n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)

la Regione Calabria è commissariata dal 2009 a causa di un elevato disavanzo sanitario e del mancato raggiungimento della soglia minima di sufficienza nella griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Nonostante questo commissariamento, il disavanzo è cresciuto ogni anno fino a raggiungere e a superare i 160 milioni nel 2019 e il punteggio della griglia LEA fino al 2019 era ancora sotto soglia.

una sanità in cui sono stati tagliati i posti letto ospedalieri e non sono state previste strutture di cure primarie e cure intermedie; una sanità in cui le assunzioni clientelari erano la regola; una sanità vittima di un alterato rapporto pubblico-privato a discapito dei cittadini calabresi, che hanno dovuto far fronte ai costi aumentati per tutte le prestazioni sanitarie; una sanità in cui per accedere a prestazioni di qualità i cittadini erano costretti a emigrare in altre Regioni, incidendo in maniera ancora più importante sul bilancio sui conti regionali, conti in rosso per assenza di bilanci - voglio ricordare come l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Reggio Calabria dal 2013 al 2017 abbia presentato bilanci orali, che non si capisce bene cosa siano cosa siano - e per forniture pagate a costi altissimi con le stesse fatture liquidate più volte; una sanità vittima di gestioni manageriali poco oculate, per non dire incompetenti. Certamente, senatore Mangialavori, non è colpa dei cittadini calabresi, che sono vittime di questo sistema. Nel 2019, però, per la prima volta lo Stato è intervenuto a tutela dei cittadini calabresi, per i quali fino ad allora non era stato garantito un diritto fondamentale come quello sancito dall'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute. Il primo decreto a favore della Regione Calabria è scaduto però il 3 novembre scorso, eppure tutte le criticità perdurano. Per questo c'è la necessità di un nuovo intervento normativo a favore della Calabria, un nuovo decreto-legge con durata biennale biennale (o ridotta rispetto ai due anni, qualora vengano raggiunti in anticipo tutti gli obiettivi previsti). Questo nuovo decreto attribuisce al commissario *ad acta* individuato nel prefetto Guido Longo - cui tutti facciamo gli auguri di buon lavoro - poteri e mezzi straordinari e mette in campo risorse importanti per raggiungere finalmente la soglia di sufficienza nei livelli essenziali di assistenza. I punti focali di questa norma sono diversi e ne riprendo solo alcuni. Innanzitutto, il rafforzamento della struttura commissariale

Prevede l'assunzione straordinaria di personale sanitario in deroga ai limiti di spesa, fino a 12 milioni di euro per ciascun anno, attingendo innanzitutto alle graduatorie di idonei e stabilizzando i precari. La norma prevede per la prima volta la verifica degli esiti, dei risultati raggiunti e degli obiettivi, che verranno valutati ogni sei mesi con una relazione sullo stato di attuazione delle modifiche e delle attività dei commissari straordinari di tutti gli enti del servizio sanitario regionale.

riprendere in questa replica alcuni degli spunti che sono stati offerti dagli interventi dei miei colleghi in discussione generale. Il senatore Marinello parlava della necessità di rafforzare l'emergenza-urgenza, sia territoriale sia ospedaliera, di potenziare la medicina territoriale anche con l'istituzione dell'infermiere di famiglia; tutte misure che sono state previste anche in questi mesi per far fronte all'emergenza Covid-19. Condivido con la senatrice Granato la necessità di rivedere i criteri di nomina dei dirigenti degli enti del servizio sanitario regionale, perché abbiamo bisogno che a capo degli enti di tale servizio ci siano persone illuminate, competenti e non debitrici ai politici che le hanno nominate. Condivido con la senatrice Granato anche la necessità di rivedere il rapporto tra Stato e Regioni in ambito di sanità, rafforzando il potere di indirizzo dello Stato centrale, per garantire lo stesso diritto alle cure a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale.

riferimento alle necessità di prevedere un termine ridotto del commissariamento, vorrei sottolineare che è già previsto nella norma che la durata possa essere inferiore ai due anni nel caso in cui vengano raggiunti tutti gli obiettivi previsti. Riguardo a quanto affermato dalla senatrice Cantù, condivido l'urgenza di intervenire in maniera decisa su una riforma della formazione medica specialistica e, aggiungo, anche dei medici di medicina generale. Ricordo che il Governo ha colmato finalmente l'imbuto formativo che si era creato negli anni in cui non veniva programmata la necessità di specialisti in base al fabbisogno di salute della popolazione. Oggi invece questo avviene, anche grazie alla tecnostruttura che nella scorsa legge di bilancio abbiamo creato tra Agenas e Osservatorio delle scuole di specializzazione. Voglio però sottolineare che quanto detto dalla senatrice Cantù, e cioè che bisogna investire sul reclutamento delle giovani leve, riferendosi ai medici in formazione, non deve significare rendere costoro manovalanza a basso costo, per evitare di assumere personale nelle strutture pubbliche o private, perché per noi la qualità della formazione è al primo posto. Vorrei sollecitare l'opposizione e anche la stessa senatrice Cantù a lavorare insieme al disegno di legge n. 1519, che ormai è incardinato in Commissione sanità da più di un anno, che prevede proprio la riforma della formazione medica post laurea. Infine, riferendomi a quanto detto dalla senatrice Rizzotti, vorrei rilevare che anche io condivido l'esigenza di rafforzare la prevenzione, perché è l'arma più potente che abbiamo per passare dalla medicina di attesa a quella di iniziativa. È l'arma più potente che abbiamo, ad esempio, in ambito oncologico: se infatti i tumori vengono diagnosticati in tempo e trattati in maniera precoce, l'esito è certamente migliore.

la possibilità di accedere a diagnosi tempestive e cure innovative, senza dover emigrare per ricevere prestazioni sanitarie all'altezza degli *standard* garantiti in tutto il resto del Paese.

Normalità significa trovare un ospedale vicino casa aperto, non chiuso, come invece purtroppo si vede in molte parti d'Italia e soprattutto in Calabria; significa trovare un medico vicino; significa trovare qualcuno che ti ascolta. I calabresi hanno bisogno di questa normalità, questa normalità, che tutti auspichiamo. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi rappresenta il mezzo verso questa normalità che ognuno di noi deve volere, perché siamo italiani, ma siamo anche tutti calabresi.

Non dobbiamo però illuderci, perché è evidente che, se per undici anni di commissariamento non abbiamo ancora raggiunto il risultato e abbiamo bisogno di un ulteriore provvedimento, la strada è in salita.

quella normalità che ho detto poc'anzi, che si ottiene con il dialogo fra tutte le istituzioni locali e centrali. Infatti, quando si sbaglia, la responsabilità non è mai di uno,

che arriva in Calabria. I cittadini calabresi hanno bisogno di trasparenza e di sapere cosa accadrà per ogni singolo centesimo che esce dalle loro tasche per per lo Stato. Hanno il diritto di sapere questo: quindi, quando sento parlare di contabilità orale, chiaramente mi vengono i brividi. Queste cose non devono più accadere e chi ha sbagliato dovrà pagare, ma - si oltre a far pagare, dobbiamo vigilare e aiutare: si aiuta con il dialogo e si costruisce insieme. Vi ringrazio davvero della vostra attenzione.

Mi sia inoltre permesso di ringraziare la Regione Calabria, che sempre ieri mattina ha intitolato a suo nome il palazzo della Regione: un gesto certamente simbolico, ma necessario, per onorare la memoria di una grande presidente, di una grande donna, di una grande amica e alleata personale e della Calabria, un modello virtuoso di abnegazione e competenza, che tanto bene ha fatto alla mia terra nei pochi mesi in cui ha potuto operare. Buon compleanno, Jole, ovunque tu sia, e grazie. Tornando al tema oggetto della seduta, il destino vuole che proprio in questi giorni si parli di Calabria e che se ne debba parlare per uno degli aspetti che più ferisce il cuore di ogni cittadino calabrese, ovvero la sanità, la sanità, che versa in condizioni disperate, nonostante lo Stato ne eserciti il controllo da oltre dieci anni. Per questo motivo, la proposta di non passare all'esame degli articoli NP1 che abbiamo presentato pone all'attenzione dell'Assemblea un tema davvero serio, riguardante il rispetto di alcuni tra i più importanti principi dettati dalla nostra Costituzione. In effetti, signor Presidente, siamo ancora alla ricerca dei presupposti legislativi e costituzionali su cui il decreto-legge in esame si basa, visto che sostanzialmente non fa altro che imporre il proseguimento senza soluzione di continuità, per ulteriori due anni, degli effetti del commissariamento *ad acta* della sanità calabrese. Come già detto dai miei colleghi, di fatto sono ben undici anni che lo Stato in Calabria esercita l'intera competenza in materia di tutela della salute, quasi a renderla esclusiva, espropriando completamente la Regione di ogni funzione e potere, finanche normativo, in violazione dell'autonomia legislativa regionale. Il decreto-legge in esame prevede l'attuazione di misure speciali così pervasive per l'ordinamento di un ente regionale, quale appunto il commissariamento, che impongono necessariamente una durata delimitata nel tempo, proprio in virtù della sospensione di alcuni tra i più importanti princìpi costituzionali.

Nell'attuale decreto vengono descritte le disposizioni urgenti volte a portare avanti gli obiettivi previsti nei programmi di prosecuzione del piano di rientro. Tali interventi si configurano come provvedimenti straordinari, con i quali si intenderebbe accompagnare, come diceva anche il vice ministro Sileri, la sanità calabrese verso situazioni amministrative normali. Ora, pensare di proporre tramite un ulteriore decreto-legge il prolungamento dell'originario termine di diciotto mesi di ulteriori ventiquattro è una palese violazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della nostra Costituzione, in base al quale i diversi livelli di Governo devono cooperare fra loro. È vero, il dettato costituzionale, in alcuni specifici casi di inadempimento, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi della Regione e dei Comuni, attribuendo però a una legge ordinaria la definizione delle procedure, proprio in virtù del pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Bisogna invece constatare come nel decreto-legge in esame non vi sia alcuna traccia, né tantomeno riferimento specifico, ai criteri di cautela fissati in materia di autonomia delle Regioni. constatiamo ancora una volta che, tramite i provvedimenti straordinari, il Governo ha deciso di delegare un commissario *ad acta* e i subcommissari a gestire di fatto tutta

alle direttive governative. Questo senza tenere minimamente in conto l'evidente fallimento dello strumento commissariale, il quale in undici anni ha contribuito a peggiorare l'assistenza sanitaria in Calabria, senza ridurre il debito, che - ricordiamolo - nel 2010 è stato stimato intorno ai 150 milioni,

La Calabria, ad oggi, è una regione fanalino di coda in tutta Europa, in cui i livelli essenziali di assistenza non possono essere garantiti, come detto da tutti noi. La conseguenza di questa situazione è una mobilità passiva di 320 milioni di euro all'anno, *trend* purtroppo sempre in crescita. Coloro i quali non sono nelle condizioni economiche di potersi permettere trasferte (e ce ne sono veramente tanti), continuano invece a subire lunghe liste d'attesa per le visite specialistiche, nonché le precarie situazioni degli ospedali, talvolta non a norma e non in grado di accogliere tutti. Piuttosto che ritrovarsi a esaminare un ulteriore decreto-legge, ci si sarebbe aspettati di avviare insieme un percorso condiviso, volto a limitare, o del tutto eliminare, lo strumento del commissariamento, che al contrario è stato nel tempo irrigidito e ampliato, attraverso l'istituzione di un supercommissario, che, seppur con un *curriculum* di tutto rispetto (mi riferisco al prefetto Longo), non potrà garantire il cambiamento richiesto dai miei concittadini: il diritto alle cure nel proprio territorio. Colleghi, non dobbiamo dimenticare che, senza salute, tutto è niente. La situazione che stiamo attraversando ha contribuito a confermarlo e ci ha aperto gli occhi, facendoci comprendere che non importa chi siamo e cosa abbiamo fatto nella vita: di fronte ai problemi che riguardano la salute, siamo tutti uguali, condividiamo le stesse ansie e preoccupazioni, siamo tutti impotenti e dobbiamo totalmente affidarci nelle mani di altre persone e fidarci di un sistema, quello sanitario, che determinerà le nostre sorti. Prevedere per altri due anni il commissariamento in Calabria con la sola logica di rientro del debito, peraltro anch'esso fallito, continua a essere uno smacco, anche nei confronti del personale medico e infermieristico, che continuerà a lavorare privo dei macchinari, dei medicinali e del personale di di cui si ha necessità. Il precedente decreto è stato tanto voluto dai colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle per salvare la gestione sanitaria calabrese. In realtà,

Se in altre Regioni, in molto meno tempo, si è riusciti, tramite il sistema dei commissari, a recuperare il debito e ristrutturare la sanità, è evidente che in Calabria tale sistema non funziona. Alla luce di questi presupposti, nonché dell'evidente situazione attuale, che mostra una Regione indebitata, priva delle strutture necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza, amministrata da undici anni dai commissari imposti dai vari Governi senza alcun minimo coinvolgimento della Regione, violando con estrema noncuranza la Carta costituzionale, chiediamo di non passare all'esame degli articoli. Il commissariamento ha fallito la sua missione, condannando la mia terra a non avere un'offerta sanitaria degna di un Paese occidentale. È il momento che il Governo se ne assuma la responsabilità, che rimetta nelle mani delle istituzioni calabresi la gestione della salute dei suoi cittadini. Oltre a stimare il debito della nostra sanità, stimeremo anche il vostro nei confronti dei calabresi, che sarà irreparabile.

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

non pretenda la vostra presenza, ma la vostra attenzione sì. possa superare il commissariamento e restituire alla sua popolazione il diritto alla salute. Troppe volte la Calabria non ce l'ha fatta; ora dobbiamo farcela. Lo dobbiamo alle cittadine e ai cittadini calabresi che da anni sono costretti a spostarsi per i loro bisogni in sanità. Lo dobbiamo ai giovani e ai ricercatori, che studiano fuori dalla loro terra e devono trovare una realizzazione altrove. Lo dobbiamo anche ai professionisti della sanità che invece scelgono di rientrare in Calabria per contribuire allo sviluppo del loro territorio e portano eccellenza e qualità in quello stesso territorio (perché ce n'è molta in Calabria). Lo dobbiamo alla classe dirigente politica, sì, anche alla classe dirigente politica, a quella che vuole cambiare le cose (guai a fare di tutta l'erba un fascio). Abbiamo ripercorso la malasanità in Calabria; ora bisogna cominciare una nuova era e quindi lo dobbiamo anche ai giovani che si vogliono impegnare in politica in quella terra, alla classe dirigente amministrativa e ai sindaci. Abbiamo sentito ieri le parole del mio collega, sindaco e senatore, Magorno. Ho ricevuto anch'io, nelle settimane scorse, una delegazione di sindaci calabresi, che mi ha spezzato il cuore, portando il grido di dolore della popolazione. Lo dobbiamo a loro, ai sindaci, che sono sempre in prima linea. Questa potrebbe essere l'opportunità giusta per non trovarci, tra ventiquattro mesi, a dover rinviare ancora una volta il commissariamento e per tornare a quella normalità, che evocava poc'anzi il Vice Ministro, perché la normalità della Calabria deve essere la normalità di tutta la comunità nazionale. Intanto, per la prima volta, nel provvedimento in esame non c'è solo l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario, per il quale ci troviamo in queste condizioni, ma anche quello dell'esigibilità e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza. deputati ha rafforzato il provvedimento, prevedendo un piano assunzionale di personale medico, sanitario e socio-sanitario, affidando al commissario *ad acta* il compito di rafforzare i LEA, così calpestati anche in questa difficile emergenza da Covid-19. Facciamo della Calabria anche un esempio di ripristino delle cure primarie e della medicina territoriale, un esempio di come il sistema sanitario in Italia debba funzionare.

la preghiera di uscire, se non si ha intenzione di ascoltare o di seguire con un po' più di buon gusto e attenzione l'intervento

sono sempre e comunque in prima linea e sono i primi cittadini delle comunità territoriali. Lo Stato impegna risorse economiche

di risollevare le sorti della nostra bellissima terra calabrese, per ripartire con un futuro migliore. Per queste ragioni, il Gruppo Italia Viva voterà la fiducia sul decreto-legge Calabria.

6 milioni di abitanti ed ha ricevuto 40.000 dosi in prima battuta; non parliamo della Germania, che ne ha ricevute 150.000. Noi ne abbiamo ricevute 9.750. Peggio di noi solo la Serbia.

cellulare. Le Regioni stanno predisponendo dei piani vaccini (già lo ha fatto il Lazio, e tutte le altre Regioni vi stanno ottemperando in questi giorni), senza un quadro di riferimento nazionale, che non c'è.

tutta questa grancassa e tutto questo andare a vantarsi di non si capisce bene che cosa, o meglio andare a vantarsi di quello di cui ci si dovrebbe letteralmente vergognare, è una cosa che grida vendetta al cospetto della politica. Grida vendetta, perché l'Italia, colleghi, come voi sapete, si è macchiata di *record* scandalosi: l'Italia oggi registra il maggior numero di decessi, la maggiore caduta di PIL rispetto a tutti gli altri Paesi del mondo, del mondo, la maggiore spesa Covid rispetto a tutti gli altri Paesi europei (95 miliardi, ad oggi). Vergogna! State a casa invece che andare da Mara Venier a vantare non si capisce bene che cosa.

nel ricordare la presidente Santelli; è assolutamente apprezzabile lo spirito, ma sarebbe necessaria maggiore coerenza, visto che certi bizzarri personaggi ancora si aggirano nei meandri delle istituzioni e nessuno ha provveduto a convincerli che sarebbe meglio restituire decoro a quelle istituzioni che invece ancora bazzicano, e sarebbe opportuno che smettessero di farlo.

con due criteri: il debito e la griglia della somministrazione dei LEA. Ad oggi, questi due criteri non sono solo peggiorati, ma sono notevolmente peggiorati. Con riguardo

Ciononostante, avete lasciato cadere il primo decreto, forse perché anche voi vi vergognate di quello che scrivete e forse alla fine un po' di pudore ce l'avete anche voi. quel primo decreto che discutemmo in quest'Aula, quando noi anticipammo che non avrebbe prodotto nulla (come nulla ha prodotto), l'avete lasciato decadere i primi giorni di novembre.

A che cosa serve una gestione regionale senza la sanità da undici anni? Con quale criterio richiamiamo alle urne gli elettori (quando finalmente deciderete di farlo) quando lo Stato espropria, con un banale decreto, o meglio con il susseguirsi di banali decreti convertiti, letteralmente il 70-80 per cento del bilancio di una Regione? A che serve quell'amministrazione regionale? La storia di questi commissariamenti, peraltro, è assolutamente paradossale. C'è una transumanza sanitaria - perché di questo bisogna parlare, non di mobilità, perché voi trattate i calabresi come pecore

che era uno dei motivi per commissariare, è peggiorata. Oggi in Calabria si vive mediamente cinque anni in meno rispetto alle Regioni del Nord come Lombardia e Veneto. Cinque anni.

con la reiterazione di provvedimenti che non hanno alcuna logica e alcuna natura se non quella di espropriare una Regione, oggi a maggior ragione perché è governata dal centrodestra, dell'80 per cento del proprio bilancio.

voglio concludere con la parola «vergogna», elencando i nomi che ci avete propinato in questo valzer di candidati che avete speso a beneficio dei giornali: Cotticelli, Zuccatelli, Varratta, Gaudio, Strada, Mostarda, Miozzo e, *dulcis in fundo,* Rosy Bindi. Questo siete voi. Vi

credo che, con onestà intellettuale, sia giusto riconoscere che dieci anni di commissariamento non hanno prodotto alcun risultato positivo. risultato positivo. Va bene scagliare le prime pietre, però, come sapete, il percorso di questi dieci anni ha visto diversi protagonisti, da una parte e dall'altra. È, tuttavia, altrettanto sbagliato non vedere che la situazione attuale della Calabria, senza bilanci, in una situazione di gravissima emergenza sanitaria pre-Covid, richiede un intervento straordinario.

darsi due obiettivi: il primo, superare assolutamente il commissariamento entro i prossimi due anni; il secondo, provare a condividere, le diverse forze politiche, una strategia per raggiungere questo obiettivo. Sono tre le condizioni, a mio parere, che il decreto risorse; dopodiché, la necessità di costruire una squadra. Nemmeno Nembo Kid da solo sarebbe in grado di governare e risolvere i problemi della Calabria; ci vuole una squadra di tecnici, di professionisti, di competenze. Da questo punto di vista spero che Agenas sia in grado di mettere a disposizione del commissario le migliori competenze italiane per costruire un piano di fuoriuscita dal commissariamento nei prossimi due anni. Ci vogliono competenze. Insieme alla Regione Calabria - voglio ricordare anch'io Jole Santelli perché sono certo che lei lo avrebbe fatto - bisogna costruire le competenze della Regione Calabria per gestire la sanità. Quelle competenze che, purtroppo, per le ragioni che conosciamo, oggi non sono a disposizione.

Mi piacerebbe che da questo punto di vista vi fosse la possibilità di discutere tra le diverse forze politiche il piano di rientro, di discuterne con i cittadini calabresi e di fare in modo che questo piano diventasse parte importante del salto di qualità della Calabria: un piano per la Calabria, della Calabria. dall'alto, senza un sistema partecipativo, il problema della Calabria non si risolverà; bisogna esserne consapevoli. Lo dico anche al Governo e alla maggioranza: se non coinvolgiamo la Calabria, ogni obiettivo, anche il più giusto, rischia di non essere realizzabile.

ma sono necessarie alcune riflessioni complessive. Io penso che occorra prendere definitivamente

diversamente, anche le assunzioni straordinarie del piano Covid non potranno essere realizzate. Io prego il Governo davvero di fare questa scelta al più presto. In secondo basta con la fase ragionieristica della sanità. Il problema della Calabria (e non solo della Calabria) non è solo il *deficit* di bilancio. Il primo problema della Calabria è che non ci sono i livelli essenziali di assistenza e non si può avere un atteggiamento che cominci dalla dalla parte sbagliata, cioè dalle risorse. Prima di tutto dobbiamo costruire un sistema che sia in grado di assicurare i livelli essenziali

ma non abbiamo direttori sanitari, non abbiamo direttori d'azienda, non li forniamo, non c'è una consapevolezza, non c'è una formazione sui medici di medicina generale.

senza una riorganizzazione del sistema, utilizzando le nuove tecnologie, come la telemedicina, non andremo da nessuna parte, nemmeno dopo il Covid.

e poi i cittadini di quelle Regioni vanno a curarsi in Lombardia, in Emilia-Romagna o in altre Regioni. Capite quanto sia assurdo. l'idea che io vi propongo è quella di pensare ad una riforma complessiva del sistema.

a partire da un punto. Abbiamo visto la complessità, la criticità del rapporto tra Stato e Regioni; avremo modo di discutere della riforma del Titolo V, sul quale certamente bisogna intervenire, ma facciamo una riforma

ci troveremmo sempre di fronte alle contraddizioni che abbiamo incontrato in questi mesi. La ragione per cui ci troviamo all'interno di questa dinamica

Regioni a dover occuparsi della gestione. Proviamo a fare questo sforzo insieme con tutto il Parlamento. Ho già proposto di fare un momento di riflessione sulla sanità in quest'Aula. Facciamola questa riflessione riflessione in modo tale da misurarci anche rispetto alle diverse posizioni tra maggioranza e opposizione e tra le diverse forze politiche. Costruiamo questo momento di riflessione perché la sanità, a volte, è come il calcio: ciascuno fa la sua formazione, ma la sanità prima di tutto è competenza e noi dobbiamo dimostrare di avere competenza per avviare la discussione e riformare, come è necessario, la sanità nel nostro Paese. Senatore Errani, ho ascoltato con attenzione il suo intervento. Se mi consente una battuta, per quelli della nostra generazione è chiaro chi è Nembo Kid, ma sotto i

l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, di cui oggi ci occupiamo, reca misure di natura eccezionale ovviamente e, dunque, con vigenza limitata nel tempo per la gestione commissariale del sistema sanitario della Regione Calabria.

riorganizzare, rendendo ovviamente impossibile vedere riconosciuti i diritti garantiti dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Il contesto generale della Regione Calabria mette in luce un sistema sanitario anche se sottoposto - come dicevo - da tanti anni a piani di rientro, presenta ancora una grave situazione e, addirittura, un peggioramento di alcuni indicatori, una mancanza di assistenza territoriale, con conseguente aumento di tassi di ospedalizzazione, del numero delle indisponibilità di posti letto, degli ospedali che ancora non sono stati che sono inefficienti. Tante risorse non si sono mai spese. In questi anni si sono accumulati ritardi e con questo decreto si vogliono creare le condizioni per poter spendere tali risorse nel modo più veloce ed efficace possibile. Per questo le disposizioni degli articoli dall'1 al 7 del decreto sono È necessario rimettere ordine a questo disordine amministrativo e gestionale, che ha messo in evidenza casi di sovrapposizione di interesse della criminalità che giustificano un intervento straordinario e rendono necessario un intervento verso una discontinuità immediata affinché vengano garantiti quei famosi livelli essenziali di assistenza anche per i cittadini calabri. Oggi, quindi, in assenza di altri strumenti giuridici - ricordo che l'altro decreto ha terminato la sua efficacia perché durava diciotto mesi - siamo di fronte a uno stato di necessità, che è considerato dagli indirizzi del decreto con un rafforzamento

Calabria, ad assicurare l'adempimento dei livelli essenziali, il rafforzamento strutturale della rete ospedaliera, delle emergenze-urgenze e anche delle infrastrutture di posti di terapia intensiva e subintensiva.

un uomo che ha fatto della lotta alla criminalità organizzata la sua missione e nel quale riponiamo non solo la massima fiducia, ma anche la gratitudine per non essersi sottratto ad un impegno così gravoso. Speriamo possa avvalersi di collaboratori capaci e di subcommissari competenti, che sappiano cosa significa parlare di *management* sanitario, di regole della pubblica amministrazione e anche di indirizzi del Ministero. L'obiettivo che sottende al provvedimento in esame è quello di rafforzare un percorso finalizzato a una prima rimozione dei principali fattori di criticità, dotando il commissario *ad acta* di poteri straordinari che consentano tempi certi tempi certi e definiti e il ripristino di quella normalità amministrativa e gestionale di cui ha parlato anche prima il vice ministro Sileri, garantendo la trasparenza nel settore sanitario e superando quindi gli ostacoli burocratici e ambientali. Il commissario *ad acta* nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi del corpo della Guardia di finanza, anche per contrastare le violazioni o il pregiudizio degli interessi economici e finanziari. La centralità sta comunque in capo al Ministero della salute e sono molti i vincoli che doverosamente sono stati introdotti, affinché non ci sia mai un vuoto di responsabilità.

opache e dalla collusione del passato finalmente con questo decreto si possa incanalare la sanità calabrese in una condizione di normalità, quella normalità che vuol dire riconoscimento di un'azione di investimenti nel campo della salute attraverso risorse umane, strutture e sistemi tecnologici, che non significa investire solo nel campo della sanità, ma

L'auspicio è di iniziare bene, facendo in modo che tutti si sentano coinvolti in una collegialità e in una missione che non può fallire, perché questa non è una sfida solo calabrese, ma di tutta l'Italia. Dobbiamo recuperare la fiducia nelle istituzioni, che per molti calabresi ormai è persa da anni.

mi chiedo per quanto tempo questo Esecutivo continuerà a fare scelte sulla pelle dei cittadini. La Calabria è di gran lunga la Regione italiana con il peggiore sistema sanitario. Durante questi anni di commissariamento sono stati pesantissimi i tagli dei posti letto (diminuiti del 40 per cento fra il 2000 e il 2013) e del personale sanitario (meno 17 per cento tra medici, infermieri e operatori sanitari fra il 2010 e il 2017). In Calabria mancano i medici, gli infermieri, gli operatori, ma anche le ambulanze, i consultori, gli studi medici e questo i cittadini calabresi lo sanno bene. infatti, come ricordava il vice ministro Sileri, un cittadino su cinque si è spostato in altre Regioni italiane per il ricovero ospedaliero. La sezione di controllo della Corte dei conti ha parlato di collasso della sanità calabrese per evidenziare che nel sistema sanitario niente va bene. Si è parlato di patologia della sanità proprio perché negli ultimi undici anni di commissariamento il *deficit* sanitario della Regione è stato ridotto di soli 6,2 milioni di euro. Pensate che sono stati i cittadini calabresi che, attraverso sacrifici finanziari, con il versamento dei tributi dell'Irpef e dell'IRAP, hanno contribuito alla riduzione del debito.

Pensate che gli anni di vita in buona salute dei cittadini calabresi è in media pari a 52 anni, contro i 67,7 dei cittadini che vivono in Trentino-Alto Adige. Questo è inaccettabile e nonostante il quadro molto preoccupante, in data 4 novembre, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Conte e del ministro Speranza, ha approvato il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare. Nonostante ci troviamo di fronte ad un esempio lampante di malasanità, essenziali di assistenza al di sotto della soglia di sufficienza, che non garantiscono ai cittadini il diritto alla salute, la proposta è quella di continuare con il fallimento, con il fallimentare sistema per non risolvere l'annoso e preoccupante problema. problema. Il totale fallimento della gestione commissariale è palese, anche se il decreto prevede il rafforzamento dei poteri del commissario *ad acta*, con l'incarico di attuare i programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro del Servizio sanitario regionale. Tutto questo naturalmente per conseguire l'obiettivo del riequilibrio finanziario, economico e contabile. Noi naturalmente facciamo il nostro augurio all'ex prefetto, dottor Longo, al lavoro a Catanzaro, in cui il piano Covid è la priorità. Ascoltiamo però anche le parole di Gino Strada, fondatore di Emergency, che dice che per la sanità calabrese servirebbe una vera e propria rivoluzione. Il problema della Regione Calabria è strutturale. Va modificato il sistema, dando più potere alla Regione e non a *task force* o commissari *(Applausi),* inviati dal Governo per tamponare la situazione, concessioni disastrose che non fanno altro che indebitare ancora di più la sanità pubblica e la Regione stessa. I calabresi devono recuperare fiducia nel loro sistema sanitario, iniziando dalla formazione, come proposto dall'emendamento 6.0.1, della collega Cantù, trasformato in Commissione sanità in un ordine del giorno, approvato da tutto il centrodestra. ripensare il sistema delle specializzazioni per contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi, con formazione e praticantato, *teaching hospital* e telemedicina sotto la guida di *tutor senior* riconosciuti dal Consiglio della scuola di specializzazione. Occorrerebbe estendere il modello alle specializzazioni afferenti a tutte le professioni delle dirigenze sanitarie, biologi, farmacisti, odontoiatri, veterinari, fisici e chimici. Tutto questo allo scopo di non trovarsi più in mancanza di materiale umano formato e qualificato. In un mondo che va molto veloce e che purtroppo viene anche travolto da eventi epocali, come la pandemia che stiamo vivendo, non possiamo permetterci di imporre delle limitazioni specie nel campo della sanità. È impensabile che proprio in campo sanitario ci siano situazioni poco chiare e non corrispondenti alle stesse esigenze. Mi riferisco, ad esempio, all'aggiornamento dell'Albo nazionale dei direttori generali delle aziende sanitarie, che viene aggiornato ogni due anni. Un'enormità di tempo in relazione al momento che stiamo vivendo. La possibilità di un aggiornamento con scadenza annuale rappresenterebbe l'esigenza di molte realtà, compresa quella sarda, con la possibilità di inserire nuove risorse indispensabili per il rilancio del Sistema sanitario nazionale, specie in quelle Regioni più fragili come la Calabria che, dopo il periodo del commissariamento *ad acta*, avrà la necessità di poter scegliere qualificati *manager* a cui affidare la guida delle Aziende sanitarie regionali. Queste sono solo alcune delle proposte migliorative che noi avremmo voluto che fossero ascoltate. membri del Governo, ogni vostro atto è caratterizzato da interventi fumosi, con decreti-legge che si trasformano in scatole vuote, lontani anni luce dai reali problemi. Anche in questo caso si vorrebbe cambiare qualcosa, senza cambiare nulla e perseverando su un modello fallimentare, a spese del popolo calabro che si trova, ancora una volta, a pagare sulla propria pelle la malasanità

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi senatori, l'anno che sta per terminare ha messo a dura prova il mondo intero, stravolgendo le abitudini di ciascun uomo e i progetti di ogni Paese. Il 2020 è l'anno dove è accaduto l'imponderabile: un virus instancabile ha distanziato fisicamente le persone e reso invalicabili i confini geografici di ogni singolo Paese, sollevando barriere invisibili; ha provocato la più grave crisi economica globale dal Dopoguerra ad oggi e portato la Cina a essere la più grande potenza economica mondiale in tempi *record*. È l'anno in cui il sistema sanitario di ogni singolo Paese è stato messo in crisi e ha visto perdere la vita di milioni di nostri concittadini, colleghi medici, infermieri, operatori e tecnici sanitari, a cui vanno il nostro sentito pensiero e ringraziamento.

il 2020 sarà ricordato anche dei calabresi come l'anno in cui lo Stato, per il tramite del Governo, ha decretato la Calabria figlia di nessuno e orfana di Stato. i calabresi si sentono figli di un dio minore. Questo accade proprio mentre l'Europa, considerata grande, gigante, distante e fredda rispetto alle esigenze dei cittadini europei, sotto continui *input* politici - anche da parte del nostro *leader* Silvio Berlusconi e del vice presidente del Partito popolare europeo Antonio Tajani - riesce a dare, nel momento più difficile della sua storia, attraverso il Vax-day, il giorno della vaccinazione, una grande lezione di solidarietà, unione, speranza, vita e rispetto verso ogni singolo cittadino europeo di fronte al diritto alla salute: esattamente ciò che i calabresi chiedono da undici anni e che il Governo oggi non vuole riconoscere e dare.

Tajani, che ha presentato la proposta per la realizzazione di una vera Unione europea della salute attraverso la creazione di un istituto europeo per la ricerca,

Per tornare al decreto Calabria, vorrei sapere con quale logica state riproponendo un decreto che ha dimostrato il suo completo fallimento, anche attraverso le diverse televisioni un decreto che non è altro che la proroga dello strumento commissariale che tanto stiamo criticando e che continuiamo a criticare anche in quest'Aula, dai banchi della maggioranza, ma che viene confermato.

Calabria. Sono certo che almeno questa passeggiata quest'anno sarà evitata. Stiamo parlando di quel decreto Calabria che in due anni ha portato 21 indicatori che misurano l'efficienza sanitaria di una Regione a registrare valori talmente scarsi che, nonostante la Calabria forse la Regione con meno contagi e meno morti da Covid, ha subito l'umiliazione di essere decretata zona rossa per l'incapacità e l'impossibilità di assistere i malati calabresi. Parliamo di quel decreto Calabria che non piace nemmeno agli esperti in materia sanitaria, chiamati dal *premier* Conte per essere nominati commissari che, una volta letto il decreto Calabria, sono stati costretti a rinunciare a quell'incarico, e abbiamo dovuto assistere ai balletti per la nomina del commissario. *(Applausi)*. Colleghi, quello che non riesco a spiegarmi, inoltre, è come sia possibile che in nove mesi cambia il mondo; cambia la storia del mondo e dei singoli Paesi; cambia anche la storia dell'Europa, che improvvisamente si materializza e riesce a mettere d'accordo 27 Paesi membri di storie e di culture diverse, con 24 lingue diverse parlate al Parlamento europeo, per tutelare 446 milioni di cittadini europei, mentre questo Paese, che conosce benissimo le problematiche di un territorio difficile e complesso, non si è impegnato in due anni a trovare una vera soluzione per risolvere l'emergenza sanitaria e il diritto alla alla salute dei calabresi. *(Applausi)*. Non riesco a capacitarmene. Eppure nel piccolo, nella quotidianità, un imprenditore - anche una famiglia, ma soprattutto parliamo di aziende e quindi di impresa di impresa - per fare delle valutazioni anche strategiche rispetto alle decisioni da prendere, valuta lo storico degli ultimi due anni di attività di un'azienda; valuta l'efficacia della *governance*; valuta le scelte strategiche fatte negli ultimi anni e quelle da fare negli anni successivi

che invece ha la responsabilità di garantire i diritti sanciti dalla Costituzione, e soprattutto il diritto alla salute, che è l'unico diritto affiancato dall'aggettivo «fondamentale» (articolo 32 della Costituzione), non si sia impegnato - per me il dibattito politico, il confronto non c'è stato né in Commissione, né in quest'Aula, perché c'è la maggioranza - e non abbia voluto trovare il confronto per garantire il diritto alla salute in Calabria,

Stiamo parlando di undici anni di aumento di addizionali regionali a carico dei cittadini calabresi, che pagano le tasse per finanziare il servizio sanitario regionale, che però non garantisce assistenza sanitaria. anni di aumento della migrazione sanitaria obbligata per quei calabresi che sono costretti a curarsi altrove perché non trovano assistenza in Calabria; undici anni di disavanzo gestionale provocato dai commissari, undici anni in cui lo Stato non ha mai messo in ordine i conti e, quindi, la responsabilità non è dei calabresi: sono i commissari che non hanno mai presentato i bilanci in questi undici anni, non i calabresi. anni che hanno creato la mancanza di 1.400 medici e 2.800 operatori sanitari; undici anni di ingiustizia sanitaria; undici anni di occupazione del nostro diritto alla salute. Questo salute. Questo decreto non funzionava, non funziona e non funzionerà. Il Governo vuole convincere i calabresi che si sta andando nella direzione giusta, ma i calabresi hanno compreso, oramai, che si trova sullo stesso *tapis roulant* di undici anni fa: dice di andare avanti, ma rimane sempre fermo. Non ha mai tracciato la rotta da seguire veramente per raggiungere il traguardo tanto atteso dalla Calabria. Questo decreto rappresenta non una cura per la sanità calabrese, ma un palliativo per distrarre i cittadini dal loro dolore, provocato dall'assenza dello Stato. In ultimo, per quanto riguarda il decreto Calabria, saluto con stima il dottore Longo, servitore dello Stato che - permettetemi di dirlo - meriterebbe una medaglia solo per avere accettato l'incarico. Essendo un uomo dello Stato, con grande senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni ha detto sì a Conte, sicuramente con la volontà di fare del bene alla Calabria. Come sapete, ho sostenuto che il commissario deve essere un esperto in *management* e programmazione sanitaria, per riorganizzare il settore ospedaliero, la medicina generale del territorio, l'assistenza domiciliare integrata, la telemedicina. La nostra difesa del diritto alla salute non inizia oggi, ma è iniziata già nel 2018. Il 5 giugno di quell'anno, in quest'Aula, in occasione della presentazione del Governo, abbiamo chiesto

Lo abbiamo chiesto anche il 18 giugno di quell'anno, con la prima manifestazione organizzata a piazza Montecitorio a Roma, alla quale hanno partecipato cittadini calabresi, medici e operatori sanitari. Adesso siamo delusi anche noi parlamentari calabresi per l'ennesima occasione persa da questo Governo. Da ultimo, il vostro piano vaccinale non funziona e non funzionerà, perché, se si vuole vaccinare - come da voi annunciato - l'80 per cento della popolazione italiana entro l'inizio del nuovo anno scolastico, cioè entro settembre, significa che occorrono 110 milioni di vaccini per 50 milioni di cittadini italiani. In nove mesi, da oggi a settembre, occorre inoculare vaccini a 400.000 persone al giorno per duecentosettanta giorni. In sostanza, servono 400.000 vaccini al giorno e non 400.000 vaccini a settimana. A proposito di decreto Calabria e del piano vaccinale, considerando che i 21 parametri che misurano l'efficienza della qualità dell'assistenza sanitaria hanno dato esito completamente negativo, significa che nel piano vaccinale deve essere data priorità alla Calabria, perché i cittadini non hanno le strutture dove curarsi e non possono subire l'ennesima umiliazione decretando la zona rossa.

e i cittadini calabresi stanno pagando da anni gli errori di chi li ha amministrati. Senza andare lontano, vi leggo alcuni stralci della relazione redatta dal magistrato Stefania Anna Dorigo, in occasione della teleconferenza della Corte dei conti sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria. Per l'esercizio finanziario 2019, il *deficit* sanitario cui dare copertura si è ridotto, in valore assoluto, di soli 6,291 milioni di euro, passando da oltre 104 milioni, al 31 dicembre 2009, a 98 milioni al 31 Gli abitanti della Calabria stanno da dieci anni colmando una voragine finanziaria che cresce e si alimenta di anno in anno. A fronte di sacrifici finanziari, però, i medesimi cittadini non godono però di servizi sanitari adeguati. Rammento - ha ricordato Dorigo - che i livelli essenziali assistenziali sono giudicati adeguati quando raggiungono un punteggio di 160 o un livello compreso fra 140 e 170 in assenza di criticità. Ebbene, dopo molti anni, solo nel 2018 la Regione Calabria parrebbe aver raggiunto un punteggio complessivo adeguato di 162, che comunque tradisce ancora numerose anomalie, come *screening* oncologici inadeguati e scarsità di posti letto. La sanità in Calabria continua a essere una vera e propria voragine e i commissari che si sono succeduti, i quali - è bene ricordarlo - erano stati chiamati quale compito originario a risanare proprio gli aspetti finanziari del settore, malgrado diciotto ospedali chiusi, blocco del *turnover* e tagli indiscriminati, non hanno raggiunto alcun obiettivo significativo, consegnando all'emergenza pandemica del coronavirus una sanità che era già in terapia intensiva. Ecco perché la Calabria è finita in zona rossa. La gestione anomala della sanità calabrese per la Corte dei conti risiede nella gestione dei contenziosi.

(complessivamente oltre 55 milioni di euro) avrebbero potuto essere destinate a incrementare prestazioni sanitarie piuttosto che - come purtroppo è avvenuto - a compensare i creditori per il ritardo nel pagamento dei loro crediti. E questo solo per quanto attiene alla mala gestione. Ma c'è molto altro: due ASP commissariate per infiltrazioni mafiose, quella di Catanzaro e quella di Reggio Calabria, e un'inchiesta che ha portato ad arresti nei vertici dell'azienda ospedaliera di Cosenza, con accuse di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e abuso d'ufficio. Il decreto di scioglimento dell'ASP reggina parla di presenza di parenti di personaggi di spicco della malavita organizzata, pregiudicati con incarichi nella stessa azienda; mancanza di procedimenti regolari nell'affidamento di appalti e lavori; mancata vigilanza sul patrimonio immobiliare: un elenco lungo e dettagliato di ipotesi di reato, che rivela una situazione molto compromessa, che ha portato al commissariamento dell'ente. Nelle intercettazioni in merito all'azienda ospedaliera di Cosenza si parla invece di una tangente da centinaia di migliaia di euro della Coopservice. Dalle indagini emergono oltre 177.000 ore di lavoro retribuite e mai effettuate, a fronte di ore reali effettuate inferiori anche alle 132.000 minime annue previste dal capitolato di appalto. Poi abbiamo il presidente del Consiglio regionale della Calabria Tallini, coinvolto nell'inchiesta sul *business* dei farmaci della cosca Grande Aracri di Cutro. Tallini è stato posto agli arresti domiciliari, accusato dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso. Secondo l'accusa, i rapporti di Tallini con la cosca Grande Aracri avrebbero riguardato la costituzione di una società con base a Catanzaro finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie. Tallini avrebbe fornito supporto alla cosca, specie nelle varie fasi di avvio del progetto, e il suo intervento sarebbe stato ricambiato anche con il sostegno della cosca alle elezioni regionali del 2014. Il contributo del politico sarebbe stato decisivo per favorire e accelerare l'*iter* burocratico iniziale per ottenere le necessarie autorizzazioni per la costituzione della società per la distribuzione di medicinali. E mi sono limitata solo alla cronaca degli ultimi mesi. Quanto ci vorrà per rimediare a tutto questo sfacelo? Non poco. Non sono bastati gli ultimi diciotto mesi di commissariamento precedente e i poteri dati. Quindi, c'è bisogno di altro tempo e di ulteriori strumenti, che mettiamo a disposizione in questo decreto-legge. Il neocommissario Longo avrà molto da fare ed è partito con il piede giusto; ha già messo in luce annosi problemi e disordine contabile, economico e finanziario. Mancano i documenti relativi all'adozione dei bilanci: quello del 2018 per l'ASP di Cosenza e addirittura dal 2013 al 2017 per quella di Reggio Calabria. Calabria. Vorrei ricordare al senatore Siclari che tale mancanza attiene ai direttori generali di quella ASP e non al commissario nominato dal Governo. È la stessa ASP di Reggio Calabria il vero buco nero della sanità calabrese il neocommissario ha chiesto dettagliate relazioni su queste carenze, da produrre in tempi brevissimi, con documenti scritti e non con relazioni orali. I cittadini calabresi meritano di più: meritano ospedali funzionanti e puliti, forniti di tutto il necessario e di personale in numero adeguato. Il personale sanitario merita di lavorare nelle giuste condizioni, per poter svolgere attività così importanti e delicate. I malati meritano di trovare risposte e cure vicino casa, senza bisogno di dover migrare lontano. Con il decreto-legge in esame facciamo un passo in avanti e forniamo strumenti affinché tutto quello che a un un abitante di Bologna sembra normale da domani sia normale anche per un cittadino di Crotone. La cattiva gestione - per non dire altro - è però così diffusa e radicata che un uomo solo, un Longo, potrebbe non bastare. C'è bisogno che i calabresi onesti, che sono una maggioranza silenziosa, facciano squadra insieme a lui e si ribellino finalmente a quello che sembra un destino ineluttabile. Noi, da parte nostra, facciamo tutto il possibile, anche votando a favore del provvedimento Voi ricordate chi ha ridotto in questo stato la vostra sanità! Il MoVimento 5 Stelle, da quando è al Governo, ha invertito la rotta dei tagli che si sono susseguiti negli anni, e non solo,

ad adottare un piano di assunzioni straordinario di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza e urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, con una spesa di 12 milioni di euro, a decorrere dal 2021. Oggi tutti si riempiono la bocca parlando di risorse da dare alla sanità, ma abbiamo visto che negli ultimi dieci anni i Governi che si sono succeduti hanno tagliato circa 37 miliardi di euro. Alla sanità serve non propaganda, ma politiche di investimento, programmazione e garanzia dei servizi che arriveranno ai cittadini, attraverso il potenziamento della medicina territoriale, attraverso il potenziamento del pubblico e una gestione che certamente non può essere a velocità diverse, come abbiamo visto anche in questi mesi; motivo per cui il prossimo passo sarà ripensare il Titolo V della Costituzione, per poter dare finalmente a ogni cittadino italiano le stesse possibilità di cura.

perché vi meravigliate? Non è neanche una novità assoluta. PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, è il dissenso che dà fastidio e lo capisco. Colleghi, avete parlato di eccellenze sanitarie e ospedaliere in Calabria... Avete sottolineato il sacrosanto diritto dei cittadini calabresi a godere pienamente del diritto costituzionale alla salute. Ma poi, quando si è trattato di nominare l'ennesimo commissario, avete dato dimostrazione di tutto il vostro stato confusionale. Non mi metto qui a ricordare che razza di bestiario - per usare un'espressione cara a Giampaolo Pansa avete messo in campo e il ritardo con cui poi l'avete rimosso. Non è solo questo, però, il punto. Parlate di rilancio della sanità e delle professionalità, ma qual è il profilo del commissario scelto? Si tratta Quindi, ricapitoliamo: a governare la sanità calabrese con i poteri del commissario c'è un poliziotto; a guidare la Banca popolare di Bari avete messo un super-poliziotto, Giovanni De Gennaro; le tensioni all'interno della maggioranza riguardano il controllo dei servizi segreti ed è per questo che siete intolleranti al dissenso. Vorrei dunque capire se pensate di schierare l'Esercito quando i cittadini vorranno difendere i loro diritti; se lo schiererete contro chi difenderà il lavoro, contro chi chiederà di non dover chiudere le proprie attività, contro chi chiederà anche di conoscere la verità sulle vostre responsabilità in tema Covid. Infine, voglio capire se schiererete l'Esercito contro chi si opporrà all'ennesimo vaccino obbligatorio, perché voi volete il vaccino obbligatorio per fare l'ennesimo regalo alle multinazionali del farmaco. Vi ricordo che nel buco nero della Calabria ci sono anche le creste fatte per pagare due o tre volte i prodotti sanitari. La Calabria ha bisogno di non chiudere gli ospedali e ha bisogno di più sanità pubblica, ma con quali soldi lo volete fare se state dentro il sistema sistema contabile dell'Europa? Italexit quindi vota contro questo vostro decreto-legge che sta ancora dietro la logica contabile e, soprattutto, umilia i professionisti seri e preparati che ci sono in Calabria, professionisti che si dovranno misurare con un commissario ex questore.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Non è una tombola natalizia, ma quasi. *(È estratto a sorte il

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore

Vanin

dei voti).* Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2045, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge 150. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 13,30 con la discussione del disegno di legge di bilancio. *(La seduta, sospesa

anziché oltre 300, sarebbe stata la stessa cosa: non ci sarebbe stato il tempo di discuterli né tantomeno di valutarli, non certo per una mancanza da parte dell'opposizione del cosiddetto clima costruttivo, ma semplicemente perché è la prima volta, come ho ricordato anche ieri, che la manovra economica è arrivata

quadra. Immagino gli interventi dell'attuale sottosegretario, senatore Misiani, gli strali del capogruppo Marcucci e degli altri esponenti dell'attuale maggioranza sull'inadeguatezza

ai progetti e alle risorse che l'Europa ci dà, perché, se non siamo capaci di fare una manovra di bilancio, dubito seriamente si possa pensare di progettare

e tutti possano sapere effettivamente cosa sta accadendo in Parlamento, ma soprattutto come sta operando questo Governo.

preciso che non sta alla Presidenza esprimersi nel merito dei contenuti specifici dei singoli provvedimenti, rispetto ai quali, naturalmente, il Governo si assume ogni responsabilità, anche nei rapporti con il Parlamento. rispetto ai futuri provvedimenti di iniziativa governativa - che sta anch'essa nelle cose - ogni valutazione sarà svolta nelle forme e nelle sedi appropriate. Naturalmente, come noto, il Governo potrà intervenire nel corso della seduta e anche all'esito della discussione generale.

qui presente il vice ministro Misiani, che è responsabile dell'Economia, chiediamo che sia lui a darci una risposta. È evidente. Non può liquidare un fatto così grave con un intervento da parte sua, che non chiarisce alcunché.

quindi rimane nella facoltà del Governo interloquire e rispondere. *(Commenti)*. Mi sembra di essere stata estremamente chiara: chiara: il Governo avrà la facoltà di intervenire quando lo riterrà opportuno.

un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Ecco, quest'oggi, leggendo il testo del disegno di legge di bilancio, che, peraltro, ci è stato sottoposto in modo frettoloso, abbiamo avuto la prova, ma soprattutto l'hanno avuta gli italiani, sui quali ricadranno i suoi effetti: il testo non ha più alcuna linea politica tesa alla crescita del Paese né una sua visione futura. Ancora, abbiamo avuto la prova dell'incapacità del Governo di gestire la grave crisi pandemica sia sul piano sanitario sia gettando il Paese in un evidente squilibrio sociale, spaccandolo a metà, affossando interi comparti produttivi, con misure che, nonostante le nostre continue grida d'allarme dei mesi scorsi, rimaste colpevolmente inascoltate, sono risultate del tutto insufficienti, perché fondate su un principio di mero assistenzialismo, assolutamente improduttivo e inefficace. D'altronde, cosa potevamo aspettarci da un Governo il cui partito di maggioranza relativa ha approvato la più grande misura assistenziale indiscriminata che il nostro Paese abbia mai visto e i cui risultati sono ormai sotto gli occhi di tutti? Hanno purtroppo dimostrato il suo completo fallimento, in termini sia sociali sia economici; ormai è cronaca, sono fatti. Oggi, a causa delle scelte scriteriate del Governo e della sua maggioranza, abbiamo due Italie: quella di chi percepisce il reddito di cittadinanza e che, a causa dei ritardi e delle falle delle amministrazioni che sono state incapaci di garantire la loro ricollocazione lavorativa, alcun pregiudizio da questa pandemia, rimanendo comodamente seduto sul divano, poi in alcuni casi permettendosi anche qualche lavoretto extra in nero. è poi l'Italia del tessuto produttivo, spina dorsale di ogni Paese, che è stato fortemente compromesso, per non dire dilaniato. Penso ai ristoratori, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti, alle piccole e medie imprese, al mondo dell'imprenditoria, agli agenti di commercio, alle partite IVA in genere, che in modo fiero e dignitoso, ma allo stesso tempo con forza e tenacia, hanno chiesto al Governo una cosa semplicissima, quella su cui si fonda la nostra Repubblica: poter lavorare. Non è bastato sprecare 140 miliardi con i vari decreti-legge ristori che si sono susseguiti, il cui unico risultato è stato quello di umiliarli ancora di più,

Colleghi, siamo in pochi, ma ben rumorosi, e la collega non riesce a completare l'intervento tranquillamente, quindi vi pregherei

ormai affossate, perché impossibilitate a ripartire e con i lavoratori in mezzo alla strada, accrescendo i cinque milioni di nuovi poveri. Il disegno di legge di bilancio destina ulteriori risorse al contrasto degli effetti del Covid sulla nostra economia, ma è difficile individuare un chiaro indirizzo di crescita per l'Italia. Ancora una volta, assistiamo al riaffiorare del principio di base di questo Governo: l'assistenzialismo improduttivo. Ancora una volta, riemerge l'antico vizio di frammentare in troppi rivoli i circa 40 miliardi della manovra, che si disperdono in tanti nuovi fondi di scarso effetto moltiplicatore sulla crescita. Ora è chiaro: ciò che conta è buttare fumo negli occhi agli italiani con *bonus* e lotterie varie, che certamente non possono rappresentare le misure strutturali di cui il nostro Paese ha bisogno. Infatti, a nostro avviso, la manovra in questione non rappresenta lo sviluppo coerentemente con quanto avanzato nella Nota di aggiornamento al DEF, né nel documento programmatico di bilancio. Ad esempio, riteniamo che ben difficilmente la variazione percentuale annua del PIL 2020 possa fermarsi a meno 9 È innegabile che tale situazione sia dipesa in gran parte dell'insorgere della grave epidemia che il nostro Paese ha subito e sta continuando a subire, ma è altrettanto vero che quella attuale è conseguenza dell'improntitudine, dell'imprevidenza e dei ritardi con cui il Governo ha affrontato la prima ondata, ma soprattutto la seconda, che, a differenza della prima, era largamente prevista. Anche questa non è una semplice considerazione, ma la triste realtà. Ne è riprova il fatto che ci sono voluti tre decreti-legge per reperire risorse, con un indebitamento netto aggiuntivo di 100 miliardi di euro per affrontare la crisi economico-sanitaria, con il risultato non proprio lusinghiero che nell'Eurozona l'Italia è il Paese con il maggiore aumento del debito, terzultima nel recupero del PIL. Peggio di noi hanno fatto solo la Spagna e il Portogallo. Il nostro giudizio su questa legge di bilancio non può che essere negativo: è una manovra che vale poco meno di 40 miliardi, 23 dei quali provengono da *deficit* aggiuntivi e i restanti 17 dalle risorse del *recovery plan* europeo (sebbene, allo stato, queste siano solo previste e auspicabili). Infatti, già si parla di un nuovo scostamento di bilancio tutto caricato sul 2021, che potrebbe valere circa 20 miliardi di *deficit* aggiuntivo e si associa a un incremento annuale medio del PIL verosimilmente inferiore al 6 per cento. Ancora una volta, il Governo ha dimostrato di rincorrere il virus e i suoi effetti, non di anticiparli. Ciò che viene portato in quest'Aula è l'ennesima manovra d'emergenza; ce ne saremmo aspettati invece una di ripartenza, ma così non è stato, a causa dei pregiudizi ideologici del Governo e della sua maggioranza, fondata sull'illusione che l'assistenzialismo sia una soluzione, anziché creare lavoro, investimenti e, quindi, sviluppo. per questi motivi voteremo contro questa legge e, forse, è opportuno che il Governo, insieme al vaccino sanitario, cominci a pensare anche a quello economico. Grazie

Colleghi, si chiude un anno molto intenso, in cui il Parlamento ha lottato tenacemente per salvaguardare il proprio ruolo. Non si contano più i decreti-legge che abbiamo convertito e il denaro che abbiamo contribuito a stanziare per affrontare le conseguenze della pandemia sulla vita dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e, non ultimi, dei lavoratori. Si è trattato di manovre importanti, cui si aggiunge adesso la legge di bilancio. I numeri di cui parlerò, però, non corrispondono solo alle somme di denaro.

Un milione e mezzo di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 è la somma che viene stanziata per finanziare quella legge che da ben nove anni prevede che le detenute madri e i loro figli debbano risiedere in case-famiglia protette, per evitare che anche un solo bambino varchi la soglia del carcere. Ricordo che parliamo di bambini da zero a tre anni e, nell'ipotesi dolorosa di assenza di famiglie che possano accoglierli, la loro detenzione può arrivare fino a sei anni. tale legge più volte abbiamo invocato la completa attuazione e ora potrà dispiegare finalmente e pienamente i suoi effetti. È un primo, piccolo passo per un obiettivo irrinunciabile di civiltà. L'emergenza sanitaria ha avuto effetti drammatici nelle carceri italiane. La solitudine e l'isolamento sono stati resi ancora più duri dalla pandemia. La limitazione delle visite è stata compensata solo in parte dall'ampliamento della possibilità di comunicazione all'esterno. La sospensione delle attività formative e culturali e di molte altre a sostegno e supporto alle detenute e ai detenuti ha messo a rischio l'obiettivo del reinserimento sociale del reo, imposto dall'articolo 27 della nostra Costituzione. La tutela della salute non sempre è stata garantita appieno. Siamo in tempi di pandemia e la salute è un diritto per tutti. La concreta esperienza di vita in carcere si è davvero impoverita fino all'estremo. Troppo poco è stato fatto - lo sottolineo - per rendere più sopportabile la detenzione in questo periodo così difficile. Molto c'è da fare, a partire dalla rapida approvazione del disegno di legge sull'affettività in carcere, un testo sollecitato dai garanti per i detenuti e per il quale, come relatrice, mi batterò. Giustizia, legalità e sicurezza non possono esistere, se è violata la dignità delle persone, se è violata la dignità dei detenuti. Per questo la norma introdotta alla Camera dei deputati è così importante. Essa garantirà almeno che le madri detenute e i loro figli possano uscire dal carcere ed essere accolti in case famiglia protette. Il termine per l'adozione del decreto attuativo è di soli due mesi. Sono sicura, colleghi dei 5 Stelle, che il ministro Bonafede almeno questa volta non mi deluderà. Parliamo

Presidente, è con grave difficoltà che devo rilevare la scarsa attenzione da parte del Governo.

esame. Bisogna dire che, di fronte alla richiesta di una specificazione e di un impegno da parte del Capogruppo della Lega, presidente Romeo, vi era la necessità di una risposta immediata del Governo, dal momento che non vi era

una visione, un'indicazione che rende a chi deve investire, agli operatori economici e agli imprenditori l'immagine di un Paese nel quale potersi attivare.

vogliono andare il Paese, il Governo e la maggioranza. È solo un'indicazione di piccole cose, che possono anche essere state introdotte da un partito dell'opposizione, ma che non danno quella visione di insieme

Scusate, ma probabilmente il Governo ignora l'attività di questo Paese e quella che è stata l'indicazione negli anni del benessere - per così dire - della prima Repubblica, della Democrazia Cristiana,

- da poter utilizzare come fonte di reddito in età anziana. Qual è il risultato? Un provvedimento di blocco degli sfratti che segue quello che aveva una sua motivazione, sia pure apparente,

siamo giunti all'atto conclusivo dell'attività svolta dal Parlamento per l'anno 2020, caratterizzato dalla pandemia relativa al coronavirus. Ci Ci apprestiamo a votare una legge di bilancio per l'anno 2021 in totale assenza di democrazia. I senatori non potranno apportare modifiche attraverso gli emendamenti a causa della questione di fiducia che verrà posta e votata favorevolmente dalla maggioranza della sinistra stellata. Dissento dalle parole di una collega pronunciate nella 5a Commissione del Senato, la quale ha affermato che la democrazia è stata rispettata, in quanto gli emendamenti dei senatori sono stati inviati ai colleghi di partito della Camera dei deputati, i quali hanno potuto presentarli a loro nome.

e, come rappresentanti politici non eletti, segnalarlo ai colleghi deputati, che possono presentare gli emendamenti. Il Senato allora non serve È così? La stessa ha proseguito dicendo che è prevalso il senso di responsabilità per evitare l'esercizio provvisorio. Aggiungo che è pur vero che necessariamente, per evitare l'esercizio provvisorio, il tutto va votato entro il 31 dicembre 2020, ma non si venga a parlare di responsabilità. L'esercizio della democrazia è stato negato a una parte del Parlamento e di noi senatori. La verità è che il Governo è partito con forte ritardo - anzi, enorme - a causa delle beghe di maggioranza

partorendo un "decreto clandestini" volto a incrementare il flusso di stranieri verso la nostra Italia per foraggiare la mangiatoia delle cooperative impegnate con l'accoglienza. Ma quale democrazia! D'altra parte, cosa ci si poteva aspettare? I presupposti c'erano tutti. Dove è il ministro Lamorgese, assente quando qui è stato discusso e convertito il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza? Voi della maggioranza avete inghiottito la democrazia per dare la priorità all'immigrazione. Anche il presidente Pesco, poco fa, in Commissione

i rappresentanti della ONG Sea-Watch per dialogarci, come se un sindaco di un Comune accogliesse nel municipio chi ha speronato l'auto dei Carabinieri del proprio territorio. Vergogna!

quanto serve solo la volontà; l'ultimo dei funzionari in telelavoro può concepire un cartello su indicazione delle politiche del Governo di maggioranza. Spero venga fatto qualcosa perché le donne, le associazioni e le commissioni pari opportunità se lo aspettano.

sempre, ma di più quella del 2021 - la carta d'identità politica della maggioranza, con la sua idea di Nazione e una visione organica, di cui invece manca. Approvata in fretta e furia alla Camera, con tempi di discussione compressi in Commissione, arriva al Senato, com'è noto, un testo blindato sul quale si impedisce la discussione parlamentare e si chiede l'approvazione in tempi *record* per evitare l'esercizio provvisorio. La spunterete con l'ennesimo voto di fiducia, ma l'Italia vi guarda e vi giudica insieme a noi. Si tratta di un disegno di legge di bilancio che vale 40 miliardi, tecnicamente e politicamente sbagliata, che non è una sintesi, ma una sommatoria frammentaria di *bonus* improduttivi improduttivi e microinterventi tra i più disparati, frutto di compromessi tra le forze di maggioranza e, un *bonus* dopo l'altro, volete gettare sabbia negli occhi per nascondere i buchi neri ed i grandi esclusi dalla manovra, i convitati di pietra, i gruppi più vulnerabili e fragili colpiti dalla pandemia, i meno garantiti, ma anche i malati oncologici e i bambini. Su questo voglio dire una cosa: in tutti questi mesi funesti, non ho mai sentito parole per i bambini privati della libertà di giocare e di socializzare, di andare a scuola nella normalità, non ho sentito parlare di supporto psicologico non solo per i bambini, ma anche per i tanti adulti, le ricadute della pandemia sulla qualità della vita sono importanti. Ma torniamo al punto, ovvero agli esclusi. Penso ai ristoratori, agli operatori turistici, a tutto l'indotto, anche alle famiglie dei dipendenti, al settore del *wedding* e al settore degli sport. degli sport. Penso alle imprese. Confcommercio ci ha detto che sono circa 390.000 le imprese chiuse nel 2020 per l'emergenza sanitaria e il contestuale crollo dei consumi. Tra i settori più colpiti vi sono quelli del tempo libero, le agenzie viaggi, l'abbigliamento e le calzature, gli ambulanti, la ristorazione, i trasporti. E, ancora una volta, non io, ma Confcommercio denuncia anche la perdita di imprese relative ai lavoratori autonomi e stima la chiusura per circa 200.000 professionisti. Eppure - e qui viene il punto - in dieci mesi avete avuto a disposizione circa 140 miliardi, evidentemente spesi in mille rivoli, perché nessuna categoria è stata né ristorata, né tutelata e la povertà è aumentata: cinque milioni

cosa avete fatto con tutti questi soldi per i quali abbiamo indebitato figli, nipoti e anche pronipoti? Evidentemente, tutte spese prive di criterio e gerarchie di priorità. E al banco di prova che rappresenta per tutti i Governi ogni manovra finanziaria, ci siete arrivati con il fiato corto, anzi con il fiato sul collo delle divisioni interne alla maggioranza - minacce, litigi, ricatti - e la legge di bilancio è lo specchio di tutto questo. C'è poi la pioggerella di buoni spesa, ne cito solo quattro tra i tanti: buoni spesa per rubinetti, per mobili,

rispetto alla crisi economica profonda. Paradossalmente, lasciate che dica che, alla fine, le uniche idee buone sono quelle venute dalle opposizioni e da Fratelli d'Italia, che ha lavorato per migliorare questa legge di bilancio. Tra Tra i tanti interventi, penso all'incremento di 50 milioni annui del Fondo sull'autismo, all'intervento per le scuole paritarie, ai nostri ordini del giorno su fondi e poteri per Roma Capitale e all'esonero minimo contributivo INPS per commercianti e artigiani: solo una parte di quello che è stato il contributo di Fratelli d'Italia alla manovra. Nella manovra c'è qualcosa di utile, sicuramente: la proroga della cassa integrazione

l'assegno unico per i figli. Premesso che alla Camera la proposta è passata con il voto unanime (quindi, anche con il nostro), io, prima di suonare le trombe, starei attenta. stanziato tre miliardi, quando tutti sanno che ne servono almeno sei per evitare che, togliendo il sistema vigente e introducendo quello dell'assegno unico, le famiglie vengano penalizzate. Lo vogliamo dire oppure vogliamo reclamare e decantare questo aspetto?

Lo vogliamo dire che prima ci deve essere la riforma fiscale? Non vi vendete quello che ancora non avete dato alle famiglie. Insomma, speriamo bene. Intanto, di certo c'è che avete stanziato solo quattro miliardi per la sanità, che continuate a buttare milioni per l'Expo di Dubai, che tanto piace a Di Maio, e che avete rifinanziato il fallimentare reddito di cittadinanza. Vi vantate, poi, della lotteria degli scontrini, quel gioco di Stato che dovrebbe combattere l'evasione fiscale e, intanto, dichiara guerra al contante e traccia le nostre spese. Ancora, avete lanciato il *cashback* come fosse un regalo di Stato, quando sono soldi nostri. D'altronde, voi siete quelli che, con il decreto Natale, avete deciso che Gesù doveva anticipare di due ore la sua nascita e avete sostituito l'evento Natale con la spettacolarizzazione dell'avvento del vaccino e del V*-*day. *(Applausi).* Questo lo voglio dire perché avete dato un clamore mediatico alla consegna dei vaccini. Fratelli d'Italia ringrazia i militari impegnati nel trasporto, ma vedere Ministri e supercommissari

forse una manovra diversa. Per questo, però, servirebbe un altro Governo, un Governo diverso, patriottico, di centrodestra, innamorato dell'Italia e degli italiani: tutto quello che voi non siete.

legge rappresenta la base della programmazione economica del prossimo anno e del prossimo triennio. Sicuramente sarà all'insegna della solidarietà, ma anche del lavoro. L'opposizione ha già espresso il suo voto contrario alla Camera e naturalmente lo confermerà al Senato. È legittimo e fa parte della dialettica democratica. Tuttavia, vorrei credere che, almeno in questa circostanza, il significato del voto non si esaurisca in un semplice no. Spero raccolga anche la storia di un lavoro comune e di una buona volontà, che sappiamo essere stata operosa in tutte le parti dell'emiciclo e che più di qualche buon frutto ha portato al Paese. Come dice Primo Mazzolari, infatti: non vogliamo portare via a nessuno il suo piccolo star bene. Vogliamo impedirgli che questo piccolo star bene determini lo star male di molti.

La legge di bilancio, in un'ottica prospettica, tiene conto della necessità di salvaguardare questo importantissimo settore, con il suo indotto che - va ricordato - rimane ingente. Già nell'articolato approvato dal Consiglio dei ministri era stata prevista una norma davvero importante, che permette alle compagnie aeree di mantenere il requisito della prevalenza dei trasporti internazionali, consentendo di beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA alle compagnie aeree che rispettavano tale requisito già nel 2019. A legislazione vigente, infatti, il requisito della prevalenza del trasporto internazionale avrebbe dovuto essere mantenuto anche nell'anno in corso, ma, con il blocco dei voli e le forti limitazioni del traffico, le compagnie aeree avrebbero fatto molta fatica a rispettare il predetto requisito, perdendo di fatto la possibilità di beneficiare della non imponibilità dell'IVA. Questo avrebbe prodotto un importante aggravio dei costi, dovendo pagare l'IVA sulle fatture ancora non emesse e su quelle già emesse. Con la norma introdotta nella manovra di bilancio, invece, i vettori che avevano tale requisito nel 2019 lo conservano anche nel 2020, evitando così un forte aggravio dei costi. Anche i gestori aeroportuali, che attendevano da tempo, hanno subito perdite considerevoli. Le perdite subite dagli aeroporti italiani nel primo semestre 2020 sono stimate pari a circa 1,1 miliardi in termini di fatturato e a circa 800 milioni in termini di ricavi al netto dei costi operativi. Già dai primi provvedimenti di ristoro delle perdite economiche il MoVimento 5 Stelle ha costantemente proposto la costituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti non solo dai gestori aeroportuali, ma anche dalle società di *handling* e manutenzione. Qui faccio un piccolo appunto: nella legge di bilancio quello che manca al momento sono le società di manutenzione, cosa che dovrà essere recuperata nel prossimo provvedimento utile. di legge di bilancio che ci apprestiamo a votare domani è prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pari a 500 milioni per la compensazione dei danni subiti da parte dei gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ente ENAC e dai prestatori di servizi aeroportuali e di assistenza a terra nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello specifico sono divisi così: 450 milioni sono destinati ai gestori aeroportuali e 50 agli *handler*. L'importo del contributo, che può arrivare fino al 100 per cento del pregiudizio subito, è calcolato sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza Covid-19, al netto delle riduzioni dei costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 dovute all'accesso agli ammortizzatori sociali, alle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza, agli eventuali importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo anno. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti, nel senso che l'ammontare dei contributi riconoscibili superi lo stanziamento, si procede a una riparametrazione del contributo in maniera proporzionale, comunque nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stanziate. Le modalità operative di fruizione del contributo dovranno essere fissate con uno o più decreti ministeriali del MIT e del MEF, da emanare entro il 31 gennaio 2021 (quindi con una certa rapidità, che mi auguro ci sia), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sette giorni. Il parere delle Commissioni rappresenta un passaggio veramente importante, durante il quale poter valutare i criteri che vengono definiti per l'accesso al contributo (quelli che io definisco paletti), per garantire la giusta trasparenza e finalizzazione delle risorse pubbliche. Il contributo ha la finalità di ripianare, almeno in quota parte, le perdite subite e non può essere utilizzato come un contributo a pioggia, a fondo perduto e senza vincolo di destinazione. Infine, un'altra importante novità introdotta nella legge di bilancio riguarda la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per il settore anche da parte delle imprese del settore che hanno accesso alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) e non solo da parte di quelle che hanno fatto ricorso o ricorrono attualmente alla Cassa integrazione straordinaria, come previsto dalla disciplina vigente, che regola il funzionamento del Fondo stesso. Come è evidente, si tratta di un intervento in favore dei lavoratori, che, ricevendo l'indennità CIGD, grazie alla misura introdotta nelle legge di bilancio, possono anche avere l'integrazione da parte del Fondo per il settore Il mio personale auspicio, alla luce dell'esperienza, è che l'incremento delle istruttorie non rallenti il complessivo andamento del Fondo e delle relative erogazioni in favore dei lavoratori, che nei mesi precedenti hanno purtroppo scontato dei ritardi.

In definitiva, si tratta sicuramente di misure volte a mitigare gli effetti negativi della crisi, in attesa di un riordino complessivo dell'intero settore del trasporto aereo, che mi auguro possa presto vedere la

ma si chiude con una speranza di rinascita e di rinnovamento, grazie all'arrivo del vaccino e alla prospettiva dell'imminente disponibilità di ingenti risorse europee per la ripresa. una prospettiva che lascia intravedere importanti opportunità di crescita, alcune delle quali iniziano a delinearsi già con la legge di bilancio al nostro esame, anche se, per forza di cose, ci troviamo a votare un bilancio che non può che essere molto diverso da quelli degli anni passati, anche solo per il fatto che dobbiamo fare i conti, quest'anno, con un calo del PIL che presumibilmente si attesterà attorno a -9 per cento: un inedito per il nostro Paese. Come Italia Viva siamo orgogliosi di avere spinto per far approvare delle misure, che non rappresentano solo un beneficio economico per i comparti direttamente interessati, ma che sono, prima di tutto, provvedimenti di equità, di giustizia sociale e di sostegno alla ripresa. Mi riferisco per esempio all'introduzione dell'assegno unico per ogni figlio: uno strumento che, a partire dal primo luglio prossimo, rappresenterà l'architrave di una nuova politica per le famiglie, attraverso la dotazione iniziale di tre miliardi di euro, grazie all'impegno del ministro Bonetti. è stata studiata allo scopo di supportare la genitorialità, conciliarla con la vita lavorativa e far fronte a quell'emergenza demografica, che rischia di venire ulteriormente aggravata dal Covid. misura a cui abbiamo voluto affiancare ulteriori sostegni per le famiglie, a partire dall'estensione del congedo di paternità, al rinnovo del *bonus* bebè, alla previsione di 50 milioni di euro per favorire il rientro delle lavoratrici dopo il parto. Particolarmente significative sono anche le misure di decontribuzione, introdotte per favorire l'occupazione femminile e giovanile, soprattutto al Sud, sulla scia di quanto avevamo previsto sotto il Governo Renzi, per ridurre il costo del lavoro e favorire nuove assunzioni. Pure è molto positiva l'istituzione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 40 milioni di euro per i prossimi due anni. due anni. Tra i risultati conseguiti da Italia Viva, siamo contenti anche di quello che abbiamo chiamato il cosiddetto reddito di libertà, cioè lo stanziamento di sei milioni di euro da destinare alle donne maggiormente vulnerabili, vittime di violenza ed in condizioni di povertà, in modo che, grazie ad un contributo mensile, possano prendere parte a percorsi di formazione, riuscendo così ad emanciparsi e ad acquistare una propria autonomia che consenta loro di uscire da situazioni di dipendenza sia emotiva che economica. Un bel segnale che arriva da questo disegno di legge di bilancio, grazie all'impegno di Italia Viva, sono anche le diverse misure a beneficio della proiezione del sistema Paese nel mondo, con evidenti ricadute a livello nazionale. Innanzitutto, va salutato con favore il fatto che il Governo abbia risposto positivamente alla nostra richiesta di dotare il Fondo cultura di risorse idonee a sostenere l'insegnamento della lingua e cultura italiane all'estero. Con la previsione di 132 milioni di euro per il prossimo triennio si ripristina sostanzialmente quanto venne a suo tempo stanziato dal Governo Renzi, con conseguenti e tangibili vantaggi per la promozione culturale del sistema Paese all'estero. poi riusciti a reintrodurre l'esenzione IMU per il 50 per cento dell'importo per un unico immobile di proprietà posseduto in Italia da quei connazionali residenti all'estero che percepiscono una pensione in convenzione internazionale. Si tratta di un bel risultato ad un anno dalla sua soppressione in sede di legge di bilancio. È un risultato che risponde alle tante richieste che ci sono pervenute nei mesi scorsi dalle nostre comunità in giro per il mondo, ma anche da numerosi Comuni, al Sud come al Nord. Tutte amministrazioni che hanno deliberato in giunta per chiedere l'abolizione dell'imposta e che si sono fatte carico, spesso a proprie spese, dell'esenzione, perché consapevoli di quanto questa misura possa rappresentare un'ancora per arginare lo spopolamento ed il degrado di tanti splendidi borghi, località che in questo modo non cadranno preda dell'abbandono architettonico e, allo stesso modo, potranno fruire di quel ritorno economico prodotto dai concittadini all'estero a beneficio delle proprie terre d'origine. Siamo contenti di avere potenziato ulteriori interventi volti a contrastare la cosiddetta fuga dei cervelli. È stata infatti ampliata la platea dei beneficiari del fondo cosiddetto controesodo, una misura di sostegno al rientro rivolta a lavoratori altamente qualificati, docenti, ricercatori e scienziati che, anche se rientrati in Italia prima del 2020 grazie al nostro lavoro, potranno usufruire degli incentivi che mirano ad evitare nuove partenze. È poi una soddisfazione il fatto che, grazie al nostro intervento, siano state stanziate le risorse necessarie per il rinnovo dei Comites (Comitati degli italiani all'estero), un importante strumento di democrazia di base, le cui elezioni meritano la nostra giusta attenzione. Insomma, signor Presidente, come Italia Viva ci siamo impegnati per misure coraggiose, eque, capaci di dare un importante contributo anche in termini di sviluppo e di crescita. crescita. Crediamo che sia necessario poiché ci troviamo di fronte ad un passaggio epocale, in cui sta a noi la scelta se entrare nei libri di storia come il Parlamento che, al pari del Dopoguerra, è riuscito a fare buona politica e ad investire per ricostruire un Paese un Paese che sia degno di una delle maggiori potenze mondiali, oppure se vogliamo essere ricordati come coloro che hanno buttato alle ortiche l'occasione storica di rigenerare il Paese. Ecco, signor Presidente, noi di Italia Viva scegliamo di essere parte della prima categoria e ci auguriamo che tutte le forze di maggioranza vogliano fare, insieme a noi, lo stesso. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, oggi interveniamo in quest'Aula a pochi giorni dal 31 dicembre

meritata. Voi, di fatto, avete esautorato questo ramo del Parlamento. Di fatto, il Senato della Repubblica in questa occasione è stato messo all'angolo, cioè non esiste più. Capisco che siate siate molto indaffarati nelle lotte intestine all'interno della maggioranza di cui leggiamo costantemente sui giornali. Le vediamo poco in Aula, magari quando interviene qualche *leader* politico,

Di fatto non serviamo a granché oggi, tranne che a ribadire, come stiamo facendo adesso noi del Gruppo Fratelli d'Italia, la nostra posizione e le nostre argomentazioni per far sapere al popolo italiano quello che avremmo pensato sulla manovra di bilancio non abbiamo potuto fare nelle sedi opportune, in Commissione e in Aula, attraverso i nostri emendamenti. Cari amici del Governo e amici del centrosinistra e della maggioranza che governa questo Paese, allora avete un gran bel dire quando parlate - lo avete detto molto spesso

per i cittadini italiani. Per questo dobbiamo ringraziare voi che fino all'ultimo avete continuato a discutere, a patteggiare e a dividervi su come accontentare questo o quell'altro all'interno della maggioranza. Niente, però, a favore dei cittadini, a favore del popolo italiano che con questa manovra

dell'anniversario della nascita del Partito comunista italiano; su queste cose siete sempre pronti e sicuri di trovare i contributi.

Signor Presidente, prima abbiamo fatto una richiesta precisa. Vorremmo capire se la risposta del Governo avverrà prima della fine della discussione generale per per evitare che si creino problemi, visto che già i tempi sono molto compressi sulla discussione. Spiegherà il Governo qual è il problema dell'eventuale errore contenuto nella manovra; vorremmo, però, che ci fosse almeno un minimo di discussione su questo tema perché troviamo corretto e doveroso

non in sede di replica - visto che ciò impedisce alle minoranze di poter eventualmente discutere del tema - ma in via incidentale prima. Se è così, ripeto, non c'è alcun problema; l'importante è che si discuta dell'aspetto. Se, però, la forzatura è: replichiamo e facciamo finta di niente, va bene, trarremo le nostre dovute conseguenze.

anche dopo l'intervento che il senatore Pichetto Fratin ha svolto a nome del nostro Gruppo, ha ora ribadito il presidente Romeo, sia la questione di fondo: avete ammutolito il Senato, che farà soltanto una registrazione notarile di ciò che è avvenuto alla Camera. Non c'è alcuna discussione di merito, la fiducia immediata è stata annunciata, non ci sono coperture; ci dovrebbe essere, quindi, il meccanismo dello scostamento di bilancio con la maggioranza assoluta, che difficilmente avreste, e quindi c'è una prevaricazione totale. Nei pochi minuti che mi spettano in questo dibattito voglio richiamare una questione specifica, quella di Roma, una delle grandi assenti di questo disegno di legge Il nostro Gruppo - io per primo - aveva presentato alcuni emendamenti riguardanti delle infrastrutture fondamentali per la Capitale, molto provata da anni difficili, anche con altre amministrazioni, ma adesso devastata dall'ultima amministrazione Raggi, priva di prospettive, di strategie, e anche di ascolto nel Governo, all'interno del quale il suo partito svolge un ruolo importante, sebbene i 5 Stelle nulla abbiano fatto per Roma nelle leggi di bilancio che hanno gestito in questi anni stando comunque al Governo. avevo presentato due emendamenti che la fiducia "trancherà", cancellerà: uno riguardante il piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana di Roma, che prevedeva stanziamenti significativi; un altro per il famoso completamento della linea C della metropolitana di Roma. Questi emendamenti non saranno discussi, come non sono stati discussi alla Camera, dove *in extremis* è stato approvato un ordine del giorno che noi abbiamo sostenuto con le firme dei nostri colleghi

possono comunque esercitarsi vanamente con tali atti di indirizzo. Noi abbiamo firmato l'ordine giorno che comunque impegnerebbe il Governo a stanziamenti per Roma. le celebrazioni dei centocinquanta anni di Roma Capitale d'Italia sono state organizzate dal Governo o dall'amministrazione comunale in modo decoroso. La Capitale appartiene a tutti, alla storia della Nazione: non è un problema di campanilismo. C'è l'assoluta ignoranza di queste esigenze. Nel 2009 abbiamo varato una legge, che chiediamo si porti ancora più avanti, per dare alla Capitale d'Italia i poteri che altre capitali nel mondo occidentale e non solo hanno, ma servono anche stanziamenti. Avete detto di il sindaco di Roma Raggi sta dicendo che aprirà un tavolo dopo l'approvazione dell'ordine del giorno alla Camera. Tuttavia, l'ordine del giorno, che noi abbiamo sostenuto, sottoscritto e votato, serve a ben poco: dovevate approvare delle norme per la Capitale d'Italia nella legge di bilancio. È inutile che il sindaco Raggi, che non ha mai ascoltato nemmeno i parlamentari nella sua totale incapacità e negazione della democrazia del territorio, oggi dica di aprire un tavolo per la Capitale d'Italia. Faccia le metropolitane. La Raggi ha annunciato una seconda funivia, quando della prima non si è visto neanche un bullone nella

La Raggi ha abbandonato Roma. Voi grillini non avete fatto nulla per Roma. Il disegno di legge di bilancio in discussione non concede nulla alla Capitale e ha preso per i fondelli tutti gli italiani. Il Governo agisce privo di coperture e, invece di rispondere al Senato, risponde agli amici. Siete minoranza nel Paese. Avete fatto affondare questo Paese. Non andrete avanti a lungo Signor Presidente, onorevoli colleghi, concentrerò il mio intervento sulle misure legate alla sanità che in questa manovra di bilancio 2021 hanno rafforzato le risposte alla drammatica emergenza che stiamo affrontando, ma al tempo stesso ci hanno portato a ripensare l'intero sistema, per investire maggiori risorse agendo su aspetti di grande fragilità. La tutela della salute è un diritto costituzionalmente garantito, il più importante, e il nuovo coronavirus ha riportato al centro del dibattito politico la qualità del sistema sanitario del nostro Paese e i princìpi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità. Si tratta, dunque, non di affrontare solo la crisi in corso, di avviare un percorso che ci consenta di irrobustire e consolidare la sanità del futuro, che di fatto rappresenta un settore della vita pubblica che sarà sempre più decisivo. Certo, avremmo potuto - come abbiamo tante volte detto - fare di più e dovremo farlo, ma credo che la manovra contenga passi importanti per andare verso quell'impegno che tutti ci siamo assunti di utilizzare molte delle risorse che arriveranno dall'Unione europea per rafforzare la sanità pubblica. L'Italia ha destinato quest'anno alla sanità risorse economiche pari al 6,5 per cento, se si considera la spesa finanziata solo con fondi pubblici e, quindi, in linea con la media OCSE del 6,6 per cento, anche se emergono ancora segnali di difficoltà. Dobbiamo ancora migliorare e investire tenendo in considerazione i tre fattori segnalati dalla Commissione europea e l'efficacia, l'accessibilità e la resilienza. Ritengo - per esempio - che, proprio nell'ottica del miglioramento del sistema, vada anche affrontato in modo non ideologico il tema della riforma del Titolo V cercando di risolvere alcune delle criticità emerse palesemente in questa fase di emergenza. Nel breve tempo a disposizione mi posso solo limitare a porre l'accento su alcune tra le principali misure della manovra, come l'incremento di un ulteriore miliardo del fondo sanitario; misure specifiche per il personale; risorse per l'assunzione; un ulteriore aumento del numero di contratti di formazione dei medici specializzandi; i 400 milioni destinati all'acquisto dei vaccini e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti Covid-19; gli ulteriori 70 milioni di tamponi antigenici rapidi e naturalmente i due miliardi in più per l'edilizia sanitaria. poi aggiungere alcune questioni della manovra che ritengo importanti e mi stanno particolarmente a cuore. Sono questioni disseminate nei vari commi, ma riconducibili a tre aree di indirizzo molto importanti. In primo luogo, vi è la valorizzazione degli interventi sulle categorie più fragili, e sto parlando del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, dell'incremento del fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, dell'istituzione di un fondo per l'Alzheimer e le demenze per garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva. Importantissimi sono poi gli investimenti per patologie che colpiscono le donne, che vanno dai test genomici per il carcinoma mammario in stadio precoce al sostegno della ricerca sull'endometriosi. In secondo luogo, ritengo importante che venga valorizzata l'integrazione interprofessionale tra le professioni sanitarie. Va bene, quindi, la valorizzazione di tutti i dipendenti appartenenti alle professioni sanitarie. infine, l'innovazione, consapevoli che la medicina del futuro avrà un ruolo decisivo. Penso - per esempio - alla telemedicina, che consente di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto. L'apporto, dunque, di diverse competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute deve essere riconosciuto, rafforzato e ampliato. Presidente, la legge di bilancio rappresenta un segnale positivo che va nella direzione auspicata di destinare, come priorità assoluta, maggiori risorse alla sanità per avviare, grazie ai fondi dell'Unione europea, il più grande piano di investimento di cui il nostro Paese ha tanto bisogno. *(Applausi)*.

sediamo noi come rappresentanti del popolo italiano è chiamato non a discutere della legge più importante di quest'anno, ma solo a ratificare le decisioni già prese altrove dal Governo e dalla maggioranza. Noi votiamo una legge di bilancio scritta con trentacinque giorni di ritardo, approvata in corsa tra Natale e Capodanno, approfittando del fatto che gli italiani - per fortuna - hanno ben altro a cui pensare che al mercimonio delle poltrone e delle marchette elettorali fatto all'interno della compagine di Governo.

vengo da una terra che purtroppo dall'attuale Governo è considerata di frontiera, la parte Sud del Piemonte, della provincia di Cuneo, enormemente penalizzata a livello infrastrutturale, dove i cantieri, come quello della Asti-Cuneo, sono bloccati ormai da oltre otto anni, dal 2012. Nonostante i milioni di chiacchiere del ministro De Micheli, ad oggi è tutto fermo.

Per quell'alluvione abbiamo avuto dal Governo 15 milioni di euro per tutto il territorio. C'è però un problema enorme, perché il collegamento transfrontaliero con la Francia, il tunnel di Tenda (strada statale 20), è interrotto: mancano le risorse per il completamento e manca la nomina di un commissario che sveltisca la pratica burocratica. Bisogna avviare i cantieri per completare l'opera e per ricongiungerci con la Francia e con la Liguria dal Sud del Piemonte: è fondamentale.

(dati del 2018) rispetto a quello che riceve in termini di servizi e di investimenti: non dimentichiamolo mai. Voi dovevate gettare le basi per la ripresa della nostra economia, ma avete continuato con la politica dei *bonus*, il sostegno agli amici degli amici, che poi spesso sono i nemici del nostro Paese, sono i nemici dell'Italia. Una misura che avrebbe aiutato le nostre imprese e le famiglie - lo abbiamo detto più volte - sarebbe stata la riduzione dell'IVA sui consumi

nulla di tutto questo. Avete ammesso che il reddito di cittadinanza non funzionava e non va bene: non ha consentito di assumere nessuno, se non forse i *navigator*, che devono ancora essere formati. Oggi è stato rifinanziato per 4 miliardi di euro. Il rapporto tra assistenzialismo e sostegno a chi vuole lavorare è di 8 a 1: 500 milioni di euro per le politiche attive sul lavoro. È una vergogna per tutti gli italiani. qui c'è non la formica, ma la cicala, che spende tutto quello che ha e spreca le risorse di cui dispone, e voi lo fate semplicemente per rimanere attaccati alla poltrona. Dovete andare a casa, e non solo per Capodanno: ve lo chiediamo con tutto il rispetto che abbiamo per i milioni di italiani che con voi non vogliono più avere nulla a che fare. Prima gli italiani, sempre. *(Applausi)*.

Sulla famiglia abbiamo fatto solamente dei proclami; sulla scuola *idem*. Noi parliamo dello stanziamento di un fondo sull'assegno unico; sicuramente una manovra

una quota sicuramente irrisoria rispetto alla necessità. Parliamo inoltre di un intervento che tiene conto della valutazione ISEE

Abbiamo un progetto per il futuro? Si utilizzano molto termini come visione, progettualità e resilienza. Qual è però la nostra visione? Martin Luther King direbbe «*I have a dream*». Qual è il nostro sogno? Noi siamo andati avanti quest'anno con i famosi *bonus*; anzi, devo dire che è da qualche anno che si va avanti in questo modo. Ci vuole una progettualità condivisa, dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Quando noi parliamo di attenzione alla famiglia, teniamo conto di questo soggetto, di questa prima agenzia educativa e, quindi, della crisi economica a Parliamo spesso di crisi economica e in questi giorni si parla di *recovery plan* e di *recovery fund*.

Con i debiti. Questi ultimi però, per poter essere sostenuti, hanno bisogno di un progetto di risanamento. E qual è il nostro progetto di risanamento? Qual è il bandolo della matassa se non quello demografico?

acquistando automobili e case, mettendo su famiglia, procreando. Abbiamo detto mille volte che ogni bambino nel PIL nazionale annuo incide positivamente di 35.000 euro annui. Noi in undici anni abbiamo perso oltre cinque miliardi. Sono tanti gli interventi che anche personalmente ho proposto alla legge di bilancio e che sono rimasti assolutamente inascoltati. Quindi, tornando al mio intervento introduttivo, è chiaro che viene detto di

anche scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio e al Ministro della salute e cercando di interpellare il Vice Ministro. L'errore grave che voglio portare alla coscienza di tutti voi è la cancellazione dalla legge di bilancio

un test che viene fatto in tutta Italia - perché inserito nei livelli essenziali di assistenza - a tutti i bambini alla nascita, il quale permette di diagnosticare in modo precocissimo l'eventuale affezione da malattia rara. È un fatto di democrazia e giustizia e riflette un principio di ordine costituzionale (il diritto alle cure, se non il diritto alla salute).

quella visibilità che - mi si permetta di sottolineare - il Presidente del Consiglio ha voluto tenere per sé come delega, ma di cui non mi sembra si sia tenuto affatto conto in questa occasione. Per di più, dall'altra parte abbiamo munificamente lasciato che le grandi imprese produttrici di tabacco pagassero il risibile aumento di pressione fiscale del 5 fiscale del 5 per cento. Abbiamo tolto ai poveri per dare ai ricchi; abbiamo tolto ai bambini perché li abbiamo lasciati del tutto sprovvisti dell'unica possibilità che hanno di avere una vita normale, per lasciare che si arricchiscano alcuni altri perché rappresentano *lobby* di potere.

e perché nei prossimi giorni lavoreremo soprattutto per la ripresa e la rinascita del nostro Paese. Sappiamo quanto difficili durante i quali tutti i settori - e le famiglie *in primis* - sono stati duramente colpiti dalla pandemia, ma dobbiamo guardare avanti. Accanto ai provvedimenti come i vari decreti ristori e a quello che arriverà dopo e alla legge di bilancio oggi, si iniziano comunque a delineare degli aiuti concreti, a cui ogni Gruppo parlamentare, a cominciare da quelli di maggioranza e dal mio Gruppo Italia Viva, ha sicuramente cercato di contribuire nella maniera

però non portano certamente a cambiare il volto duramente provato di questo Paese, dell'Europa e non solo. Abbiamo certamente bisogno, invece, di ridisegnare una visione, una strategia per il 2021, soprattutto pensando alle fondamentali risorse che arriveranno

parere essenziali, di avanzare delle proposte che vanno proprio nella direzione di avere una visione strategica, perché parliamo di investimenti davvero ingenti per

Per quanto riguarda la scuola, faccio due brevi accenni. Sicuramente c'è un importante intervento sull'incremento del personale e, nello specifico, di docenti di sostegno e di docenti da impiegare nella scuola dell'infanzia, di assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo e di collaboratori scolastici. altre disposizioni che vanno ad incrementare le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innovazione digitale, alla didattica laboratoriale e al cosiddetto fondo 0-6,

per occupazione, per il sistema di volontariato, in modo particolare con il fondo di 50 milioni per potenziare l'attività sportiva di base. Infine, finalmente finalmente c'è anche il riconoscimento di un esonero anche parziale della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo. ancora poco, ma è un segnale che va nella giusta direzione. Sta a noi adesso, nei prossimi provvedimenti, pensare davvero ad avere una strategia in grado di aiutare e cambiare il volto di un Paese che è stato duramente

culturale di un Paese che ha un patrimonio straordinariamente ricco che non ha uguali nel mondo. Il Gruppo Italia Viva voterà ovviamente a favore della legge di bilancio.

Presidente, la legge di bilancio in esame arriva con oltre un mese di ritardo. Siamo solo a due giorni dal baratro del bilancio provvisorio e tutto questo per colpa di una maggioranza litigiosa, che pensa ai rimpasti e alle poltrone. È chiaro che è una semplice e bieca spartizione del potere. Avremmo voluto confrontarci su questo provvedimento. Avremmo voluto portare il nostro contributo, che mai è mancato per il bene della Nazione e anche degli italiani. Ma c'è stato impedito, in particolare qui in Senato, dove saremo costretti a fare un esame rapidissimo, in meno di

concertazione su questa sessione di bilancio. Invece domani apporrete l'ennesimo voto di fiducia a una legge di bilancio che manca di una visione e di una identità nazionale capaci di parlare agli agli italiani e soprattutto di dare loro una prospettiva. Non sono bastati i 140 miliardi degli scostamenti di bilancio di bilancio, che sono stati in qualche modo anche sperperati in mille rivoli. Ora, anche i 40 miliardi andranno ad aggiungersi

imprenditori, di ristoratori e famiglie che non sanno qual è il futuro che li attende. Avreste dovuto parlare alle imprese. Avreste dovuto parlare ai lavoratori, a chi è caduto in disgrazia e in povertà, offrendo soluzioni e possibilità di rialzarsi, e non certo l'elemosina dei ristori. Avreste dovuto dare risposta alle tante imprese, piccole e grandi, sulle quali si è abbattuta la crisi

Avreste dovuto affrontare la grande questione dei costi fissi, che continua purtroppo a rimanere il grande tema inevaso. Ne parliamo quotidianamente e, invece, anche qui zero opportunità. Mi chiedo e vi chiedo: che senso ha dare un ristoro, se poi costringete a pagare gli arretrati delle tasse per mesi e mesi? Questa è una domanda alla quale non riusciamo ad avere è una domanda alla quale non riusciamo ad avere risposta. Con quali entrate, che non ci sono, pensate che potranno essere coperti quei costi? Sono queste le domande alle quali neanche in questa manovra avete dato una risposta. Parlate di riaprire le scuole, ma non avete fatto nulla per migliorare il trasporto pubblico locale. Sicuramente il trasporto pubblico locale è un elemento essenziale, strategico per far ripartire il settore scolastico. Ci abbiamo pensato noi con un nostro emendamento nel decreto-legge ristori, grazie al quale abbiamo stanziato Questo consentirà di aiutare il trasporto pubblico attraverso delle convenzioni con gli NCC, con i taxi e le aziende di bus che sono ferme. Tutto questo sicuramente aiuterà. Che dire del settore turistico e ricettivo, che è uno dei tanti che lamenta l'inadeguatezza del vostro operato? Per il settore turistico, tra le risorse più importanti del nostro Paese, non è stato fatto nulla. Soprattutto, non è stato fatto nulla per le agenzie di di viaggio. Non è stato alcun tipo di sostegno. La stessa domanda potremmo farle anche per il settore degli eventi. È un mondo che da quasi un anno è fermo, con migliaia di professionisti

che non possiamo essere soddisfatti, così come non lo sono gli italiani. Ma non vi illudete: prima o poi - speriamo prima - il popolo vi giudicherà e ribadirà con forza lo stesso no che noi oggi annunciamo in quest'Aula.

una legge di bilancio importante (40 miliardi), che approviamo a conclusione di un anno sicuramente complesso e tormentato. un primo tassello di una strategia che riguarda l'anno prossimo e gli anni a venire, a cui contribuiranno il prossimo decreto ristori, che è all'orizzonte, ma soprattutto il Piano nazionale di recupero e resilienza, che affronteremo nei primi mesi dell'anno nuovo. Tramite tale Piano dovremo definire in modo strategico gli orizzonti e gli obiettivi verso cui orientare il cammino di questo Paese. Tale consapevolezza è generale e lo è sicuramente in modo molto forte per quanto riguarda il comparto agricolo; un comparto che, in questo anno sicuramente molto complesso, ha comunque lavorato, fornendo ai cittadini italiani - e non solo - prodotti di altissima qualità, di grande sostenibilità ambientale e di grandi contenuti salutistici. Nel corso dell'anno si è cercato di accompagnare questo settore

che ci ha permesso di portare l'anticipo PAC dal 50 al 70 per cento; credo che questa sia stata una svolta straordinaria per il mondo agricolo in termini di immissione di liquidità alle imprese. C'è poi tutto il tema dei *bonus*, del fondo perduto,

una serie di misure generali, dall'esenzione IRPEF per i redditi dominicali e i redditi agrari al 50 per cento per le imprese all'esonero dal versamento dei contributi INPS per due anni per le nuove imprese che stanno partendo. una serie di interventi molto puntuali, dall'IVA al 10 per cento sui prodotti da asporto, che interessa moltissime aziende agricole, ai fondi di sostegno per le filiere dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,

per la prima volta nella storia della Repubblica una manovra economica arriva qui in Senato, in seconda lettura, a soli tre giorni dalla fine dell'anno e solo grazie alla responsabilità delle forze d'opposizione si scongiurerà l'esercizio provvisorio. Ormai, purtroppo, non ci stupiamo più dell'operato del Governo, troppo impegnato a risolvere i molti dissidi al suo interno. Il Governo ha presentato la manovra di bilancio con più di un mese di ritardo, lasciando poco spazio per l'esame alla Camera dei deputati e praticamente nessuno al Senato. Questo è veramente inaccettabile per la democrazia del nostro Paese. poche ore per discutere il principale atto di politica economica, nel momento più difficile per la nostra Nazione dal dopoguerra. Questa legge di bilancio doveva gettare le basi per la ripresa da una crisi economica e sanitaria senza precedenti. Doveva essere l'occasione per condurre il nostro Paese verso un futuro di speranza e obiettivi di crescita. Un provvedimento da 40 miliardi di euro senza un quadro di insieme ben delineato: così l'ha definito l'Ufficio parlamentare di bilancio e noi della Lega non possiamo che condividere. Tuttavia, durante il passaggio alla Camera dei deputati, abbiamo cercato di migliorarlo, con senso di responsabilità nei confronti del Paese e delle tante categorie, che in questo momento stanno soffrendo. Lo abbiamo sempre fatto e dimostrato in questi mesi, dando il nostro voto agli scostamenti di bilancio, per un ammontare complessivo di indebitamento netto che supera i 100 miliardi di euro. tante risorse, ma prive di una visione di insieme, come state dimostrando in questo momento: tante idee e ben confuse. dunque la progettualità necessaria per una ripartenza solida, con la possibilità di utilizzare le risorse anche derivanti dal *recovery fund* per rimediare alle politiche lesive degli anni passati e cogliere l'opportunità di ridisegnare il futuro, tenendo conto dei cambiamenti nella società, composizione dei nuclei familiari, delle esigenze economiche, della rigenerazione urbana e dell'erogazione dei servizi. Cambiare, rinnovare e ricostruire: dovevano essere queste le linee guida, ma forse è troppo per questo Governo. Visione e prospettiva sono parole completamente sconosciute. Fuori da questi palazzi esiste il mondo reale, che aspetta risposte concrete, soprattutto dopo i vari *lockdown*. Avete fermato l'Italia in vari modi, colorando il nostro calendario e la nazione, creando confusione, ponendo i cittadini, quando quando si svegliano la mattina, nella condizione di dover consultare i siti Internet o i giornali per sapere cosa possono o non possono fare e lasciandoli nell'incertezza. Incertezza: questa è la parola con cui i cittadini devono convivere in attesa dei vari DPCM, che arrivano la sera con le conferenze stampa ed entrano in vigore la mattina. modo, chi deve organizzare e programmare il lavoro non sa come fare gli acquisti, stabilire i turni di lavoro o mettere in cassa integrazione i dipendenti. Ne è un esempio la gestione della questione del turismo invernale: tutte le Regioni alpine hanno presentato un protocollo per ripartire in sicurezza, ma solo in questi giorni, quindi dopo un mese, il È evidente che la questione sanitaria è prioritaria, ma è altresì evidente che sono necessarie risposte certe, con indicazione di data e modalità. Soprattutto, voglio sottolineare come l'importanza della stagione invernale sia stata liquidata da molti con la frase: «È solo una sciata». Invece c'è un intero comparto che vive di questo. È noto che le aziende legate al prodotto montagna generano l'85 per cento del fatturato annuo nel periodo concentrato tra dicembre e marzo. L'attuale chiusura sta comportando la perdita del reddito per mantenere attive le imprese fino alla stagione invernale 2021. Tale perdita non sarà in alcun modo recuperabile se non a fronte di adeguate misure di ristoro e compensazione. Quindi, le ricadute su imprese, lavoratori e famiglie saranno gravissime. Sulle nostre montagne, Alpi e Appennini, c'è un comparto economico con 400.000 occupati, che vale un fatturato tra i 10 e i 12 miliardi. Chi ha amministrato un ente pubblico sa che meno introiti per le casse pubbliche derivanti da queste scelte significa meno servizi erogati ai cittadini. Quindi anche chi si occupa d'altro avrà ricadute, soprattutto le famiglie più in difficoltà.

si perde sul PIL nazionale il 5,8 per cento di un settore che ne pesa il 13 per cento. Il mondo della ristorazione registra una perdita nel 2020 di quasi 41 miliardi: una situazione che ha fatto chiudere il 14,4 per cento di bar e ristoranti, con relative conseguenze sulla filiera. Le misure messe in campo dal Governo prevedono nella legge di bilancio solo 505 milioni: sono assolutamente insufficienti. È una manovra fatta di microbonus senza una visione di insieme. *bonus* idrico, con una dotazione di 20 milioni, con 1.000 euro a beneficiario per cambiare rubinetti e sanitari. La dispersione dell'acqua è per l'Italia uno dei parametri che ci rende peggiori a livello europeo: la dispersione sulla rete idrica è al 47,9

Poi ci sono i *bonus* televisori e i *bonus* cellulari, e si rifinanziano le misure assistenzialistiche: in emergenza possono essere uno strumento, ma spiace constatare che per questa maggioranza esse rappresentano misure strutturali. Peccato non mettere in campo misure che incentivino investimenti e lavoro: mi riferisco a decontribuzione e semplificazione, soprattutto in un Paese dove l'articolo 1 della Costituzione dichiara: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Inoltre, in questi giorni invito il Governo a fare attenzione al nuovo regolamento europeo di *default*, a porre in atto una pianificazione di emergenza per gli arretrati fiscali delle aziende e di posticipare di almeno due anni l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Altrimenti, dal 1° gennaio, per classificare un'impresa in *default* basterà un arretrato di pochi euro, superiore all'1 per cento dell'esposizione totale verso la banca: in piena pandemia e con le chiusure imposte, questo sarebbe un'ulteriore beffa e un ulteriore danno per le imprese. conclusione, va bene il *bonus* sugli occhiali, ma per il Governo consiglierei l'acquisto di un binocolo. se non si ha una visione a lungo termine, il futuro per i nostri figli rischia di essere davvero incerto e difficile. La responsabilità sarà vostra che avete avuto l'opportunità di investire più di cento miliardi in un solo anno e avete sprecato questa grande occasione.

ci occupiamo del disegno di legge di bilancio per il 2021 alla fine di un anno davvero difficile per l'Italia e per il mondo intero. Lo scoppio della pandemia ha causato una crisi economica con pochi precedenti nella storia e per scongiurarne gli effetti sulla carne viva degli italiani, dei lavoratori, degli artigiani, delle piccole e medie imprese, noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo messi subito al lavoro. E così nei mesi scorsi abbiamo approvato, insieme alle altre forze politiche, provvedimenti, misure, aiuti, finanziamenti, ristori ed erogazioni che ammontano a 100 miliardi di euro per dare risposte immediate a tutti coloro che si trovavano e si trovano ancora in situazioni di difficoltà. È stato uno sforzo enorme di cui siamo orgogliosi. Abbiamo cercato di interpretare al meglio le istanze dei cittadini, che chiedono a noi tutti un impegno assoluto per risolvere i loro problemi. Di certo i cittadini non vogliono sentir parlare di crisi o di verifiche. Oggi, come dicevo, ci occupiamo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 e nei primi mesi dell'anno prossimo continueremo a lavorare nel solco di quanto fatto finora e definiremo tutti gli aspetti del *recovery plan*, Next generation EU, il che ci consentirà di investire nel nostro Paese i 209 miliardi di euro assegnati all'Italia, un ammontare particolarmente ingente, com'è facile vedere, di cui 81 miliardi a fondo perduto, non dimentichiamolo mai, ottenuti grazie all'azione del presidente del Consiglio Conte, del MoVimento 5 Stelle e di questa maggioranza. Fondi che consentiranno di rilanciare il nostro Paese, di superare carenze e mali atavici e di riprendere a produrre in modo sostenibile, di creare ricchezza e benessere e di ridurre le ingiustizie sociali. di legge di bilancio che oggi ci occupa prevede interventi per circa 40 miliardi che, come detto, si aggiungono ai 100 approvati negli scorsi mesi. La nostra azione si è indirizzata sostanzialmente lungo quattro direttrici che riteniamo fondamentali, cioè interventi immediati per affrontare l'emergenza, misure e investimenti mirati per costruire l'Italia del futuro, all'avanguardia nei settori strategici dell'ambiente, della sanità, della scuola e dei servizi pubblici, e poi un pacchetto fiscale che si rivolge ai lavoratori e alle famiglie italiane e norme che garantiscono la protezione sociale delle fasce più deboli della popolazione. Queste direttrici si sono tramutate in alcune misure che passo ad elencare velocemente: la proroga al 31 marzo 2021 del blocco dei licenziamenti e ulteriori dodici settimane di cassa integrazione Covid; conferma fino a giugno 2021 della moratoria sui mutui, prestiti, *leasing* e della liquidità garantita dal fondo centrale per le piccole e medie imprese e da SACE: 4 miliardi aggiuntivi per la sanità; 24 miliardi in poco più di due anni per rilanciare gli investimenti delle imprese private, con particolare riguardo per i macchinari, i beni immateriali e per la formazione innovativa dei lavoratori. vi è lo sgravio al 100 per cento per chi assume donne disoccupate e per chi assume *under* 35, la conferma di un lungo periodo dello sgravio del 30 per cento dei contributi previdenziali per le imprese del Sud che assumono, e ancora, conferma e stabilizzazione della diminuzione delle tasse fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti che hanno redditi annui compresi tra 8.000 e 40.000 euro. Questa è una misura che interessa 16 milioni di italiani.

Un miliardo per dare il via al cosiddetto anno bianco sui contributi previdenziali di autonomi e professionisti. Queste due ultime misure, che ho appena elencato, sono importantissime perché abbiamo introdotto un nuovo ammortizzatore sociale, riconoscendo agli autonomi diritti e tutele che fino ad oggi avevano solo i lavoratori dipendenti. Mai prima d'ora in Italia a quattro milioni di partite IVA era stato garantito un aiuto concreto in caso di calo del reddito mai - si era intervenuti per sostenerle garantendo l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali. Continuando nell'elenco, l'assunzione di 3.000 medici e 12.000 infermieri assistenti sanitari in vista del grande piano vaccinale anti-Covid; 4 miliardi di euro dal 2021 al 2029 per il fondo per il reddito di cittadinanza, che in questi mesi drammatici ha evitato il collasso sociale per 3,5 milioni di cittadini italiani, tra cui 700.000 minori, e che, come noto, è una misura di giustizia e di inclusione sociale checché ne dicano i detrattori - che il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto e che i fatti, non le chiacchiere, hanno dimostrato essere stata decisiva per superare questa crisi economica per oltre 3,5 milioni di nostri connazionali. Proroga fino al 2022 del superbonus al 110 per cento: provvedimento che il MoVimento 5 Stelle ritiene strategico per la nostra economia, per il rilancio di un settore importantissimo per il nostro Paese, che era in sofferenza da anni, senza che i nostri attuali detrattori, allora al Governo, muovessero un solo dito per aiutare questo settore vitale per il Paese. Si tratta di una misura importantissima per la sicurezza delle nostre abitazioni e per rispettare i parametri di minore impatto ambientale, minore inquinamento e salvaguardia dell'ambiente e del Pianeta. In questo disegno di legge di bilancio ci sarebbe molto piaciuto aggiungere altri tre provvedimenti - davvero concludo - che abbiamo proposto e che riproporremo con forza

e alla regolamentazione dell'utilizzo della canapa industriale, un settore che già oggi dà lavoro a migliaia di cittadini e imprese. Ripeto, canapa industriale, cioè l'utilizzo della pianta per produrre tessuti, carta, materiali per l'edilizia, plastica biodegradabile per l'industria dei cosmetici e per quella alimentare. *(Applausi)*. La canapa industriale non ha nulla a che vedere con la droga o con gli stupefacenti, e chi afferma il contrario è ignorante o vuole sfruttare l'ignoranza di alcuni a fini ideologici e di propaganda. Infine, la rottamazione *quater* delle cartelle esattoriali, almeno fino al 31 dicembre 2019, che personalmente ho proposto sotto forma di emendamento al cura Italia e ai provvedimenti... È un provvedimento che darà respiro ai cittadini incorsi nelle cosiddette morosità incolpevoli e che sicuramente non sono evasori. In conclusione, il 2020 sarà ricordato per la scoppio della pandemia, ma anche per l'inizio della vaccinazione; sarà ricordato per una difficile crisi economica, ma anche per le misure imponenti e senza precedenti in quanto a risorse stanziate in pochissimo tempo per superare la crisi. Confidiamo che riusciremo presto a lasciarci alle spalle quest'anno difficile, questo momento drammatico, nella convinzione che, anche grazie all'azione del MoVimento 5 Stelle, l'Italia, la nuova Italia, sarà un Paese più dinamico, più sostenibile, più giusto e più equo. *(Applausi).* la nuova Italia che prima veniva citata è un'Italia senza Parlamento, dove il Parlamento non esiste più, è stato cancellato con un decreto, con un atto di fiducia. Alle ore 13,30 di oggi

per la inettitudine e la sfrontatezza di questo Governo sostenuto, reclamato e guidato dai 5 Stelle. Cancellata la democrazia rappresentativa, cancellato il ruolo del Parlamento

cioè quanto mai nessuno ha potuto fare in questo Paese nei decenni precedenti; sono cifre che corrispondono a circa sei leggi di bilancio in un solo anno. Inoltre, concludete quest'anno con una legge di bilancio che avete trasformato

milleproroghe), 10 deroghe e 20 microbonus*.* In questi numeri c'è l'inettitudine di un Governo che realizza provvedimenti a pioggia, disperde le risorse, piega il Paese sotto montagne di debiti senza consentire la ripresa economica: 50 proroghe, 10 deroghe, 20 *bonus,* a questo avete ridotto la legge principale dello Stato, che dovrebbe dare indirizzo, prospettiva e strategia a tutta l'attività economica del Paese. Ebbene, in tutto ciò vi è però un *bonus* che nascondete e che si erge su tutto. Mi rivolgo soprattutto ai cittadini che hanno votato per i 5 stelle: si tratta di un *bonus* che si erge su tutto per coprire tutto e che nascondete con il resto del provvedimento. Mi riferisco al *bonus* che deve servire al Partito Democratico italiano per pagare con il denaro dello Stato una banca e comprarne due; al *bonus* che serve alla fusione tra Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, tax asset* (DTA), che non ha un preciso stanziamento di bilancio. È una norma a fisarmonica che potrebbe essere di 1, 2, 3, 4, 5, 6 miliardi, seconda di come poi si realizzeranno le fusioni in questo anno, e che dovrebbe servire a consentire al Partito Democratico, coprendo gli scandali del passato che stanno dietro il dissesto finanziario di Monte dei Paschi di Siena, acquisire finalmente, secondo le ambizioni da tempo della ditta di Bersani, Fassino ed eredi, non una, ma due banche in una,

poi c'è la manleva di 10,2 miliardi. Stiamo parlando, colleghi parlamentari, di qualcosa che denunceremo in ogni passaggio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Parliamo del più grande ammanco della storia della Repubblica italiana; italiana; di un salvataggio di Monte dei Paschi di Siena, che è già costato 5,7 miliardi quando fu fatta la nazionalizzazione,

Ebbene, nel 2017 già accadde, a fronte di una maxiperdita di oltre 11 miliardi di euro, di iscrivere nei bilanci 3 miliardi di euro di credito di imposta nel computo del capitale. Tale manovra è già stata effettuata dallo stesso Padoan nel 2017. Accadde

Qualcuno per questo cadde da una finestra. Recentemente la Camera ha deliberato una Commissione di inchiesta. Ebbene, per coprire quello scandalo l'allora Ministro dell'economia nazionalizzò Monte Paschi di Siena con una montagna di miliardi (5,7 prima, 3 miliardi dopo), 8 miliardi di crediti deteriorati furono acquistati da AMCO ed ora ci sono altri 3 miliardi almeno di DTA, almeno altri due miliardi e mezzo di ricapitalizzazione, altri 10,2 miliardi di manleva da garantire. A quanto ammonta il sacco che state preparando agli italiani? A quante decine di miliardi ammonta l'operazione di salvataggio della banca del Partito Democratico, che deve essere fusa con Unicredit e affidata a Padoan? Ho presentato un'interrogazione per capire come mai - sarà pubblicata domani domani - il ministro Gualtieri abbia sbianchettato una norma di direttiva europea, cancellandola dall'ordinamento per consentire a Padoan di superare fittiziamente e arbitrariamente con raggiro la norma sul conflitto di interesse e diventare oggi consigliere e domani presidente di Unicredit e Monte Paschi di Siena. Avete raggirato l'Europa; avete modificato e stravolto la normativa; avete sbianchettato il conflitto di interesse per realizzare il grande sacco sulla finanza e sulle banche italiane. Noi non ve lo possiamo consentire e non ve lo consentiremo. La manovra di bilancio serve solo a nascondere quell'operazione.

e alle imprese italiane delle regole che porteranno al *default* dell'impresa italiana, come hanno denunciato banchieri eccellenti. È una bomba cosmica sul sistema produttivo e la Banca d'Italia con il chiarimento di ieri mette una toppa peggiore del buco. Si tratta di uno sforamento di 100 euro per cittadino e di 500 euro per l'impresa, pari all'1 per cento di quello sforamento in novanta giorni. Almeno un terzo del sistema produttivo italiano incapperà in quelle regole e salterà. Di questo non vi interessa nulla purché vi appropriate delle due banche che questo siete ridotti: la finanza speculativa italiana è diventata la bandiera della sinistra italiana.

se la recessione economica preoccupa, non preoccupa meno la recessione democratica in atto. Le liberaldemocrazie stanno arretrando in tutto il mondo: non sono state mai così poche numericamente negli ultimi cinquanta I principi liberaldemocratici stanno arretrando nelle coscienze dei popoli d'Occidente. Questo ci dicono i sondaggi. Se esiste un termometro per misurare la febbre delle democrazie e l'insorgere di incombenze autoritarie e/o

popolare. Che il Parlamento vada difeso ce lo ricordano gesta recenti dei nostri amici e colleghi della maggioranza. Ce lo ricordano le sceneggiate, e parlo di sceneggiate perché evidentemente erano delle messe in scena che non afferivano a valori realmente avvertiti. Le sceneggiate del MoVimento 5 Stelle - le ricordiamo - sul tetto di Palazzo Montecitorio, brandendo copie della Costituzione in difesa del Parlamento della Repubblica, a quei tempi minacciato da governi che mai si sarebbero sognati di fare quello che questo Governo sta facendo oggi. Ce lo ricordano le gesta molto più recenti del Partito - cosiddetto - Democratico che appena due anni fa, esattamente in questi giorni di due anni fa, raccolse le firme di senatori attualmente seduti in questo emiciclo per presentare ricorso alla Corte costituzionale e per protestare contro la violenza subita da questo ramo del Parlamento, quindi dal Senato, da parte di un Governo (il Governo era il Conte 1) che aveva impedito a questo ramo del Parlamento di valutare, giudicare ed emendare l'allora legge di bilancio. Siamo oggi in condizioni analoghe a quelle, ma non mi pare che i colleghi della maggioranza avvertano tutto questo *pathos* democratico. Siamo in condizioni persino peggiori rispetto a quelle di allora, perché ce lo dicono i dati: degli oltre 430 atti di Governo relativi alla pandemia solo il 2,7 per cento ha avuto natura parlamentare; dei tanti decreti-legge approvati dal Governo il 62 per cento è passato con voto di fiducia. Il Governo si è degnato di rispondere ad interrogazioni e interpellanze parlamentari

assistiamo oggi a una manovra che nell'arco di ventiquattr'ore dovrà essere fintamente valutata, realmente approvata e di sicuro licenziata da questo ramo del Parlamento. Colleghi, siamo di fronte alla classica eterogenesi dei fini: un Governo nato per ristabilire gli equilibri costituzionali e democratici e dare lustro alla buona politica, coartata dalla cattiva demagogia, sta abusando di demagogia, non ha alcuna sostanza politica e sta mettendo sotto i piedi la Costituzione e la prassi democratica. Non so infatti se vi rendete conto che non solo nella storia repubblicana, ma nell'attuale cronaca d'Europa l'Italia ha raggiunto un nefasto primato: siamo il Paese in cui più il Parlamento è stato svuotato delle proprie funzioni Un liberale non dovrebbe dirlo, ma sono un liberale realista: si potrebbe anche accettare tutto questo; viviamo in uno stato d'eccezione e si può accettare che in uno stato di eccezione circoscritto nel tempo, in ragione di un'evidente e grave emergenza nazionale, i diritti e le prerogative costituzionali vengano compresse a favore di una maggiore efficacia ed efficienza del Governo. Non è questo il caso con tutta evidenza e non è un'opinione, ma sono i numeri a dirlo: siamo il Paese europeo con il maggior numero di morti per Covid; siamo il Paese europeo nel quale la recessione è più grave. Devono ancora essere promulgati il 64,5 per cento dei decreti attuativi, cioè di quegli strumenti, varati all'interno dei Ministeri, per dare concreta attuazione alle decisioni del Governo. una cosa talmente enorme che l'Ufficio per il programma di Governo, con grande scorno del sito Openpolis che svolge un'azione di trasparenza meritoria, ha smesso addirittura di pubblicare i dati di avanzamento dei decreti, aggiungendo così a una mancanza di spirito democratico, a un'evidente violazione dei diritti e delle prerogative parlamentari e a un'oggettiva incapacità ed inefficienza del Governo anche una rara e grave mancanza di trasparenza. Assistiamo così a una legge di bilancio che l'Ufficio parlamentare di bilancio racconta come un milleproroghe qualsiasi, una sequenza di interventi di natura puramente assistenziale che sono proiettati al presente, che nulla dicono del futuro e che mancano totalmente di senso politico. Se questo era, com'è ragionevole attendersi, un antipasto del Piano di ripresa e resilienza che il Governo varerà, è chiaro che non ci sarà alcuna ripresa e non ci sarà alcuna resilienza. Credo che senza democrazia e senza politica non potete e non possiamo pensare che questo Governo abbia un futuro. Credo che senza democrazia e senza politica

Signor Presidente, intervengo con riferimento ai quesiti posti da una serie di colleghi in relazione ad una correzione necessaria alla legge di bilancio. Confermo che è necessario un intervento normativo

100 euro, come già deciso per il secondo semestre del 2020, stabilizzando questa norma a decorrere dal 2021. La relazione tecnica, che fa riferimento ai valori corretti, quantifica

nel disegno di legge di bilancio che stiamo discutendo in questa sede, modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, cioè quello che ha previsto per il secondo semestre del 2020

scrivendo che nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione, di cui al comma 1 - che è però la detrazione relativa solo a sei mesi - spetta per le prestazioni a decorrere dal primo luglio 2020. Se rimane questo testo, la detrazione non è più di 1.200 euro a decrescere, con tutti i parametri che conoscete, ma diventa di 600 euro, cioè la metà. Questo è il punto. Quindi non solo non c'è un problema di copertura, ma se la norma rimanesse così come è scritta, avremmo circa 1.600.000.000 di euro che non verrebbero in realtà impegnati perché la detrazione, a norma di legge, sarebbe la metà di quella che era nell'intenzione del Governo e di quello che è scritto peraltro nella relazione tecnica che fa riferimento a 960 euro più 240, quindi 1.200, con tutti i parametri che conoscete. Per intervenire è necessaria una norma di legge e il Governo ha intenzione di farlo il prima possibile, sostanzialmente immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio, con un decreto-legge che interverrà in questo senso.

credo che quanto espresso dal vice ministro Misiani, che almeno dalle verifiche che stiamo facendo corrisponde alla realtà, possa chiamarsi davvero pressapochismo nelle norme. Può sfuggire infatti su un singolo emendamento da parte di un parlamentare in alcuni casi, però non su un provvedimento e per un'entità di questo genere su una manovra finanziaria. *(Applausi)*. Crediamo che la giustificazione e la soluzione proposta dal Governo in questo caso non sia peraltro corretta, perché la norma rende strutturale

voglio interloquire in modo molto sereno e voglio essere obiettivo. Possiamo discutere se la mancanza di copertura turba l'equilibrio di bilancio,

Non è possibile liquidare tutto ciò dicendo che non ci sono più fondi e che c'è la riduzione a 600 euro.

molto meravigliato - per non dire sbigottito - l'intervento del vice ministro Misiani che, purtroppo per lui, deve portare sulle spalle il peso della responsabilità collettiva di questa pessima figura. Vorrei rivolgermi non tanto a lui, quanto ai colleghi della maggioranza che ancora conservano un minimo di onestà intellettuale, chiedendo loro non è il momento di dire basta allo scempio delle istituzioni e del Senato in particolare. Colleghi, ci rendiamo conto del punto a cui siamo arrivati? Stiamo facendo in Senato, nel bel mezzo della discussione generale, un dibattito tecnico che andava svolto in Commissione, perché è in quella sede che si affrontano questi problemi, ma voi non ce l'avete consentito. Colleghi, questo non è più accettabile. Questo è il Senato della Repubblica e stiamo discutendo non di un provvedimento qualsiasi, ma del bilancio dello Stato.

Ma vi immaginate cosa può pensare di questo Governo e di questo Paese un investitore internazionale che, per sua sventura, sedesse oggi qui, in Senato, di fronte a un Esecutivo che, a quarantott'ore dall'esercizio provvisorio, sbaglia i conti della manovra

La fretta è conseguenza delle vostre divisioni, dei vostri litigi e dei ricatti all'interno della maggioranza. Ricordo che a definire scandaloso il metodo con cui al Senato è stato imposto questo *timing* non sono Luca Ciriani di Fratelli d'Italia o i colleghi di Forza Italia o della Lega, ma è stato il senatore Renzi non più tardi di ventiquattr'ore ore fa. Se è scandaloso per lui, lo è sicuramente anche per noi. dall'esercizio provvisorio, che sarebbe una tragedia non per il Governo, ma per le famiglie, i cittadini e le imprese, l'Esecutivo ci annuncia che deve ancora tagliare, cucire, aggiungere, ripensare e rivedere. Ora basta, siamo giunti a un momento e a un punto oltre i quali le istituzioni non possono essere calpestate. Mi rivolgo a lei, signor Presidente, perché faccia valere nelle sedi più opportune il grido di dolore che giunge almeno dai banchi dell'opposizione.

perché su una questione di questa importanza indubbiamente era necessario un intervento che non poteva ridursi alla sola replica, quindi grazie al Governo per questo chiarimento. ci risulta da alcune notizie che sono apparse o che circolano anche nei corridoi che non sia solo questo l'elemento del decreto-legge correttivo, ma che ci siano anche altre questioni, ad esempio il fatto che sia stata duplicata una norma che sostanzialmente era già contenuta ristori-*quater*, che comprendeva un po' tutti i decreti ristori, che è stata replicata anche sulla manovra di bilancio con due coperture differenti. Sembra cioè che i 50 milioni sul *quater* e i 50 milioni previsti sulla manovra di bilancio si sommino e che diventino 100 milioni. Questo riguarda l'intervento sugli affitti. Ricordo al senatore Errani che era uno degli interventi che la maggioranza si era prefissata di migliorare nella fase emendativa all'interno del Parlamento. C'è quindi questa duplicazione, anche se non penso che sia questo poi il tema principale. Qualcuno parla anche della questione legata ad una norma sull'istruzione

se sono anche altri gli eventuali interventi correttivi, ma mi pare di capire dal suo intervento che l'elemento principale resta questo. Io non ho motivo per

A questo punto, per chiarire bene la situazione nell'interesse degli italiani - questa è la cosa principale - abbiamo bisogno che sia lei, a darci, dopo una valutazione attenta, la chiarezza della norma per capire se effettivamente non c'è bisogno di un ulteriore scostamento e di un ulteriore passaggio alla Camera, ma sia solo sufficiente un decreto correttivo. So che lei è sempre molto attenta nel verificare anche i maxiemendamenti, direi che una verifica ulteriore su questo maxiemendamento è necessaria prima ancora che il Governo ponga la fiducia, così almeno facciamo le cose fatte bene, perché non vorremmo trovarci a votare la fiducia

precisione e con grande trasparenza, come era doveroso fare in quest'Aula, perché di fronte ad un quesito come quello che è stato posto era corretta una risposta del Governo. Credo che la risposta sia trasparente e precisa e mostri anche il volto delle difficoltà all'interno delle quali il Governo si sta muovendo per gestire - e io credo che questo sia un punto politico essenziale che anche tra di noi dovremmo cominciare a condividere una situazione emergenziale, per attraversare una pandemia come questa, che ha avuto bisogno di una quantità di provvedimenti molto ampi, composti da numerosi articoli e commi, dove l'errore tecnico non è qualcosa che può essere attribuito io dico - politicamente, con responsabilità politica nei confronti del Governo e della maggioranza, perché amministrare il Paese e governarlo per attraversare questa crisi richiede inevitabilmente l'assunzione di una pluralità di responsabilità. Qui il vice ministro Misiani ha correttamente riportato una decisione altrettanto responsabile del Governo, assunta ad invarianza di saldi, nel pieno rispetto dell'equilibrio di bilancio, e dunque nel pieno rispetto della legge di bilancio sulla quale stiamo intervenendo, quindi senza modifica degli equilibri e dei saldi di finanza pubblica, perché la matematica ancora non è un'opinione: se quella norma aveva un tiraggio di 3,3 e così come è scritta ha un tiraggio di 1,6, è inevitabile che la correzione serve per poter applicare la volontà politica del Governo, che peraltro era già stata in diverse occasioni ribadita e sottolineata. Lo dico con estrema amicizia e anche con grande senso di responsabilità nei confronti del collega Pichetto Fratin. Sappiamo che ci uniscono la volontà di approfondimento e di entrare nel merito. Io credo che, di fronte a questo chiarimento che il Governo ci ha portato, non ci sia bisogno di entrare in ulteriori elementi di valutazione tecnica. È stato dichiarato qui dal vice ministro Misiani che il tutto avviene ad invarianza di saldi e nel pieno rispetto degli equilibri. Per quello che ci riguarda, questa è una bella pagina di relazione tra Governo e Parlamento e anche per noi è un elemento di estrema chiarezza per poter continuare, nella legalità, nella regolarità e nella piena assoluzione della responsabilità politica, il nostro lavoro e il nostro dibattito.

il Capogruppo della Lega ha preso atto della risposta del Governo. Risposta doverosa, a fronte di notizie che potevano lasciar pensare al rischio di un problema relativo alla tenuta dell'equilibrio di bilancio. Questo problema non esiste. Non esiste un problema di copertura. Anzi, c'è esattamente il problema opposto, collega Pichetto

è un errore. Qui c'è stato un errore che va corretto, ma va corretto senza che si metta in discussione la correttezza del bilancio, la possibilità di approvarlo e di evitare l'esercizio provvisorio. Dunque, nonostante tutta l'attenzione, che non ho dubbi il Presidente del Senato metterà, non c'è la necessità di un intervento del Presidente del Senato, perché, da questo punto di vista, le cose sono chiare e trasparenti. trasparenti. Poiché io ho apprezzato, come detto anche in diversi interventi, che l'opposizione ha lavorato per evitare l'esercizio provvisorio, nonostante i tempi strettissimi, proporrei di procedere, dopo la sanificazione, con il nostro dibattito per l'approvazione del bilancio. finestra"). Vice ministro Misiani, io le pongo una domanda diretta, tenendo conto di quanto alcuni componenti di questo Senato hanno asserito: in questo provvedimento c'è copertura oppure no? Per cortesia, dia proprio una risposta secca: la copertura c'è, sì o no?

La norma, così come è scritta, invece, costa la metà di quella cifra. Quindi, c'è una sovracopertura di 1,649 e rotti

sull'equilibrio di bilancio. Il vice ministro Misiani oggi assicura che non c'è alcun problema di copertura. Alla luce di questo, del parere della 5a Commissione e del parere del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, io devo ritenere che la procedura sia corretta. Del resto noi verificheremo poi, attraverso proprio il decreto correttivo, se quello che è stato detto corrisponderà al vero.

Francesca Salvetti. Era entrata nei ruoli del Senato solo nel 2005, ma in pochi anni era diventata una delle colonne portanti della segreteria della Commissione difesa. Donna brillante e di vivace intelligenza, lavoratrice instancabile, competente e sempre disponibile, la signora Salvetti era soprattutto una ragazza piena di energie e di vitalità. e la sua capacità di affrontare le mille difficoltà quotidiane del lavoro parlamentare con spirito sempre costruttivo e senza mai perdere il sorriso l'avevano resa un punto di riferimento importante tanto per i senatori quanto per i colleghi. Quello stesso sorriso e quella stessa incredibile energia con cui la signora Francesca Salvetti ha affrontato la terribile malattia che l'aveva colpita poco più di due anni fa, subito dopo essere diventata mamma per la seconda volta. La notizia della sua prematura scomparsa è stata motivo di forte dolore. Con la signora Salvetti, il Senato non perde soltanto una collaboratrice preziosa, ma una bella persona a cui tutti erano affezionati, una ragazza in gamba, generosa, solare, dinamica e combattiva. Sono vicina alla famiglia, al marito Giovanni, ai piccoli Matilde e Leonardo, a cui rinnovo il mio cordoglio personale e sentimenti di affettuosa e commossa partecipazione, a nome di questa Assemblea e di tutto il Senato. In ricordo della signora Francesca Salvetti, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, arriviamo alla discussione di questa manovra di bilancio con la consapevolezza di aver già pagato il tributo più alto che possa toccare a un Paese e a una comunità. Portiamo sul cuore il peso delle vite umane perdute e sulle spalle l'onere di una congiuntura nefasta ed emergenziale. La fine del tunnel ancora non si vede, eppure abbiamo il dovere di immaginarla e di intuire come raggiungerla. Il Governo ha scelto di muoversi lungo un percorso a tappe che con oggi traguarda il nono provvedimento economico finanziario negli ultimi dieci mesi di legislatura. Ognuno ha completato il precedente, lo ha arricchito o anche solo corretto in meglio e l'attuale comincia finalmente a porre le basi per guardare oltre la pandemia, per vedere la ripresa oltre la crisi. Quando si parla di ripresa, inevitabilmente si finisce per parlare di lavoro, che è tema centrale di questa manovra anche grazie al rapporto costruttivo che si è venuto a creare con le forze di minoranza. Nel testo all'esame dell'Aula si è cercato di equilibrare politiche di sostegno al reddito e all'impresa con politiche attive di rilancio del sistema produttivo ed economico in generale. Registriamo infatti il prolungamento di dodici settimane degli ammortizzatori sociali e l'inserimento di considerevoli risorse sugli sgravi contributivi, sia per il lavoro dipendente che per quello autonomo, e per la prima volta i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata avranno la possibilità di un'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Questo è un passo importante sulla strada della riforma degli ammortizzatori sociali che è già nell'agenda del Parlamento per il prossimo futuro. Capitoli importanti della manovra sono riservati poi ai pensionati e agli esodati, ai cosiddetti lavoratori fragili e alle donne cui è dedicato in particolare il fondo per la parità salariale che è una sorta di implicito impegno del Parlamento a legiferare in materia. Investimenti per il futuro sono anche l'assegno unico universale per le famiglie con figli cui sono riservati oltre tre miliardi di euro, l'assegno di ricollocazione non soltanto a chi percepisce il reddito di cittadinanza ma anche ai cassintegrati e ai disoccupati in Naspi, e il contratto di espansione che in un mercato in trasformazione si pone come una sorta di patto generazionale. È evidente che in molti casi citati e in altri che mi manca il tempo di ricordare, ci troviamo di fronte al momento di avvio di politiche che dovranno poi trovare esplicitazione e concretezza. Penso, ad esempio, allo scostamento di bilancio che servirà nei prossimi mesi a rafforzare le maglie nella rete dei ristori intessuta per salvaguardare chi ha patito di più gli effetti della crisi generata dalla pandemia. Urge infatti cominciare a ragionare per filiere produttive e rivedere il concetto di attività prevalente rispetto a come è stato applicato sin qui, in modo da evitare che nell'elenco dei destinatari delle misure, taluni operatori risultino indebitamente eclissati. Da un lato, dunque, l'odierna legge di bilancio manda in porto i risultati attesi, dall'altro intraprendere nuove sfide e nuovi traguardi. Il tutto anche grazie a un mutato contesto europeo, all'interno del quale questo Governo ha saputo far tornare l'Italia tra i protagonisti. Vorrei concludere ricordando che, ancora sul tema del lavoro, proprio dall'Europa arriva l'eco di una proposta cruciale, con la quale presto saremo chiamati a confrontarci, relativa al tema dell'equa retribuzione. Si tratta di una proposta orientata a stabilire prescrizioni comuni nell'Unione affinché si tenda a una convergenza verso l'alto dei salari minimi, qualunque sia il sistema con cui essi vengono determinati nei Paesi membri. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Intorno a questo obiettivo sta maturando una direttiva che non può e non deve coglierci impreparati, a maggior ragione per l'intenso lavoro che il Senato, in particolare, ha già svolto sull'argomento nel corso dell'attuale legislatura. Quindi, nel ragionare di bilancio, di rimedi e soprattutto di futuro, è bene metabolizzare che una decisione va presa, e va presa anche alla svelta, perché possiamo accompagnare il cambiamento invece di subirlo. rappresentanti del Governo, colleghi, sulla procedura vi ricordo che esiste la legge del contrappasso: quello che fate oggi alle opposizioni o al sistema potrebbe, un giorno, ritorcersi contro di voi con gli interessi. Il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio dice che l'aumento del PIL, che voi ipotizzate nel 6 per cento, in realtà sarà almeno di un punto inferiore, e io aggiungo che probabilmente, invece, la diminuzione di quest'anno non sarà 9, come previsto, ma, purtroppo, qualcosa in più. Sempre il parere dice che è parzialmente indefinita la struttura del bilancio: non c'è un equilibrio tra le voci e c'è incertezza. Inoltre, gli 88,5 miliardi del

come fonte di copertura 2022-2023 è incerta e scorretta (andrebbe a finanziare la riforma fiscale); eventualmente gli utili derivanti da manovre fiscali da investimenti vanno nel bilancio a rendere quella omogeneità e quella maggior definizione di cui si è rimproverati. Sono 40 miliardi di *deficit*, ma sono 73,6 di fabbisogno; gli scostamenti sono a parte. Gli scostamenti sono già 108 e abbiamo altri 20 miliardi in vista.

disposizioni anche in contraddizione e di difficile attuazione. Sul 110 per cento ho sentito prima da un collega che proporrete una proroga ulteriore perché giugno 2022 non basta; bisogna andare almeno a fine 2023, altrimenti non parte - ve lo dico come constatazione, riporto le idee degli operatori del settore - ed inoltre, va semplificato. Avete fatto tanti rinvii, però le cartelle fiscali prima o dopo arriveranno e, a mio avviso, l'Agenzia delle entrate scalpita - e anche troppo - nelle dichiarazioni. Andrebbe in qualche modo tacitata con un provvedimento. Il blocco degli sfratti al 30 giugno, già citato dal collega Caliendo, mi fa pensare che ce l'abbiate comunque con i proprietari di casa, che hanno investito e non hanno rubato gli alloggi o gli investimenti immobiliari. Il divieto di licenziamento lo pagheremo caro, purtroppo, dopo il 31 marzo.

ma l'Europa la ascoltate quando volete, e quando non vi interessa, non la sentite. Perché ci deve essere un costo di miliardi a carico dello Stato per fare *cashback* quando uno può pagare come gli pare? Se poi vuol pagare con la carta di credito fa benissimo.

i sistemi di filtraggio dei rubinetti vanno nelle agevolazioni per le ristrutturazioni; sull'acqua ci sarebbe molto da dire, ma forse conta un'opera educativa.

politica industriale predomina il concetto di nazionalizzazione, come ha detto prima un collega; mi astengo dal commentare le questioni del Monte dei Paschi o della Whirlpool, che però chiude (le avete dedicato mesi, dicendo che avreste risolto il problema). I ristori hanno importi troppo bassi, che non risolvono nessun problema; dovevate chiedere istruzioni alla Merkel, quella che vuole comandarci: ha indennizzato tutti di tutto il fatturato che hanno perso, però poi comanda in Europa e comanda anche su di noi, ma i vaccini li acquista in proprio.

quel problema contabile di cui si è parlato prima potreste anche decidere che quegli 800 milioni, invece di essere destinati all'assalto della diligenza con il *bonus* occhiali, *smartphone,* *cargo bike,* coltelli per i cuochi, possano andare per l'alluvione (il mio è un suggerimento).

facciano chiaramente: siamo in difficoltà, abbiamo problemi serissimi, forse abbiamo anche sbagliato, lo si può riconoscere, però vi chiediamo un sacrificio per efficientare al meglio la sanità, per portare a termine la vaccinazione e per gestire

In conclusione, bisogna produrre in Italia: il manufatturiero, che era ed è forte, non va ammazzato; l'agricoltura deve difendere i nostri interessi, i nostri prezzi e non perequare ad Est; la Gran Bretagna lo farà del 2021. Sono necessarie poche norme, semplici e chiare: anno bianco fiscale, come dice Forza Italia, allora avremo più entrate e più occupazione

la proroga di opzione donna e il rinnovo di APE sociale, la spinta al mercato del lavoro nel Sud Italia (con un regime di fiscalità di vantaggio per le imprese del Mezzogiorno, che possono così continuare a godere di uno sgravio del 30 per cento dei *bonus* bebè, il potenziamento del reddito di cittadinanza e dei relativi controlli. La misura su cui vorrei soffermarmi, in cui credo fortemente fortemente e alla cui redazione ho contribuito, collaborando con i colleghi di Camera e Senato e con i membri del Governo in un grande sforzo collettivo e comune, è l'ormai noto superbonus. Ne sono particolarmente orgoglioso. È uno strumento di rilancio e di sviluppo che consente di ottenere una detrazione fiscale superiore alla somma spesa. Tale misura ha dato nuovo impulso all'edilizia privata e ha messo insieme - cosa mai accaduta nella storia di questa Repubblica - il mondo produttivo, l'edilizia, le associazioni ambientaliste, i sindacati, i professionisti, le banche e la finanza, realtà che non si erano mai sedute allo stesso tavolo e che ora spingono tutte insieme a supporto di questa visione di Paese. Abbiamo potenziato questa misura con l'allargamento temporale: l'abbiamo prorogata a metà 2022 e, addirittura in alcuni casi, al 2023. Sicuramente l'anno prossimo con il nuovo scostamento di bilancio troveremo i fondi per allargare a tutti questa misura fino al 2023. È un punto d'onore di questa maggioranza e un impegno che ci prendiamo adesso e che porteremo a compimento. gli ulteriori miglioramenti di questa misura. Per i cittadini abbiamo gli edifici collabenti, che prima non potevano fare superbonus, mentre adesso possono; abbiamo inserito gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche; abbiamo aggiunto per questi interventi anche le persone fisiche proprietarie di fabbricati fino a quattro unità immobiliari, che prima erano escluse. Abbiamo permesso di aumentare le somme per il sisma *bonus* di aumentare le somme per il sisma *bonus* fino al 50 per cento per coloro che sono stati colpiti da sisma dal 2008 in poi e per i Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Per i sismi verificatisi dal 1° aprile 2019 gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Abbiamo fatto inoltre un intervento molto mirato sulle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, perché il il *driver* principale dell'espansione della mobilità elettrica è l'avere a casa una colonnina di ricarica, oltre che trovarla sulle strade. Abbiamo inserito quindi un intervento mirato per le colonnine di ricarica, prevedendone una per ogni unità immobiliare nel superbonus al 110 per cento. Abbiamo rimodulato la normativa, la normativa, che fa il paio con un'altra, la quale prevede che ogni 50 chilometri nella rete autostradale debba essere presente almeno una colonnina di ricarica. Stiamo dando un impulso alla mobilità elettrica.

- ancora parlano di trivelle, inceneritori e grandi opere inutili (che sono grandi sprechi di denaro pubblico) oppure di lavoro, senza capire che ha bisogno di persone qualificate - è su formazione e riqualificazione che si giocherà la sfida più importante - che noi parliamo invece di digitalizzazione, idrogeno, intere filiere produttive riconvertite al *green,* *reshoring* produttivo e telemedicina. Vorrei che queste due visioni così distanti trovassero un punto d'incontro. Questo è un punto che dobbiamo perseguire per il bene del nostro Paese. Sono pronto e tutto il MoVimento 5 Stelle lo è. Incontriamoci e parliamo seriamente del futuro di questo Paese. Con questo spirito, auspico che

Signor Presidente, mi consenta di iniziare con un pensiero ai cittadini croati colpiti da un forte terremoto di un'esperienza che personalmente ho vissuto più volte e capisco perfettamente come possano sentirsi. Le scosse, tra l'altro, sono state avvertite chiaramente anche in Italia, con numerose chiamate alla Protezione civile e richieste di assistenza.

Venendo alla discussione in oggetto, oggi ci troviamo a intervenire su quella che dovrebbe essere una delle leggi più importanti in assoluto approvate dal Parlamento, quella fondamentale dello Stato: la legge di bilancio. Uso il condizionale perché in realtà, purtroppo, non è più così. Alcuni colleghi si sono lamentati che il nostro è diventato una sorta di sistema monocamerale.

In un sistema monocamerale, infatti, almeno una delle due Camere decide. Attualmente, invece, ci ritroviamo sempre più spesso a dover convertire in legge decreti-legge su cui il Governo

a fianco a un eccesso di decreti-legge, ci ritroviamo anche un proliferare di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, atti amministrativi con cui il Governo ci priva delle nostre libertà fondamentali e dei nostri diritti costituzionali, che tra l'altro esulano completamente dal controllo, dalla vigilanza e dalla possibilità di intervento del Parlamento. Quindi, in questa fase il Parlamento nella sua interezza, non in una delle due Camere, viene privato anche del potere attribuito dalla Costituzione, cioè quello legislativo. La maggioranza obietta che questa è una necessità determinata dalla situazione contingente, ma non è vero, perché, se vediamo i criteri con cui verrà nominato il comitato per la finanza ecosostenibile, criteri fissati dalla legge di bilancio, troviamo di nuovo il DPCM. Ma come? L'Assemblea aveva stigmatizzato l'abuso di questo strumento, la stessa maggioranza aveva auspicato che non avvenisse e, come criterio di nomina di un comitato, che sarà fondamentale nelle decisioni future del Governo e nell'impiego delle risorse fondamentali per la nostra economia del *recovery fund*, troviamo di nuovo il DPCM? Quindi, o qualcuno sta prendendo in giro il Parlamento, oppure non si dà il giusto valore alle dichiarazioni che vengono fatte in Aula. Questo è gravissimo, perché quello che diciamo qui non è rappresentanza di un parere personale, ma quello per cui il popolo ci ha chiamato a intervenire, a perorare appunto quelle cause. Sono un appassionato di storia, quindi potrei ricordare e pensare che non è una novità per l'Italia far ricorso - come ho detto prima - a fasi dittatoriali e a dittatori. dittatori. Nell'antica e gloriosa storia di Roma, ad esempio, quando ci si trovava a vivere una crisi importante, per cui le soluzioni abituali non erano sufficienti, si nominava un dittatore. Quindi già 2.500 anni fa

definito analfabeta istituzionale. A fronte della nostra storia, ci troviamo ad aver incaricato un dittatore definito analfabeta istituzionale. *(Proteste).* Colleghi, non ce l'ho chiamato io.

riguardo alle dichiarazioni del collega Renzi. Questo però può significare solo due cose. La prima è che il Governo Conte è finito, perché, se una forza di maggioranza pensa che il proprio Presidente del Consiglio sia un analfabeta istituzionale, evidentemente gli ha tolto la fiducia. La seconda, in alternativa, significa che Italia Viva è disposta a qualunque cosa, pur di rimanere al Governo. *(Applausi)*. Il prossimo futuro ce lo dirà. Il presente però ci lascia con un Presidente del Consiglio dei ministri preoccupato più per la propria immagine che per le proprie misure, che sono quasi sempre *spot*, a dimostrazione del fatto che va in televisione ad annunciarle, prima ancora di venire in Parlamento e illustrarle a noi. Misure *spot* come era il *click day*. *(Applausi)*. Misure *spot* com'è il *cashback*, per cui si è annunciato che si sarebbero restituiti agli italiani 150 euro a persona ed emerge che, con la dotazione finanziaria prevista, al massimo arriveremo a un terzo. Tuttavia, non avendo imparato nulla da questo, si introduce il *bonus* idrico,

Si sono mortificati i Comuni. Nella manovra è prevista la possibilità di ottenere un finanziamento per l'efficientamento termico delle scuole, escludendo però i Comuni. Ho avuto il privilegio, l'onere e l'onore di indossare la fascia tricolore per tre mandati ero in trincea, come tutti colleghi sindaci: tutti i colleghi sindaci, quelli che danno le prime risposte alla popolazione, si vedono esclusi dai finanziamenti per le scuole. *(Applausi)*. Per tale ragione avevo presentato un ordine del giorno, che è stato bocciato. dall'Imu: avevo chiesto, sempre con un ordine del giorno, l'esonero per le case distrutte dal terremoto; dal 2022 si tornerà a pagarla su case che non esistono più. Lo dimostrano tante altre misure demagogiche e senza senso, come il finanziamento alle associazioni che danno assistenza alla fauna selvatica. Benissimo,

dissesto idrogeologico, uno dei problemi della nostra Nazione: lo vogliono risolvere con assunzioni a tempo determinato, che scadranno fra un anno. Vi è poi il superbonus, su cui si soffermeranno altri colleghi. Ci sarebbe ancora tanto da dire. Vi ringrazio per l'attenzione e speriamo che le nostre proposte di buonsenso

da ridere a trovarsi oggi, 29 dicembre, a dover votare una legge di bilancio per il prossimo anno quasi senza aver avuto nemmeno la possibilità di discuterla e visionarla. Ci sarebbe ancor più da ridere, cari colleghi, se pensiamo che, mentre l'opposizione interviene in quest'Aula nel merito del provvedimento in esame, che riguarda il programma economico e sociale del Governo per il 2021,

parte di questa maggioranza, ieri abbia presentato, con tanto di *slide*, quello che i giornali hanno definito un nuovo programma economico, ben differente da quello che il Governo attuale vuole presentare agli italiani. ci sarebbe davvero da ridere, colleghi, ma noi, che siamo un'opposizione seria, che mette al primo posto gli interessi degli italiani, in queste ore vediamo troppi nostri connazionali piangere per le conseguenze di ciò che avete fatto negli ultimi mesi e di ridere non abbiamo proprio voglia.

Quali sono, dal punto di vista tecnico, i provvedimenti adottati per aiutare quelle categorie che la pandemia ha distrutto e che rischia quasi di far sparire?

devono combattere sempre più contro la concorrenza sleale di piattaforme straniere che in Italia fanno il bello e il cattivo tempo? Quali sono le scelte che potranno aiutare gli operatori turistici italiani, che sono sempre più in ginocchio e non sanno come riuscire a sopravvivere a questo infinito periodo? Quali decisioni avete preso, colleghi della maggioranza, per aiutare gli enti locali che nei prossimi mesi dovranno affrontare spese correnti sempre maggiori per far fronte alla crisi sociale, mentre le entrate saranno estremamente minori, a causa di una crisi sociale che tutti potevano prevedere, ma che voi non siete in grado di contrastare?

Avete preparato un pacchetto di provvedimenti, in parte anche condivisibili, in cui emerge la vostra unica ossessione, che è quella di continuare a sopravvivere. Ho letto ogni capitolo del provvedimento in esame e, quando ho visto che ancora trovate centinaia di milioni di euro per il reddito di cittadinanza (previsto addirittura fino al 2029,

e la capacità di ammettere che il rilancio del Paese deve passare attraverso la ricchezza prodotta dal lavoro, dalle imprese, dagli artigiani, dalle partite IVA, dai commercianti,

manca il coraggio di dire agli italiani che avete fallito; manca il coraggio di dire al Paese che avete sbagliato; manca il coraggio di dire che negli ultimi mesi avreste dovuto pensare a come salvare il Paese e non avete fatto altro che pensare a come salvare le vostre poltrone. Certo è che il vostro tempo politico è ormai finito e gli italiani, che l'hanno capito, quando verranno chiamati al voto, sapranno a chi affidare la guida del Paese, e non sarete certamente voi.

un quarto delle misure di questa legge di bilancio, praticamente 7,6 miliardi, è legato al finanziamento di misure emergenziali per i settori che stanno ancora scontando questa gravissima crisi. Parliamo di sostegno a imprese e famiglie, ma soprattutto ai settori del turismo, della cultura e dello spettacolo, nonché delle risorse per la scuola e i trasporti pubblici, a cui dobbiamo aggiungere anche i 18 miliardi dei vari decreti ristori: ritengo quindi impensabile impensabile dire che l'Italia non ha messo in atto una risposta fiscale adeguata. È stata la seconda risposta più grande d'Europa per entità e per dimensione, quindi credo che qualsiasi accusa che la risposta economica dello Stato non sia stata adeguata sia da rigettare assolutamente. I restanti tre quarti della manovra (23 miliardi) vanno a finanziare invece interventi non emergenziali. Va detto che il testo è stato migliorato enormemente, anche grazie al lavoro di Italia Viva, che, oltre alla defiscalizzazione dei contributi dei lavoratori autonomi e delle partite IVA per quasi un miliardo, ha ottenuto un'indennità di non occupazione anche per i piccoli autonomi. Oltre all'aiuto ai lavoratori autonomi che in questi mesi hanno perso un terzo del loro reddito, voglio sottolineare ed evidenziare anche un importante risultato ottenuto sul congedo di paternità obbligatorio, che passa da sette a dieci giorni. Un altro importante contributo di Italia Viva è arrivato sul credito di imposta per le minusvalenze del PIL, i piani individuali di risparmio, validi solo per il 2021, per cercare appunto di incentivare gli investimenti nelle piccole Penso anche alla proroga dell'implementazione della *plastic tax* e della *sugar tax* al 2022, appunto per permettere alle aziende di riconvertirsi nella produzione di materiali più eco-compatibili e nella produzione di sostanze che non favoriscano l'obesità infantile, una missione che è stata resa ancora più complessa dalla pandemia. Sempre per parlare di cose concrete, nel merito, il nostro supporto a queste aziende per avere più tempo per riconvertirsi è più che tangibile. In questi mesi, Italia Viva sta restituendo il senso di una politica che sa ascoltare: ascolta le parti sociali e il grido di dolore che arriva da molte categorie e prova a trovare risposte, perché continuare ad alimentare l'idea di una politica lontana dalla vita delle persone, che non guarda e non ascolta, è sbagliato. Solo qualche minuto fa è arrivato l'ennesimo grido d'allarme lanciato da Confindustria, che prega il Presidente del Consiglio di fare uno sforzo in più per dare risposte al motore produttivo del Paese, che attende con speranza di avere una visione strategica per la rinascita da qui ai prossimi vent'anni. Il *recovery plan* è un'occasione storica e le sue immense opportunità non devono essere usate per distribuire alla cieca risorse che non avremo mai per i prossimi cento anni. consegnando agli italiani un programma strategico-operativo per l'utilizzo corretto di quelle risorse, Italia Viva ha dimostrato cosa vuol dire fare politica ed esercitare la democrazia con la forza delle idee, anche in contrasto con le altre forze politiche della maggioranza. Si è assunta una responsabilità. Ora spetta al presidente Conte fare tesoro della bontà dei nostri suggerimenti. Le idee di una forza della maggioranza vanno rispettate e, qualora non condivise da tutto il Governo, vanno comunque motivate. Le nostre proposte sono concrete e realizzabili, frutto di un'attenta e costruttiva elaborazione politica dei contributi che arrivano dal mondo delle imprese, dagli autonomi, dalle partite IVA, dalla scuola, dalla cultura e dal turismo: sono idee che possono trasformarsi in realtà e sono condivise, sì, da un silenzio-assenso di molti parlamentari di quest'Aula, da destra e da sinistra. Concludo, signor Presidente, facendo un'ultima riflessione, che il *Premier* e la maggioranza ne facciano tesoro. In questo caso, mi preme sottolineare

Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, la legge di bilancio che oggi stiamo discutendo affronta la situazione economica più difficile dalla Seconda guerra mondiale. Sarebbe stato necessario far fronte a questo grave momento proponendo una chiara visione su come aiutare gli italiani a risollevarsi al più presto dalle gravissime difficoltà in cui versano. Ci saremmo aspettati un progetto coerente, in considerazione delle ingentissime risorse a disposizione del Governo, ottenute anche grazie all'opposizione, che ha votato scostamenti di bilancio, senza essere obbligata a farlo, per 140 miliardi. Al contrario, purtroppo, mancano completamente un progetto di futuro e un'idea di società. Avete vanificato i sacrifici degli italiani in un'accozzaglia di misure raffazzonate e incoerenti, disperdendole in centinaia di *bonus*. Finanziate persino la propaganda *gender* nelle scuole, erogando tre milioni di euro alle associazioni LGBT. L'unica cifra che emerge è l'improvvisazione, frutto di vecchie logiche assistenziali e clientelari. Voi, cari colleghi, state spendendo risorse prese in prestito dalle future generazioni. Sarebbe stato vostro dovere concentrarle per sostenere le attività produttive, sbloccare i cantieri e gli investimenti in infrastrutture, il lavoro autonomo come quello dipendente. Invece, avete fatto un piano senza anima. Non lo diciamo noi, ma Renzi, che fa parte della vostra maggioranza. Avete fatto un *collage* raffazzonato, che non risponde alle esigenze degli italiani. Vi abbiamo chiesto di ridurre le tasse e di sospendere, ad esempio, il pagamento di 31 milioni di cartelle esattoriali che stanno arrivando agli italiani, già prostrati ed esausti. Ma voi, niente. Avete però trovato il modo di agevolare ancora una volta gli immigrati, abolendo la tassa sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo dei cosiddetti *money transfer*.

fiume di denaro guadagnato in nero, frutto molto spesso di attività illecite. Sappiamo benissimo che ad esempio, attraverso i *money transfer*, vengono trasferiti all'estero i fondi della mafia nigeriana. Lo sapete, cari colleghi, qual è l'importo *pro capite* che ogni nigeriano presente in Italia trasmette all'estero ogni anno? 11.806 dollari. Ed è una cifra ricavata da un'inchiesta di qualche mese fa della Gabanelli pubblicata sul «Corriere della sera», non di qualche cattivo sovranista. sovranista. Ogni nigeriano, oltre a sostentarsi, riesce a risparmiare in Italia quasi 12.000 euro: gli italiani dovrebbero imparare dai nigeriani come si fa a fare i soldi. L'uso dei contanti, però, lo prevedete per loro, ma non per noi, in modo che i loro loschi affari continuino come sono continuati fino a oggi. Per venire alla giustizia, che è la materia di mio principale interesse, la situazione è ancora peggiore, se possibile. Nel triennio 2021-23 non ci saranno interventi di rilievo: le

di giustizia e di buon senso, secondo la quale le spese legali di chi è assolto in un processo penale debbano essere restituite dallo Stato che ha inquisito ingiustamente quel cittadino - non sia adeguatamente finanziata. Eppure sappiamo benissimo che la condizione della giustizia italiana è fondamentale per consentire di venire

anche nel 2021 non verrà assolutamente diminuita, a prescindere ovviamente dalle difficoltà dell'amministrazione della giustizia che dipendono dall'emergenza Covid. Covid. Cari colleghi, vorrei concludere con una considerazione. Vedete, la questione sanitaria non è indipendente da quella economica. Ormai abbiamo capito benissimo che l'economia ripartirà soltanto quando ci saranno le condizioni sanitarie perché la società possa riprendere a camminare e gli investimenti e il lavoro possano riprendere. Mentre le altre grandi Nazioni come la Germania, il Regno Unito gli Stati Uniti stanno procedendo di gran passo attraverso la vaccinazione di centinaia di migliaia o di milioni di loro concittadini, noi oggi non abbiamo nemmeno ancora un piano chiaro e preciso di come saremo in grado di farlo. Oggi si chiude il bando per assumere il personale sanitario che sarà necessario per le vaccinazioni. Allora ha fatto bene la presidente Giorgia Meloni a chiedere che il Governo renda pubblico, giorno per giorno, come procedono i vaccini. *(Applausi)*. È una questione fondamentale non soltanto per la salute degli italiani, ma anche per la ripresa vera della nostra economia, che non può rimanere indietro, a causa della vostra incapacità, rispetto alle economie degli altri grandi Paesi europei e occidentali.

è la prima volta che intervengo sulla legge di bilancio, quindi il timore di dire qualche inesattezza c'è, ma il signor Vice Ministro me lo perdonerà e cercherà di cogliere il senso generale dell'intervento.

cosiddetto patrimonio privato, che ammonta più o meno a 10 *trillion*. Queste sono due riflessioni che, secondo me, dovremo fare molto a breve e che anzi avremmo già dovuto fare.

crediti non riscossi, nelle loro diverse categorie - non chiamiamolo condono, ma una sanatoria intelligente - così come non vedo, dall'altra parte, un contributo straordinario. Riporto gli indici di Oxfam,

strutturale della microimpresa a reperire professionalità digitali, in grado di sostenere la crescita e la competitività. Aggiungo peraltro un dato veramente preoccupante, relativo al fatto che la scarsa offerta di competenze si accompagna ad una debole domanda da parte delle imprese e questo è un dato che deve far riflettere. In secondo luogo, ho visto tanti fondi oltre ai *bonus*, tra cui mi pare ci sia anche un Fondo per la creatività.

dunque potuto pensare ad una sorta di credito di imposta, che incentivi gli imprenditori a manutenere il capitale umano, perché la manutenzione del capitale umano

occorre attingere per far nascere un'economia innovativa, flessibile, duttile e molto veloce, anche a servizio della media e grande impresa. Credo che ormai siano maturi i tempi per pensare e sostenere una nuova generazione non solo di incubatori, ma di incubatori e acceleratori, con cui prima aiutiamo queste realtà e poi le acceleriamo verso il mercato. Tutto questo all'interno di ecosistemi, che che possiamo anche immaginare a livello regionale, se ci sono le condizioni, per dare servizi, spazi fisici e relazioni di *networking* e per incentivare il cosiddetto sviluppo dei processi di innovazione aperta, per favorire non solo le economie locali, ma anche l'economia nazionale.

intravedere nella legge di bilancio. Questo ci fa preoccupare molto, per l'indirizzo strategico che l'Italia vorrà dare a se stessa e non solo, anche a livello di Unione europea. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, quella al nostro esame è una legge di bilancio in cui vediamo risorse economiche disperse in mille rivoli, alcuni anche fantasiosi o quantomeno di scarso impatto sul vissuto quotidiano dei cittadini. Trovano invece poco spazio investimenti per i lavoratori fragili, categoria di persone della quale abbiamo parlato in più occasioni, ma che a fatica viene ascoltata: malati oncologici, trapiantati, immunodepressi, la cui salute è posta ulteriormente a rischio, se esposti al contagio Covid sul posto di lavoro o sui mezzi pubblici usati per recarvisi. Ci sarebbe lo *smart working*, ma questa possibilità non è però accessibile per chiunque per via delle mansioni che spesso non possono essere modificate, stante la natura e la tipologia delle aziende per cui gli interessati lavorano. Per questo è indispensabile che venga assicurata la possibilità di assentarsi dal lavoro senza che ciò impatti sul comporto, ossia il totale dei giorni di assenza possibili nel corso dell'anno. Durante l'esame della Camera è stata posta parziale soluzione al mancato intervento del Governo, e lo si è fatto solo grazie alle pressioni della Lega e delle altre forze di opposizione; in particolare, oltre al sottoscritto, grazie alla senatrice Nisini e all'onorevole Alessandra Locatelli. stucchevole assistere al tentativo di assumersene il merito, come sta facendo qualche esponente dei 5 Stelle. Imparate dai vostri alleati del PD ad adottare la dignità del silenzio e ringraziateci per aver risolto un problema da voi creato. L'articolo 81-*bis*, seppur positivo, è però insufficiente per due ordini di motivi: non pone soluzione, con il mancato effetto retroattivo, alla carenza di copertura nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020; e soprattutto, specificando che l'assenza è equiparata ad un ricovero ospedaliero virtuale, non vi è certezza che questa non incida sul comporto, perché non tutte le tipologie di contratto lo prevedono. È necessario che questo venga specificato nella legge in modo esplicito. La Lega ha presentato, a mia prima firma, un emendamento ed un ordine del giorno che pone soluzione o, in subordine, impegna il Governo ad adottare migliorie, ma purtroppo la vostra scelta di apporre l'ennesima questione di fiducia

voi con la vostra incapacità, con il vostro immobilismo, con la vostra l'inettitudine, restate. Speriamo che il 2021 ci porti la rimozione di entrambi. Signor Presidente, il Covid ci ha messo in una situazione eccezionale, quindi è assurdo ricercare normalità in circostanze come questa e continuare a parlare di inadeguata prassi e di bicameralismo o di parlamentarismo negato, perché non sappiamo come sarebbe andata. Tutte queste chiacchiere sono pertanto Non avremmo accettato, in una condizione di normalità, una situazione così eccezionale. Questa legge di bilancio va quindi licenziata e non strumentalizzata. In questo intervento non parlerò però né dei ristori necessari e dovuti, questi 40 miliardi che vanno a sanare molte situazioni, né degli incentivi che ci potevamo risparmiare,

Parlerò di due emendamenti che non sono passati alla Camera e di uno che invece è stato approvato. Non è passato l'emendamento che posticipa la scadenza dei fondi ai giornali gestiti da cooperative che beneficiano di una quota pubblica, tra cui «il manifesto». È una questione di pluralismo di informazione intesa quale funzione di bene pubblico: mentre cresce una foresta di aiuti pubblici - sacrosanti, lo abbiamo detto in tutti i settori dell'economia, nei confronti de «il manifesto» si è fatto esattamente il contrario. Quindi a che vale parlare di difesa del pluralismo e dell'informazione se le parole vengono contraddette poi nei fatti? Si parla poi continuamente di una riforma del settore, ma si prosegue con tagli in maniera lineare. Sono stati elargiti soldi pubblici per la qualunque, lo dobbiamo dire, anche per l'ottavo centenario del presepe

leggo che sicuramente l'ideologia sull'equivalenza tra informazione e mercato è confermata e questo è un punto molto problematico. non è passato l'emendamento sulla cosiddetta patrimoniale, infelice denominazione. Essa prevedeva un'aliquota progressiva dello 0,2 per cento per la prima fascia da 500.000 ad un milione di euro di patrimonio posseduto, per cento per quelli di oltre 50 milioni di euro. Avrebbe dovuto essere vista come una fiscalità più equa e progressiva, non come un anatema. Come crediamo si debba ripagare il debito prodotto dalla pandemia? L'ultima volta la ricetta è stata chiara: tagli lineari nei servizi pubblici, negli investimenti, nella ricerca e nella salute. Il risultato è che la crisi la paga chi lavora per vivere, dal ceto medio in giù. È dimostrato che la minoranza più ricca della popolazione è diventata ancora più ricca anche in questa pandemia. Questo accade perché si sono fatte scelte politiche ben chiare negli scorsi decenni: deregolamentazione finanziaria, alienazione di patrimoni pubblici, fiscalità di vantaggio per i grandi capitali. per cento più ricco della popolazione detiene il 64 per cento delle ricchezze. Tutto questo nel nostro Paese è aggravato dal regime delle donazioni e delle successioni. Il centrodestra dice che quell'emendamento avrebbe ucciso l'economia di chi produce lavoro, ma non è così. È vero il contrario. L'enorme patrimonializzazione è una delle ragioni della bassa crescita economica. Chi aveva le risorse per investire in ricerca, innovazione e lavoro ha legittimamente preferito accumulare per un semplice motivo: conviene. Non è passato neanche l'ordine del giorno in merito. Quindi io mi chiedo se il Governo vuole ripensare a una fiscalità più equa, progressiva e semmai ecologica. Lo vedremo nella delega. è passato, invece, un emendamento della Lega che prevede che nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le maggiori entrate permanenti rimangano acquisite ai rispettivi bilanci. Un emendamento molto tecnico che è sicuramente un *assist* al principio del residuo fiscale che dispone che le maggiori entrate per gettito fiscale rimangano sul suolo territoriale. Ma la cosa davvero importante è che questo emendamento si iscrive in un quadro di continue incursioni nella definizione di federalismo fiscale prima che vengano definiti i LEP. In questa ottica si configura lo stralcio dell'ex articolo 151 della legge che differiva di un ulteriore biennio - al 2023 - il meccanismo di finanziamento delle Regioni proprio per la mancata definizione dei LEP, che poi è stato reinserito, ma per le forti pressioni, nel decreto-legge ristori-quattro. Visto che il disegno di legge di bilancio se ne occupa, vale la pena anche dire qualcosa sulla ripartizione del *recovery fund*. Nella bozza del piano di ripresa e resilienza che è stato discusso in Consiglio dei ministri, si fa ancora riferimento alla clausola del 34 per cento per il Sud come limite per gli investimenti straordinari decisi dall'Europa e non si tiene conto del fatto che l'Italia ha ottenuto 209 miliardi di risorse da Bruxelles proprio perché il divario del Sud è stato riconosciuto come il più ampio tra i Paesi europei e che il calcolo è stato fatto in base a parametri indiscutibili che sono, sì, la popolazione, ma anche il livello di disoccupazione, le diseguaglianze sociali e il reddito *pro capite*. Un principio non solo europeo, ma che è stato anche ribadito al Parlamento nella relazione della 5a Commissione, recante individuazione delle priorità nell'utilizzo del *recovery fund*, approvata in Aula il 13 ottobre scorso.

Una sperequazione enorme cui va posto rimedio al più presto, e più presto è domani. non nascondo un certo disagio nell'intervenire in questa discussione generale su uno degli atti più importanti, se non il più importante, dell'attività parlamentare: la legge di bilancio, Perché sento questo disagio, che ritengo dovrebbe essere comune a tutti noi membri di questo ramo del Parlamento, e che definirei invece imbarazzo per voi colleghi di maggioranza? Il mio disagio nasce dalla difficoltà di dover apprendere, capire, analizzare e discutere un provvedimento così importante per la Nazione in poco più di qualche ora. Poche ore in cui la Commissione di merito avrebbe dovuto analizzare un provvedimento così complesso e determinante, presentare emendamenti per correggere eventuali criticità emerse in fase di approvazione alla Camera, votare gli emendamenti, venire in Aula ad affrontare una discussione politica più approfondita e, infine, deliberare e permettere a ogni senatore di esprimere un voto consapevole, perlomeno un voto con un minimo di cognizione di causa. Niente di tutto questo. È un metodo che in questa legislatura è ormai diventato prassi: una prassi che non esito a definire il sovversiva, cui il Parlamento viene completamente esautorato e le prerogative di analisi tecnica, giuridica e politica di ogni senatore o parlamentare vengono di fatto annullate. Questo lo dico ai colleghi di maggioranza, in particolare colleghi del PD e di Italia Viva, che ritengo più attenti alle questioni di diritto e che hanno una cultura politica più radicata rispetto a chi oggi siede in maggioranza con loro, ma che non va oltre ai «vaffa», al Palazzo da aprire come una scatoletta di tonno, che pensa ai monopattini o ai banchi con le rotelle, ma che non ha alcun altro obiettivo se non quello di mantenere la poltrona. Ricordo sempre ai colleghi del PD e di Italia Viva quando loro, poco più di un anno fa, occupavano i banchi del Governo con in mano la Costituzione. Forse anche voi siete stati colpiti dalla paura del giudizio degli elettori e vi scordate di tutto pur di rimanere incollati alle vostre poltrone? Eppure, oggi siete voi che fate esattamente quello per cui contestavate l'allora maggioranza. Ciò che mi amareggia ancora di più è il silenzio, un silenzio assordante che proviene dal colle più alto di Roma, che sicuramente osserva la trasformazione del nostro sistema istituzionale, ormai ridotto a un sistema monocamerale di fatto. Mi sarei aspettato una maggiore attenzione e qualche segnale più netto, e non un silenzio - ripeto - così assordante. E lo dico davvero con il massimo rispetto. Tutto ciò non basta a questa maggioranza; anzi, siamo arrivati al punto che, per mantenere un consenso ormai finito, non esita a varare una legge di bilancio piena di mancette, con un'arroganza tale che nemmeno si preoccupa di verificarne le coperture, tant'è che, grazie al lavoro dei colleghi deputati di Fratelli d'Italia, sono stati costretti a rimandare il testo in Commissione. Insomma, un bel pasticcio, che si somma all'episodio di oggi, con il Governo che ammette di aver sbagliato i conti. L'incapacità di questo Esecutivo di gestire la Nazione e soprattutto il tirare a campare pur di mantenere le poltrone è ormai palese. Più di 100 miliardi spesi con i decreti precedenti, con misure poco efficaci non solo per tamponare l'emergenza, ma soprattutto inutili per rilanciare l'economia. Non contenti, vi siete inventati un disegno di legge di bilancio di cui i cittadini, gli enti locali, ma soprattutto le imprese non hanno bisogno; un provvedimento senza visione, senza un progetto, con poco sviluppo, poco di tutto, ma con molto assistenzialismo e molte mancette.

Anche nel disegno di legge di bilancio in esame, nonostante le misure siano abbastanza centrate, le risorse sono limitate ed insufficienti per dare respiro al settore. Penso al comparto del vino, duramente colpito dalla misure anti-Covid

Eppure si stanzia un milione di euro per le associazioni animalistiche, ma neanche un euro per compensare i danni provocati dalla fauna selvatica; non si pensa all'attività venatoria come a un'attività di pubblica utilità per il contenimento della fauna selvatica: penso in particolare agli ungulati, che sono diventati una vera e propria piaga. si ricorda della pesca, per fortuna, con un fondo specifico e 12 milioni per il fermo pesca, ma non c'è una strategia complessiva per il settore e per il rilancio dell'attività, ad esempio con un piano nazionale per il rinnovo delle attrezzature della flotta, ormai vecchia e di fatto improduttiva. Tuttavia, se questo è troppo complicato per il Ministro, almeno sollecitasse la Commissione europea a mettere lo stesso impegno che mette nel difendere gli interessi dei pescatori francesi del Nord nel difendere anche quelli dei pescatori italiani. Allo stesso modo, il Governo dovrebbe difendere non solo gli interessi ma anche il diritto alla pesca dei nostri pescatori. Tuttavia la mancanza di visione purtroppo è generalizzata per tutto il settore agricolo. In questa manovra, se veramente si voleva dare un segnale alle imprese e in particolare al mondo agricolo, si doveva avere il coraggio di eliminare la *sugar tax,* invece ci si limita a procrastinarne l'entrata in vigore e per di più si amplia la platea di coloro che sono soggetti al pagamento, così come per la *plastic tax.* In questo momento di crisi togliere le tasse e non prorogarle sarebbe stato un segnale positivo, che avrebbe creato quell'elemento di fiducia necessario agli imprenditori per pianificare gli investimenti che oggi ritengono inopportuni e rischiosi a causa di queste tasse demagogiche e inutili.

Non so se il Ministro si è reso conto che all'agricoltura sono state destinate poche briciole, forse perché troppo presa nelle trattative per il rimpasto di Governo: solo briciole, all'agricoltura niente. manovra finanziaria sono stati messi in campo quasi 150 miliardi di euro e per l'agricoltura non si arriva a 5 miliardi: 5 miliardi su 150. Il giudizio lo lascio agli agricoltori e ai pescatori. Per questo sarò anche banale e forse ripetitivo: potete cercare la fiducia in quest'Aula

alla vigilia della sua scadenza, con l'aggravante del rischio (purtroppo non tanto lontano visti i problemi emersi) dell'esercizio provvisorio, proprio nel contesto della grave e drammatica crisi che stiamo vivendo. È inaudito: di legge di bilancio pasticciato, che ha bisogno di un decreto-legge correttivo per essere sistemato. Siamo al limite Entro nel merito del provvedimento per lasciare agli atti e per non tacere sulle vostre scelte miopi, anzi cieche, rispetto all'intera manovra, che mai come in questo momento dovrebbe essere determinante per il futuro del nostro Paese. Non siamo solo noi a dirlo, ma anche autorevoli organismi indipendenti, oltre alle associazioni di categoria. Cito, per esempio, l'Ufficio parlamentare di bilancio che nella relazione definisce la manovra - che, ricordo, ammonta a circa 40 miliardi un coacervo di misure indirizzate a diverse finalità condivisibili, ma senza un sottostante disegno di politica di bilancio ben delineato. Dopo una serie di decreti che si sono susseguiti dalla scorsa primavera che non hanno fatto altro che tamponare e male gli effetti sanitari e socio economici della pandemia, ora ci si saremmo aspettati misure strutturali e concrete anche in prospettiva del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. La legge di bilancio poteva e doveva essere la sede utile allo scopo, in coerenza appunto con il piano di rilancio. Si tratta di un ennesimo appuntamento mancato perché a oggi, tra l'altro, il piano non è ancora definito; non vi sono idee chiare e il Governo e la maggioranza continuano a brancolare nel buio litigando. Con questa legge di bilancio siamo ancora di fronte a una pioggia di micro interventi, di *bonus* e incentivi (gli occhiali da vista, le cargo *bike*, i *bonus* per gli *chef*, l'Osservatorio nazionale per la valorizzazione del un milione per una serie di fondi come quello per l'antiusura, per quello sperimentale per la formazione turistica esperienziale, per il fondo per i piccoli musei). Sono tante misure singolarmente plausibili che, però, non incidono effettivamente sui settori ad essi dedicati, che non arriveranno a tutti e che tanto meno incideranno sulla ripresa dell'economia. *(Applausi)*. A oggi non è stato fatto nulla di efficace. Ricordo che le imprese italiane, a fronte di una perdita di fatturato del 13,5 per cento rispetto al 2019 per il Covid, hanno avuto aiuti diretti a sostegno pari solo al 7 per cento del crollo del fatturato dell'intero sistema economico italiano. Questi sono dati della CGIA di Mestre.

a partire dagli sgravi fiscali di rilievo per agevolare le imprese e per chi crea veri posti di lavoro. *(Applausi)*. Le misure presenti nel provvedimento per la decontribuzione per le assunzioni di donne e giovani sono importantissime, ma se sono, come in questo caso, ancora limitate alle nuove assunzioni non incidono sulle migliaia di aziende in difficoltà che, invece, devono ancora ricorrere alla cassa integrazione. Servono misure anche a sostegno di chi mantiene i posti di lavoro, per esempio. La decontribuzione, che risulta interessante per le aziende che non sono in difficoltà, è limitata perché potrebbe avere un impatto maggiore se nel contempo fosse anche abolito il famoso decreto dignità, di dignità ne ha creata davvero poca. *(Applausi)*. Ora più che mai - non è più rinviabile - vi è la necessità di creare maggiore flessibilità nel mondo del lavoro. forse, non avete capito che una volta finiti gli ammortizzatori sociali - prima o poi termineranno - e non potendo più prorogare il blocco dei licenziamenti scoppierà, purtroppo, la bomba e avrà effetti devastanti. sono poi le misure in continuità con quelle già introdotte con i decreti di maggio e di agosto, che prevedono crediti di imposta che riguardano il settore del turismo, dell'editoria, dell'agricoltura e dei trasporti. Anche in questo caso sono poche le risorse per i tanti settori in crisi che comprendono, invece, una filiera articolata e complessa esclusa anche dagli interventi precedenti individuati attraverso i famosi codice Ateco. L'ecobonus al 110 per cento è una formula che potrebbe essere vincente non solo per far ripartire il settore edile, che negli ultimi dieci anni, con la crisi, ha visto perdere oltre 600.000 addetti, ma per l'intero Paese. Il problema sta nella sua complessità assoluta, nella normativa, nella moltitudine di incombenze, certificazioni e asseverazioni costose. È una misura con una serie di pratiche rallentate anche dallo *smart working* nella pubblica amministrazione e che necessiterebbe di una tempistica ben più ampia di quella che è stata concessa. *(Applausi)*. Anche il sostegno alla liquidità delle imprese e i vari fondi - penso a quello creato per l'imprenditoria femminile di soli 20 milioni - costituiscono, come sempre, tanti bellissimi annunci, ma poca sostanza. *(Applausi)*. La riforma fiscale complessiva, tanto annunciata da Conte, è solo annunciata ed evidentemente rinviata a data da destinarsi e il perché è presto detto. È istituito un fondo con dotazione di otto miliardi per il 2022 e di sette miliardi a decorrere dal 2023: una quota di questo fondo non inferiore ai cinque e non superiore ai sei miliardi sarà destinata all'assegno universale e ai servizi per la famiglia. I conti sono presto fatti: gran poco resterà per una vera riforma del fisco, a partire dall'Irpef. *(Applausi)*. O meglio, quella che il Governo chiama riforma fiscale ha al momento sembianze molto diverse dalla riforma fiscale così come intesa e proposta dal centro-destra. Ed è una riforma, quella nostra, che è ormai assolutamente indispensabile e indifferibile per una ripresa del Paese, ma servono risorse. Occorre per questo avere una visione lungimirante e fare scelte politiche non dettate dall'immediato e dal poco, per non scontentare nessuno, ma in vista di un progetto comune per il Paese. Imprenditori, commercianti, partite IVA, autonomi e liberi professionisti hanno bisogno di aiuto. Non basta quello che è stato fatto grazie a proposte concrete di Forza Italia. Confcommercio denuncia proprio in questi giorni che nel 2020 abbasseranno le serrande circa 390.000 imprese del commercio ed è un dato sconcertante. E la prospettiva per i commercianti, prevista da questa legge di bilancio, è un aumento dell'aliquota contributiva per il 2022. Bell'aiuto. Il Governo non vuole proprio distinguere tra incentivi buoni per sostenere il lavoro e sostegni inefficienti a pioggia. Questo Governo e la maggioranza vogliono capire che le migliaia di assunzioni nel pubblico - e non parlo di medici e infermieri, ma di stabilizzazione nella pubblica amministrazione e di assunzioni a livello statale centrale - non risolvono il problema dell'occupazione, ma anzi? Bisogna cambiare filosofia, perché la filosofia assistenzialista, statalista e centralista, con cui ad oggi in questa legislatura sono stati concepiti

e non ne possono più delle vostre ideologie e dei vostri litigi. Vogliono soluzioni e fatti concreti. Signor Presidente, ieri la Confcommercio ci ha consegnato dei dati impietosi sullo stato di salute delle imprese italiane: nel 2020 chiuderanno 390.000 imprese, ne sono state aperte 85.000 e quindi il saldo è altamente negativo; 305.000 imprese non ci saranno più. Rischiano la chiusura 200.000 studi professionali e il tasso di mortalità delle imprese dal 2019 al 2020 si è pressoché raddoppiato, passando dal 6,6 per Ci troviamo qui oggi, in un clima surreale, a discutere del disegno di legge di bilancio che dovrebbe essere la carta d'identità di un Governo. In questo caso lo è, ma è una carta d'identità che che di identità ha ben poco, perché chi la fa da padrone sono la confusione e un modo di mettere insieme tanti cocci in maniera raffazzonata. Francamente non so per la vostra incapacità, che rimettiamo agli italiani di giudicare, ma sicuramente non avete una visione del nostro Paese. *(Applausi)*. È surreale, perché è una manovra di bilancio che arriva qui con un mese di ritardo. È surreale, perché avete segnato un altro *record*:

l'esercizio provvisorio è soltanto perché le forze di opposizione hanno avuto un senso di responsabilità elevatissimo al cospetto della vostra superficialità.

Veniamo qui e scopriamo che il disegno di legge di bilancio non ha copertura finanziaria. Per favore, scendete con i piedi sul pianeta Terra. Avete annunciato per bocca del Vice Ministro

C'è improvvisazione. Vado per *spot*. Era tutto pronto per i vaccini, il supercommissario Arcuri aveva detto che era tutto pronto e alla Camera le forze di maggioranza sono costrette a fare un emendamento che prevede circa 650 milioni di euro per assumere personale sanitario per eseguire i vaccini.

l'anno bianco contributivo per tutti i lavoratori autonomi. Un anno bianco contributivo che guarda ai nuovi non garantiti, che sono coloro i quali pagano le tasse con quello che guadagnano e non con il reddito di cittadinanza. riguarda i numeri, ma guardiamo in positivo anche i valori. Grazie alla Lega, non è passata la legalizzazione della *cannabis.* Vogliamo essere ignoranti, ma vogliamo credere nella vita e non nella cultura della morte.

non ha nulla; questa legge di bilancio per il Sud non ha fatto nulla ed, anzi, ha tolto due miliardi di euro sulla decontribuzione delle imprese al Sud, al Sud, stanziando però qualcosa per le scuole innovative: 300.000 euro. È una vergogna. Non c'è un disegno per il Sud, non avete il coraggio di guardare un Sud diverso, che rappresenta la porta dell'Italia sul Mediterraneo. Voi siete meridionali, come gli stessi meridionalisti che hanno inguaiato il Mezzogiorno; quando arrivavano fior fior di quattrini tramite la Cassa per il Mezzogiorno, tramite l'obiettivo uno. Se non c'è una progettualità

noi siamo tutti vaccinati nei confronti di questo cattivo modo di far politica. Accettiamo tutto, accettiamo che non si discuta, accettiamo anche che si parli di water e di bidet, invece che di crescita, di sviluppo e di soluzioni dei problemi. però rispetto non nei nostri confronti, ma nei confronti degli italiani, risparmiandoci almeno il teatrino che hanno messo su Renzi e Conte, con la comparsa di Zingaretti.

che la gestione degli interventi di tutela e conservazione del bene pubblico è contrassegnata da tempo da una logica emergenziale e non da un circuito virtuoso frutto di una programmazione pluriennale. Credo sia importante prendere atto dell'esito dell'indagine della Corte dei conti, perché noi oggi stiamo parlando di programmazione. Grazie a questo Governo

Quando parliamo di tutela, parliamo anche di rilancio e di valorizzazione delle professioni che lavorano per la tutela del nostro enorme e preziosissimo patrimonio culturale. Quando parliamo di valorizzare le professioni e toglierle dai circuiti del precariato, parliamo di rilancio del lavoro e di implementazione del bacino di lavoro e di orizzonti per i molti studenti che si dedicano a questo tipo di studi. Quando parliamo di tutela e di aumentare gli investimenti - purtroppo, dobbiamo prendere atto che siamo ancora fermi al palo dello 0,9 parliamo di tutelare quella fonte intangibile di ricchezza quotidiana che ci permette uno sviluppo armonico, come persone e comunità.

e anche verso la comunità globale che, attraverso l'organismo dell'UNESCO, ha riconosciuto molta della nostra ricchezza come patrimonio dell'umanità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che stiamo per lasciarci alle spalle è un anno complesso, che non dimenticheranno le tante famiglie che hanno dovuto subire perdite inaspettate, inaspettate, né i nostri giovani a cui è stato sottratto un tempo irripetibile. Ne siamo pienamente consapevoli noi che, con il nostro impegno, abitiamo questi luoghi e sentiamo il peso di scelte importanti in questo momento drammatico per il nostro Paese. La pandemia ha innescato una crisi sanitaria senza precedenti, che si è ovviamente ripercossa sull'economia, creando un'emergenza sociale che ha coinvolto milioni di persone. Questo periodo di straordinaria incertezza ha fatto anche emergere alcune debolezze del nostro attuale modello di sviluppo e ha portato a ripensare il sistema con una più evidente direttrice di cambio del Paese, a partire dalle disuguaglianze, dalle iniquità tra persone e territori, fino alla piena coscienza di un'idea del vivere e del produrre sempre più compatibile con l'equilibrio ecologico. L'Italia, insieme all'Unione europea, ha dimostrato in questi mesi difficili di saper rispondere con orgoglio e visione alla sfida tremenda che si è presentata. Oggi, però, siamo chiamati a una responsabilità più grande, una responsabilità collettiva e condivisa, quella di guidare una fase nuova, avviare la ricostruzione, realizzare le condizioni per un'economia più giusta, una società più equa, un'idea di sviluppo sostenibile e resiliente, dando agli italiani punti fermi. È questo il punto politico e questa legge di bilancio rappresenta un passo importante in un nuovo percorso, in vista di un equilibrio diverso, declinato al rispetto dei diritti dell'individuo, della collettività e dell'ambiente, nell'ottica di quella transizione non solo economica, ma anche umana, valoriale; un'economia del bene comune, un'economia non autosufficiente e autonoma, ma una disciplina sociale e che guarda alla transizione ecologica anche come opportunità per creare lavoro. Sono tanti gli interventi presenti nella manovra che si rivolgono a questa visione e che incardinano la transizione verde del nostro Paese, considerando appunto la sostenibilità come condizione indispensabile per garantire crescita e benessere. Viene prorogato a tutto il 2022 uno strumento di eccezionale importanza, il superbonus, un enorme incentivo all'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare nazionale che, grazie a questa legge di bilancio, potrà essere applicato a nuovi interventi. interventi. Fondamentale, tra questi, è l'eliminazione - per esempio - delle barriere architettoniche. E, sempre in tema di rigenerazione energetica e urbana, è da segnalare il rifinanziamento di tutte le misure di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio che, insieme alla proroga del *bonus* verde e degli incentivi per gli interventi di restauro, potranno dare una grande accelerazione all'opera di rinnovamento dei nostri borghi, delle nostre periferie e delle nostre città. A questi si aggiungono due misure di grande significato: le nuove risorse destinate al programma sperimentale di riforestazione urbana, previsto già dal decreto clima, per incoraggiare la creazione di foreste urbane e periurbane, e l'istituzione della fondazione per il futuro delle città, che si occuperà di alimentare l'idea di uno sviluppo del sistema produttivo nazionale coerente con la transizione verde dell'Italia. In questo passaggio verso un'economia più pulita, dobbiamo coinvolgere l'industria e le istituzioni con un corposo piano di investimenti. segnalare due imprescindibili elementi nella nuova legge di bilancio: i nuovi fondi dedicati agli interventi di decarbonizzazione e di efficientamento del settore industriale, che aiuteranno quella svolta tanto attesa sotto il profilo della produzione di emissioni inquinanti, e poi l'incremento delle risorse in favore degli enti locali, che serviranno alla progettazione e alla realizzazione delle opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio per gli interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico mirati a ridurre l'inquinamento ambientale nella rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso le fonti rinnovabili. È ovvio che la legge di bilancio prevede tante importanti misure. Abbiamo ancora davanti a noi un tempo complesso, ma dobbiamo avere piedi saldi e testa lunga. Una manovra economico-finanziaria è un atto di intelligenza che legge dentro i bisogni profondi del Paese; sceglie in nome di un rigore direi più che numerico culturale, intervenendo nelle difficoltà e trasformandole in occasioni di crescita. Abbiamo rappresentato in questo modo le precondizioni di azioni che, con coraggio e responsabilità, guardano al futuro lavorando per la stabilità del presente. Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il Senato è costretto a ratificare la manovra blindata senza possibilità di modifiche. Altro che rammarico, presidente Pesco: questo è grave, è un'umiliazione per noi senatori. A parti inverse, è accaduto lo scorso anno. Chi non ha toccato palla allora è stato Montecitorio; due anni consecutivi con lo stesso problema, che non è il Covid-19: il problema è il traballante Governo Conte! Siete voi! D'altronde, l'Esecutivo, vittima di faide nella maggioranza, ha presentato al Parlamento la manovra da 40 miliardi con un mese di ritardo, comprimendo i lavori a Montecitorio e facendo rischiare l'esercizio provvisorio; una manovra consegnata pessima al Parlamento, con oltre 30 articoli fatti fuori subito, stralciati dalla Commissione bilancio. Ne ricordo due, sciagurati. Il primo sull'istituzione della fondazione sulla *cybersecurity*: una norma sbagliata nel metodo e pessima nel merito, vista la inopportunità di affidare a privati la sicurezza dei dati. è sulla cancellazione della regionalizzazione delle concessioni idroelettriche: l'ennesimo maldestro tentativo, fallito, di centralizzazione voluto dal Partito Democratico; un regalo ai concessionari e un grave danno erariale di circa 10 miliardi per gli enti territoriali. una manovra che, dopo i lavori alla Camera, è stata infarcita di tanti micro *bonus*, veri sperperi di denaro, come i 20 milioni per il *bonus* idrico per sostituire rubinetti e *bidet*, che sicuramente saranno bruciati con la *roulette* del *click day*; day*; i rinnovati e troppi incentivi per l'acquisto di auto elettriche: una tara, quella vostra, dell'elettrificazione della mobilità. È una manovra nata senza progettualità, ma comunque migliorata dal centrodestra e dalla Lega, che ha raccolto diversi risultati. Grazie alla determinazione dell'onorevole Garavaglia, si è ottenuto che, agli 800 milioni a disposizione del Parlamento, si aggiungessero anche 3,8 miliardi previsti dal "fondone" Conte, che il *Premier* con più decreti voleva spartire. Così, con un miliardo, abbiamo garantito l'anno bianco contributivo per autonomi e professionisti con calo di fatturato. Sono stati poi stanziati 224 milioni per rifinanziare il contratto di espansione per le imprese sopra i 250 dipendenti, introdotto con la Lega al Governo. Altra grandissima soddisfazione è lo *stop* all'emendamento grillino sulla *cannabis light*. La droga, colleghi, fa male e deve essere contrastata, non legalizzata! *(Applausi)*. La manovra è stata un'occasione persa per cancellare o prorogare la *plastic tax.* È incredibile come, dopo gli usi insostituibili cui si è ricorso con i dispositivi in plastica in emergenza Covid-19, voi insistiate nel penalizzarla, bastonando così il comparto produttivo italiano. Sul superbonus, poi, si è intervenuti ancora con la norma introdotta con il decreto rilancio, con il famoso articolo 119: la quarta volta in sette mesi. Sono state, però, deluse le aspettative di imprese e tecnici che chiedevano una proroga più ampia.

Ma, dopo una settimana di tira e molla, avete dovuto abbozzare, rinunciare ai ventiquattro mesi e accontentarvi di un 6+6: ne è uscita una proroghina di sei mesi al 30 giugno 2022 più altri sei mesi, ma solo per i condomini se, a quella data, si realizzerà il 60 per cento dei lavori. Quindi, è tutt'altro che una proroga piena al 2022; anche perché, i secondi sei mesi non sono stati concessi agli edifici unifamiliari, alle villette a schiera e alle altre categorie di beneficiari. Sul superbonus una cosa ormai è chiara, vedendo le modifiche apportate e anche leggendo la bozza del PNRR: l'ampliamento della platea dei beneficiari non si farà, né ora e né mai. Addio, dunque, al 110 per cento per capannoni e laboratori industriali; nulla ci sarà per strutture alberghiere e nulla per le scuole paritarie. Cari colleghi, si sta palesando il limite di questa misura che, annunciata in pompa magna, fino ad oggi ha ottenuto un solo risultato, ma in negativo: ha rallentato gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Oltre al ginepraio tra norme primarie, decreti ministeriali e circolari dell'Agenzia delle entrate, permangono dubbi interpretativi. Tanti sono i rischi per beneficiari e tecnici che, più conoscono la misura, più la evitano, consapevoli che il superbonus, da grande opportunità, rischia di trasformarsi in una trappola pericolosa. E poi vi è l'eccessivo costo della misura, insostenibile per le casse dello Stato; se si valutasse il rapporto costi-benefici, scopriremmo delle sorprese. Insomma, la misura si è già instradata su un binario morto e non avrà futuro. Mi avvio alle conclusioni, colleghi, per ricordarvi che, accanto al dramma sanitario, cresce vistosamente la piaga della povertà e del disastro economico-sociale, che non può essere affrontata con derive assistenziali, con l'immorale reddito di cittadinanza oppure bloccando i licenziamenti e gli sfratti, peraltro senza dare alcun risarcimento ai proprietari. Bloccate invece, e subito, le 30 milioni di cartelle esattoriali pronte a partire dal 1° gennaio, che creeranno una carneficina tra le imprese e uno scontro sociale senza precedenti. Siamo nel pieno di una pandemia sociale e voi della maggioranza dovreste avere la responsabilità di operare scelte oculate, come il taglio delle tasse e investimenti capaci di creare sviluppo e occupazione, di operare scelte irresponsabili come quelle che state assumendo, sprecando le risorse del maggior debito pubblico autorizzato o quelle del *recovery plan*, che - lo ricordo - sono prestiti che le prossime generazioni dovranno restituire. Mossi da un cieco ambientalismo e noncuranti dell'impatto negativo sulle nostre imprese, sostenete il nuovo taglio della CO2 deciso dalla UE, sprecando risorse, senza il principio della neutralità tecnologica, in investimenti che rischiano paradossalmente di fare danni all'ambiente senza una sostenibilità economica e sociale. Finanziate l'auto elettrica e i monopattini cinesi, senza valutare l'impatto dell'impronta di carbonio che questo crea. Puntate al 100 per cento delle rinnovabili, del fatto che non sono programmabili e dunque, per garantire la sicurezza del sistema energetico, dovremo ricorrere a sistemi di *backup* costosi, che impattano sulle bollette, oppure a inefficienti processi di produzione di elettricità dall'idrogeno, magari quello verde costosissimo, l'unico che vorreste sostenere. Anziché lo sviluppo del Paese, all'insegna di un delirio ambientalista senza limiti, state tentando - e lo si è visto nella bozza del proroga termini - di dare il colpo mortale al comparto del gas del nostro Paese, compresa la Val d'Agri e Tempa Rossa in Basilicata, portando ancora più in miseria l'Italia, condannandola a dipendere energeticamente per il 100 per cento Sulla gestione dei rifiuti, caratterizzata nel Centro-Sud da una carenza di impianti, avete scritto nella bozza del PNRR di voler investire solo in nuovi impianti TMB, che sono l'emblema del fallimento della gestione della *monnezza* di Roma e del Lazio: è una follia. Signori della maggioranza, del fatto che state sorreggendo un Governo fragilissimo e senza visione per il Paese, inadatto ad affrontare una crisi, forse la più pesante anche tra quelle accadute nel XX secolo. Sulla bozza del PNRR Italia Viva afferma che arraffazzonate senz'anima; il *recovery plan* non può essere il terreno di scontro sulle spalle degli italiani. Siete spaccati sulla cabina di regia. Siete spaccati sui progetti, che - lo ricordo devono essere cantierabili. Siete spaccati sulla TAV. Per cortesia, fate un gesto di umiltà, per il bene del Paese: date le dimissioni e andate a casa.

citarne solamente due, chiedendo poi al Governo magari di dare a questi seguito con dei provvedimenti propri. Fratelli d'Italia ha presentato, con un emendamento a mia firma, la richiesta di aumentare il fondo destinato all'acquisto e alla diffusione dei vaccini anti-Covid, al fine di poterli destinare anche agli italiani residenti all'estero, che si trovano in Paesi dove non sarà possibile una diffusione capillare degli stessi vaccini.

garantire la vaccinazione alle nostre comunità italiane all'estero, lì dove avessero difficoltà a fare ciò. Chiedo al Governo di non cestinare questa proposta di Fratelli d'Italia, di farla propria, magari con un decreto-legge, in modo da poterla rendere immediatamente operativa e non dimenticare gli italiani che vivono all'estero.

propone l'eliminazione del minimo contributivo INPS per artigiani e commercianti. Mi rendo conto che è un argomento non semplice per chi

si prevede che gli artigiani e i commercianti, a prescindere dal reddito effettivo fatturato nell'anno, debbano versare almeno

Quindi, la partita IVA iscritta alla gestione separata non ha un minimo contributivo: se si fattura zero, si paga zero; se si fattura poco, si paga poco. All'INPS c'è invece la

Lo abbiamo chiesto in generale, ma almeno lo si faccia in questa fase drammatica, nella quale i nostri artigiani e i nostri commercianti sono in ginocchio. Qualcuno potrebbe obiettare che il minimo contributivo serve per evitare un'eccessiva facilitazione nell'accesso alla pensione, ma non è così, perché questo poteva valere nel sistema retributivo. a seconda di quanto si versa, aumenta o meno il montante contributivo che determina l'entità della pensione. Per quanto riguarda il diritto alla pensione, e cioè gli anni di anzianità, è già prevista nella cassa

di calcolo, pari a 15.500 euro all'anno di reddito, che assicura un anno pieno di contribuzione. Se si dichiara di meno, si pagherà di meno, ma si avrà meno di un anno di anzianità. Quindi, non stiamo regalando niente a nessuno,

Mi è venuto anche il sospetto che sia un'ostilità voluta nei confronti di artigiani e commercianti, visto che vengono dipinti sistematicamente come ladri, evasori, truffatori, persone che prima chiudono e meglio è. E allora

ridotto alla versione *discount*, ossia la versione scamuffa nella quale, tra le varie assurdità che adesso non ho il tempo di elencare, sono stati esclusi artigiani e commercianti. Quindi, nell'accesso a nuove forme di ammortizzatori sociali per le partite IVA,

Si tiene il minimo contributivo - non gli è stato tolto - e non gli viene dato neanche l'ammortizzatore sociale; le imprese continuano a rimanere in ginocchio e così

sono dei nemici da colpire. Questo non è ciò che pensiamo noi e, quindi, Fratelli d'Italia continuerà a battersi in ogni sede per difendere gli artigiani, i commercianti e il popolo delle partite IVA, sistematicamente colpiti da questo Governo.

rappresentanti del Governo, colleghi senatori, prima di parlare della manovra economica e finanziaria consentitemi alcune considerazioni procedurali e di tempistica che, in un sistema come il nostro, quello del bicameralismo perfetto sono non meri dettagli ma sostanza di scelte istituzionali che tanti anni fa sono state fatte dai nostri Padri costituenti.

31 dicembre, fatidica data per non andare in esercizio provvisorio. *(Applausi)*. Ci ritroviamo quindi in una strada tortuosa, in un percorso difficile. il Senato oggi ratifica un provvedimento che è stato approvato soltanto dall'altro ramo del Parlamento. Se non mi sono perso qualcosa in quest'Aula parlamentare, ritengo che una riforma costituzionale che superi il bicameralismo perfetto non sia stata ancora approvata nel nostro Parlamento. sta accadendo che le prerogative costituzionali del Senato oggi siano così compresse da evitare assolutamente il confronto politico su un atto fondamentale, perché ricordiamo che la manovra finanziaria è l'atto politico per eccellenza eccellenza del Governo. A tal proposito, mi torna in mente un episodio accaduto sempre qui quasi due anni fa, di cui fu protagonista il Gruppo parlamentare del Partito Democratico: allora, proprio sui tempi ristretti della manovra economica, sollevò un conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale. Purtroppo all'epoca il Partito Democratico era partito di opposizione e quindi si opponeva ai metodi di compressione del dibattito parlamentare. Invece questa volta è partito di Governo e ne fa pertanto un *modus operandi*. *(Applausi)*. Complimenti alla coerenza del Partito Democratico. Assistiamo - come dicevamo - a un monocameralismo alternato e anche in questo caso è giusto ricordare ai paladini

Fatte queste premesse, arriviamo a esaminare la manovra di bilancio in alcuni suoi aspetti importanti e fondamentali. La manovra al nostro esame vale 37,9 miliardi nel 2021, di cui 24,6 in *deficit*.

investimenti per riforme strutturali, aiuti diretti alle imprese, ai professionisti, agli artigiani, al commercio e alle partite IVA. Abbiamo anche chiesto meno burocrazia e, quindi, un piano burocrazia

trasporti e mobilità, che in questo momento sono fondamentali anche per il distanziamento sociale e per la limitazione del contagio, soltanto 300 milioni di euro, di cui 100 vanno a rinnovare il bonus mobilità.

vivendo. Ancora una volta, infatti, tale manovra è un atto che rincorre a fatica l'emergenza, non disegna una strategia per il futuro, per la ripartenza del nostro Paese. Ancora una volta assistiamo a un provvedimento che fonda i suoi pilastri su alcune questioni che qualche gruppo politico ritiene essenziali - pilastri che sono nuovamente il sussidio, l'assistenza le stabilizzazioni pubbliche - e non getta assolutamente le basi per una ripresa economica fondata sugli investimenti, sull'iniziativa e sul sostegno all'iniziativa economica privata e soprattutto su ciò di cui il Paese ha bisogno, e cioè una riforma fiscale. Per la ripartenza, sappiamo benissimo che a partire dalla metà del prossimo anno, il 2021, saranno a disposizione le cospicue risorse economiche che arriveranno dal programma Next generation EU, sul quale finora in Parlamento è mancato un vero e proprio confronto. Il Parlamento deve contribuire all'indirizzo e al controllo di questi progetti che devono essere condivisi con le opposizioni, con le parti sociali e con i corpi intermedi, perché i soldi che arriveranno ci sono e sono tanti, ma dobbiamo ricordare che una gran parte di essi è a debito e inciderà sui nostri cittadini, sulla popolazione, sulle future generazioni. *(Applausi)*. Quindi, noi dobbiamo essere parte integrante, oggi, del dibattito dibattito su quei fondi. La Confcommercio, in queste ore - l'abbiamo detto in molti in quest'Aula - ha dichiarato morte 390.000 imprese in Italia, per cui dobbiamo assolutamente utilizzare

Anche se alcune proposte di Forza Italia sono state prese in considerazione, noi diciamo ancora una volta sì agli italiani, ma diciamo no, ancora una volta, a questo Governo perché assolutamente non ne condividiamo né le premesse, né tantomeno i metodi di svolgimento dell'azione politica.

erano girate le bozze colorate, senza alcun valore, peraltro. Erano 229 articoli, già con una connotazione di polverizzazione degli interventi. Dopo qualche giorno, il Presidente della Commissione bilancio alla Camera aveva stralciato - già allora - una trentina di misure che con il bilancio non c'entravano nulla o perché ordinamentali o, peggio, perché particolaristiche e localistiche. Senza pudore, alcuni di quegli articoli erano riusciti a rientrare dalla finestra nel decreto-legge ristori. Ma ormai siamo abituati a piroette Questo mette in evidenza che l'azione dell'attuale Governo è confusa, con una parcellizzazione dei provvedimenti e senza una visione, e non mi stancherò mai di dirvelo. Questo modo di agire è dannoso per il Paese. Vi rendete conto? Siete arrivati al 27 dicembre a votare in prima lettura la legge di bilancio alla Camera, passata in fretta e furia al Senato. Non abbiamo avuto il tempo materiale di esaminarla, sommariamente, salvo comunque accorgerci che, probabilmente, proprio per la fretta, la legge di bilancio è viziata da errori di copertura su un singolo provvedimento e deve già essere corretta. Ciò dà la misura dell'inadeguatezza di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene. Sì, perché la maggioranza ha avuto bisogno della collaborazione delle minoranze, e non certo perché la manovra ci piaccia: semplicemente abbiamo voluto evitare di trascinare il nostro Paese all'esercizio provvisorio. L'Italia e gli italiani non se lo meritano, soprattutto in un momento di così grave crisi. E l'inadeguatezza dell'Esecutivo si vede dall'inizio della crisi, dalle tante contraddizioni. Questo è il Governo dei *bonus*, il Governo dei crediti di imposta. Ma non è più facile non far pagare alle attività in crisi tasse, contributi e tutto ciò che che vizia l'attività produttiva del nostro Paese? Persino l'assegno unico per le famiglie poteva essere un aiuto: l'avete trasformato in un'elemosina alle famiglie, con risorse insufficienti tanto che il Presidente dell'Istat ha confermato in audizione che, con questa misura, una famiglia su tre prenderà meno di quanto prende oggi con gli assegni familiari.

riconoscere che la Lega, in Commissione bilancio alla Camera, ha fatto un ottimo lavoro.

si è ascoltata la Lega e quelle risorse sono state destinate all'iniziativa parlamentare. Quindi, Lega e minoranza sono riuscite a realizzare migliorie, soprattutto a favore di autonomi e partite IVA. IVA. D'altronde, le partite IVA e gli autonomi sono quelli che, obiettivamente, in questo momento stanno soffrendo di più e sono i più fragili. Parlo, quindi, dell'anno bianco contributivo per autonomi e professionisti con fatturato inferiore ai 50.000 euro nel 2019 e che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 33 per cento (era un emendamento dell'onorevole Garavaglia).

Questi sono soltanto degli esempi che hanno tentato di portare un po' di buon senso in questa manovra, ma l'impianto rimane alquanto deludente, privo di un minimo di programmazione e disorganico, fatto di fretta. Non raccontateci poi la storia dell'emergenza Covid, perché il tempo per distruggere i decreti-legge sicurezza lo avete trovato in piena emergenza economica, quando si sarebbe dovuto pensare esclusivamente alla sessione di bilancio.

evidentemente abbiamo perso l'abitudine, perché l'anno scorso, se vi ricordate, non c'era il Covid, ma eravate in ritardo lo stesso: c'è stata un'unica lettura con fase emendativa in Senato.

abbiamo quindi segnalato gli errori di cui ho già parlato, che avrebbero dovuto essere corretti proprio in Senato, ma manca il tempo. Non ci è stato permesso di farlo. Questo Governo è inadeguato e in particolare lo è il ministro dell'economia Gualtieri, primo responsabile di questo scempio, che non si vede mai in Aula ed è pronto a promuovere, a breve, un ulteriore scostamento di

voce per voce, su come avete privilegiato una visione miope, assolutamente piena di marchette e invece priva di un piano di sviluppo che è necessario, specie in una situazione drammatica come quella attuale. C'è un punto però che desidero riprendere ed è quello che riguarda il Piano nazionale vaccini, o più in generale la questione dei vaccini. Avete visto tutti in televisione, a reti unificate, il grande evento: sono arrivate arrivate 9.750 dosi di vaccino. Ce l'hanno fatta! Sono meno di 10.000 dosi. Pensate che la Danimarca, che ha sei milioni di abitanti, poco più della Sicilia, ne ha avute 40.000. Però, noi ci affidiamo all'Unione europea

si blocca il piano vaccini. Figuriamoci che succederà quando dovremo farlo a 40 milioni di italiani! Non è questo il punto, comunque. Mentre noi ci atteniamo rigorosamente alle regole europee, la signora Merkel - che fa bene per il suo Paese

vogliono vaccinarsi. *(Applausi)*. Siamo in una fase veramente di scollamento totale e poi si chiede all'opposizione di fare propaganda. Faremo propaganda perché tutti si vaccinino, però ho consigliato alla Meloni di farlo separando la sua faccia da quella degli altri perché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. *(Applausi)*. È troppo comodo volere le nostre facce, il nostro aiuto quando si decide tutto da soli, come con questa finanziaria. Presidente, colleghi, vorremmo sapere se c'è già questo piano di vaccinazione.

si dice che saranno date le direttive di riferimento per i piani che ogni singola Regione svilupperà. Qualcuno di voi ci sa dare un numero di telefono a cui possiamo chiedere dov'è questo Piano nazionale dei vaccini? Qualcuno di voi ci può indicare un nome e un cognome, a fronte dell'affermazione «daremo il vaccino a tutti *gratis*»? Dov'è la persona, l'ente, il gruppo,

di questo non abbiamo notizie. Se ce l'avete, fatecelo sapere; siamo in attesa. Nella finanziaria, però, abbiamo scoperto tante piccole

i monopattini rimangono, come si può vedere, per esempio, a Milano in questi giorni, il mezzo di trasporto privilegiato, magari chiudendo corso Buenos Aires e facendo in modo che ci sia una coda infinita

con questa e con tutte le altre non poche marchette (perché si chiamano così) che avete fatto. Ve ne potrei leggere

il reddito di cittadinanza. Ma perché non prorogarlo fino a quando non sarete più al Governo? Per altri nove anni o non so per quanti anni l'avete prorogato. Tanto a che serve? Basta scrivere: 4 miliardi per il reddito di cittadinanza.

se continuare a stare insieme. E per stare insieme devono spartirsi meglio il bottino. Ebbene sì, il bottino, perché non mi direte è diverso l'argomento di cui discutete. Sapete come risponde il Partito Democratico? Vi dice di stare attenti, perché se cade questo Governo si va a votare e non è un richiamo alla democrazia, ma una minaccia a coloro che, pur di non andare a votare, sono pronti a dire di sì a qualunque proposta. Un atto di democrazia diventa un atto di minaccia. Ormai, se volete minacciare qualche parlamentare della maggioranza, di tutti i partiti di maggioranza, e fargli chinare la testa, è facilissimo. Basta dirgli: o voti così, oppure noi facciamo votare gli italiani. Povera democrazia italiana, povera Italia!

è l'incredibile storia di un emendamento osteggiato e torturato da lungo tempo, quello richiesto dalla sentenza della Cassazione per sistemare al meglio la legge 2 dicembre 2016, n. 242, in vigore dal 2017, che riguarda la filiera della canapa industriale. Ora non voglio parlare di droga, ma chiarire semplicemente un punto, onde evitare di fermarci a discutere su questo. In qualsiasi libro di botanica scoprirete che la cannabis è un'unica pianta con diverse varianti, alcune delle quali con effetti "droganti", come hanno definito con un italiano un po' forzato i giudici della Corte di cassazione, e che possiedono effetti stupefacenti; le altre tipologie senza effetti droganti, quindi senza effetti stupefacenti o psicotropi, sono meglio conosciute da noi da tantissimo tempo come canapa,

essendo stato bocciato questo emendamento, aggiungete al novero anche queste 3.000 imprese) dà lavoro a 12.000 famiglie e porta all'erario circa un miliardo: non da poco. Non si produce droga, ma usando la canapa da secoli (marcite e campi si estendevano da Nord a Sud), abbiamo imparato a ottenere dalla sua corteccia corde, filati, vestiti, fibre plastiche non inquinanti, combustibile, concimi naturali e carta, carta, senza abbattere foreste. Dal fusto, opportunamente trattato, abbiamo ottenuto materiale edilizio, pannelli isolanti per rendere le case più sane e con maggiore risparmio energetico; la famosa *green economy* - pensate - anticipata e promossa anche durante il Ventennio fascista. Quindi, appurato che non voglio parlare di droga, ma voglio parlare di canapa, la vicenda di questo emendamento reietto è il punto centrale. inizio, la prima volta, quando viene ritenuto inammissibile in quest'Aula nel dicembre dello scorso anno. L'ignoranza sull'argomento è tale che ci viene detto «fate una legge»; peccato che la legge c'è e l'emendamento è appunto alla legge che c'è già. il 16 ottobre 2020 avviene un fatto gravissimo, che va sottolineato; un dirigente dell'ufficio centrale stupefacenti, di cui conosco anche il nome, ma stendiamo un velo pietoso, violando l'*iter* che ogni norma segue, in maniera inaccettabile - e questo è provato - bypassando cioè il vaglio dei Ministri coinvolti, faceva arrivare sulla scrivania del ministro Speranza un fogliettino, un "decretino" in cui si metteva si metteva la canapa nella tabella relativa alle sostanze stupefacenti. Una bomba *contra legem* che avrebbe di colpo trasformato l'intero comparto produttivo in un comparto criminale. Quindi, dovremmo chiederci se oltre al Governo c'è qualcun altro che legifera, magari quelli messi in certe agenzie da precedenti Governi. La notizia esplode mandando tutti nel panico e si sospende il decreto. Si crea un tavolo di lavoro, che ancora deve dare i suoi frutti. L'operazione è importante, soprattutto scoperta la malafede della dirigente ministeriale del farmaco (AIFA), la quale, durante un incontro istituzionale, alla richiesta di ottenere l'elenco dei loro studi in possesso e la bibliografia scientifica relativa alla *cannabis*, ha risposto solo con farfugliati balbettii. L'ultimo atto di questa tragica vicenda è l'emendamento 168.03 che approda in Commissione bilancio alla Camera con parere negativo del Ministro della Salute. Incredibile. Sileri e i promotori dell'emendamento provano a dare le controdeduzioni, ma nulla, il Ministero tace; è incomprensibile. perché questa ostinazione a non regolamentare adeguatamente con un micro sforzo un settore che potrebbe crescere in modo esponenziale, recuperando terreni, agricoltura, imprese, commercio e un volume d'affari e di impiego enorme. Non so quale sia la risposta. Forse perché metterebbe in crisi multinazionali, magnati petroliferi, la produzione della plastica e la *plastic tax*, i derivati velenosi da idrocarburi.

due battute che ho ricevuto in questa Aula, gridate dalle opposizioni. Quando dissi che avevo ancora le tovaglie della mia bisnonna filate a canapa, ricevetti un urlo dai banchi dell'opposizione: «fumatele!».

risposta fu «Sì, ma la coltivano solo i drogati». Evidentemente a qualcuno in questo Parlamento, oltre alla canapa, non interessa neanche la cultura. Voglio solo rivolgere un ringraziamento dovuto per lo sforzo compiuto per cercare di risolvere questo problema annoso ai deputati Sodano, Sarli, al granitico Matteo Mantero, al Senato e a tutti i colleghi

Signor Presidente, siamo consapevoli che questo disegno di legge rappresenti una manovra finanziaria quasi *in tempore belli*, in tempo di guerra, visto il difficilissimo contesto pandemico che stiamo vivendo. In questo senso anche il nostro Gruppo sa bene che, nonostante consideriamo estremamente negativo il fatto di non poter fare alcuna modifica al testo della Camera, lo spettro di un esercizio provvisorio dello Stato durante questa crisi, ci pone di fronte ad una scelta di responsabilità verso il Paese. In riferimento alle necessità delle nostre comunità alpine, in particolare della Valle d'Aosta, che rappresento, avrei voluto porre temi per migliorare questa manovra finanziaria. ad esempio, alla valorizzazione del settore idroelettrico e, in particolare, della Compagnia valdostana delle acque (CVA), proponendo l'esclusione di quest'ultima dall'applicazione della cosiddetta legge Madia, per permettere una manovrabilità sul mercato. alla disapplicazione della stessa legge Madia agli impianti a fune a partecipazione pubblica, per salvarne le sorti in questa grave crisi, al potenziamento della nostra rete ferroviaria e alla proposta di rivalutare l'ambizioso progetto della Torino-Aosta-Martigny-Losanna, che darebbe un respiro internazionale all'intero Paese e la possibilità di una reale modernizzazione del nostro asse ferroviario. soluzione delle criticità rispetto alla manutenzione dei *tunnel* del Gran San Bernardo e del Monte Bianco; al miglioramento del funzionamento in agricoltura dell'Agea rispetto ai pagamenti a favore delle nostre aziende agricole; agli interventi per sollevare il commercio, il turismo, l'artigianato e le partite IVA da obblighi fiscali in questo difficile momento; a misure a sostegno della scuola, dell'università e della sanità. Inoltre, il mio auspicio che lo sconto previsto per le Ragioni a Statuto speciale (per la Valle D'Aosta 3,2 milioni di euro nel 2021) sulla compartecipazione al risanamento dello Stato sia rivisto in aumento durante l'anno. che nel 2020 fu di 84 milioni. Al riguardo, ringrazio il vice ministro Misiani che ha lavorato in questo senso. Vorrei sottolineare quanto mi abbia fatto male sentire nelle settimane scorse autorevoli politici e testate giornalistiche nazionali considerare il mondo dello sport invernale come semplice divertimento, o - peggio ancora - venire rimproverati di non pensare abbastanza ai nostri morti e ammalati. Sono indignato. Noi valdostani siamo un esempio di come ci si prende carico dei nostri anziani e delle persone non autosufficienti. Tutto il settore del turismo invernale rappresenta uno dei pilastri della nostra economia e il sostentamento per migliaia di famiglie. Il ritardo di un mese, ahimè, con il quale il Comitato tecnico scientifico ha risposto alla bozza di protocollo sanitario delle Regioni sulla ripresa degli sport invernali dimostra un'ulteriore mancanza di rispetto. signor Presidente, come senatore della Valle D'Aosta e rappresentante dell'alta montagna, sono a sollecitare più collaborazione e lealtà; quella lealtà che la Valle d'Aosta ha avuto in questi anni, garantendo allo Stato un contributo per il risanamento della finanza pubblica ben più alto (dovuto all'applicazione del metodo Siope, che abbiamo sempre contestato) rispetto alle nostre possibilità economiche. nostre possibilità economiche. In questo periodo, in cui bisogna muoversi con difficile equilibrio tra la tutela della salute e il diritto al lavoro, da gente di montagna con passo lento e costante andiamo comunque avanti con dignità, come abbiamo sempre fatto nei secoli,

di legge di bilancio in esame è ricco di misure che prestano attenzione all'ambiente, a partire dal rafforzamento del superbonus per le riqualificazioni energetiche degli immobili. Non cito le diverse misure che sono state rinnovate o introdotte, ma mi soffermo sull'istituzione del Fondo per il risparmio di risorse idriche, che ha una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021.

Non mi dilungo sulle finalità, che sono già state toccate da altri colleghi, e sulle modalità con le quali potrà essere fruito il *bonus*, ma voglio sottolineare che questa misura rientra in una visione più ampia della sostenibilità e del risparmio delle materie prime. Accanto all'importante misura del superbonus per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, l'efficientamento idrico è l'altro indispensabile tassello. In qualunque settore si operi, interpretare il *green new deal* europeo è un passaggio che deve vedere impegnato lo Stato, ma anche il sistema produttivo del Paese, rappresentando questa sfida anche una straordinaria opportunità. Ogni cittadino europeo è chiamato a fare la sua parte in questo senso è un contributo esponenziale quello che gli imprenditori possono offrire all'ambiente grazie all'applicazione della ricerca nei loro prodotti. Soprattutto a causa di quest'anno complicato che sta per volgere al termine, possono essere colte importanti opportunità per salvaguardare le risorse del nostro pianeta. Le aziende del nostro Paese sono terze al mondo per produzione di rubinetteria, quindi l'opportunità che viene data ai cittadini con il *bonus* è offerta anche alle nostre imprese, che grazie alla ricerca e alla tecnologia applicata potranno offrire sistemi importanti per un risparmio idrico che darà all'ambiente notevoli risultati. Voglio fare poi un accenno da ex sindaco sulle misure introdotte per i Comuni. Oltre al rinnovo di alcune misure che riguardano la contabilità, oltre alla possibilità di usare ancora avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti, c'è anche il rafforzamento di una serie di fondi, a partire dal fondo di solidarietà Credo che ai sindaci non si dica mai abbastanza grazie per il lavoro svolto: sono la prima linea, il *front office* dello Stato e qualsiasi misura noi adottiamo, qualsiasi intervento noi facciamo, alla fine è quasi sempre a loro che i cittadini si rivolgono per avere spiegazioni, per poter accedere alle misure stesse che noi offriamo. Credo che questa sia anche l'occasione per dire loro grazie per l'impegno che li ha visti protagonisti loro malgrado in questo anno difficilissimo. Credo che come Assemblea potremmo davvero cogliere l'occasione trovare una modalità per dire un grazie sentito e importante al loro impegno in questo anno speciale. dicendo che Italia Viva ha contribuito con propri emendamenti e con il confronto interno alla maggioranza e con l'opposizione a migliorare la manovra. Siamo quindi soddisfatti dell'impianto complessivo della legge di bilancio e delle misure ivi contenute.

prendo in prestito, per iniziare questo mio intervento, la dichiarazione autorevole di un collega di questa Inizio della citazione: «Siamo in mano ad una banda di cialtroni incompetenti, che prima impediscono al Senato di discutere la legge di bilancio e poi si cospargono il capo di cenere». Era il 29 dicembre 2018, esattamente due anni fa oggi, e il collega era Andrea Marcucci, il Presidente del mio Gruppo parlamentare e il riferimento era ad una modalità che è esattamente quella che oggi si ripete in quest'Aula, vale a dire la scelta di comprimere a tal punto il dibattito parlamentare da non consentire a questo ramo del Parlamento di aprire, discutere, emendare, modificare la legge di bilancio. Di fronte a quella scelta, noi ricorremmo alla Corte costituzionale.

tantomeno con i colleghi del Partito Democratico o di Italia Viva o dell'attuale maggioranza, e nemmeno aver elementi di attacco sulle scelte. Vorrei solo porre una questione, ormai gravissima e ineludibile, che ci riguarda tutti, legata allo svuotamento, che io arriverei a definire svilimento, dell'attività parlamentare in una democrazia già fragile e compromessa come la nostra. Temo che stiamo tutti sottovalutando quanto sta accadendo. Non è compito mio giudicare il cambiare idea di fronte a medesimi comportamenti a seconda di chi quei comportamenti mette in atto. Come non è compito mio giudicare chi oggi, dalla maggioranza, denuncia derive giustizialiste e assistenzialiste, dopo aver consentito a questo Governo di porle in essere. essere. Oggi scopriamo che c'è la deriva giustizialista, ma la prescrizione poteva essere fermata da questo Governo. il reddito di cittadinanza è un provvedimento disastroso (non parole mie, ma di membri di questa maggioranza), ma non è stato modificato in questa legge di bilancio. Potevate fermare l'emendamento della senatrice Lezzi sull'Ilva, ma non l'avete fatto. Oggi vedo, con grande interesse, lanciare *ultimatum* sull'utilizzo del MES, che è disponibile da giugno. È giusto avere i propri tempi per maturare *ultimatum*, ma è disponibile da giugno e siamo a dicembre. siccome non è mia intenzione fare un intervento tutto sulla polemica, voglio riprendere le parole con cui Michele Ainis, che studia e conosce la Costituzione forse meglio di quanto non l'abbia fatto io, ha denunciato e ha descritto questa legge di bilancio: «Un coacervo di misure senza disegno, dal *bonus* rubinetti al finanziamento di un *master* in medicina termale; lenzuolate di norme sconnesse l'una dall'altra, in un linguaggio arcano, mutevole come gli umori di un fanciullo». Ancora Ainis: «Perché in nome dell'emergenza sanitaria ogni autorità costituita dispensa in lungo e in largo i propri editti, senza mai curarsi del quadro complessivo. Perché questa emorragia di norme e di decreti scorre perlopiù al di fuori delle procedure stabilite, ferendo il senso della legalità, se non anche il buon senso». Ancora Ainis: «I senatori dovranno votare ad occhi chiusi questa legge, altrimenti si aprirebbe l'esercizio provvisorio del bilancio. Tuttavia, quest'ultimo - l'esercizio provvisorio è pur sempre una eventualità regolata dalla Costituzione, mentre il sequestro del Senato no, quello non è previsto. Non viene autorizzata in alcun modo la confisca dei poteri spettanti al Capo dello Stato». Spero che leggiate queste parole, non come elemento di polemica, ma come un problema che riguarda tutti noi circa le istituzioni che consegniamo al futuro di questo Paese. è poi il merito, e qui mi voglio rivolgere, con rispetto, anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, portatori di una modalità di fare politica (perlomeno questi erano gli intenti) al di fuori delle mance, degli scambi delle reciproche convenienze. Ma vi pare possibile portare così in superficie, come fatto in questa occasione, una logica di scambio e di mance? Non voglio utilizzare altri termini, signor Presidente, perché non utilizzo parole non consone a quest'Assemblea. Da questo punto di vista, anche qui, affinché non giunga una strumentalità delle mie parole, voglio utilizzare quelle di Sabino Cassese di oggi. Inizio della citazione: Decine di elargizioni e mance. L'istituzione di molti fondi. La previsione di finanziamenti fino al 2036, così parcellizzando il bilancio, irrigidendolo. Sono numerosi periodi, che contengono sei o più rinvii ad altre leggi. Secondo una consuetudine, vi erano risorse assegnate alla gestione parlamentare, quelle usate dai Governi per tacitare le voci più critiche delle opposizioni». Ancora Cassese: «Ora, il dialogo Governo e opposizioni è utile, anzi necessario, ma non se si svolge a danno del Paese, che ne paga il costo». Signor Presidente, penso che abbiamo perduto un'occasione. C'erano 800 milioni, che sono diventati addirittura di più; avremmo dovuto prendere ciò che tutti sottolineiamo nelle dichiarazioni e nelle iniziative pubbliche, l'emergenza e la carenza del personale sanitario e dei medici, e fare una scelta forte come Parlamento. Sappiamo che mancano e mancheranno medici nei prossimi anni; superare definitivamente l'imbuto formativo, cioè quei 9.000 laureati che ogni anno in medicina non hanno accesso alla specializzazione, costa 234 milioni di euro all'anno per cinque anni (altro che 800). Potevamo garantire agli italiani un servizio sanitario all'altezza e invece gli abbiamo garantito i *bonus* per i rubinetti e i sanitari. Ora ci aspetta un Capodanno di tregua; poi, così come accaduto per il Natale, tornerete a proporre agli italiani questo indecoroso spettacolo della crisi che non è una crisi, di una verifica che non finisce mai, di un rimpasto che nessuno vuole, ma senza il quale non si prosegue. Non so se è esaurita la fiducia in questo Governo; so che è esaurita la dignità di questo Governo. E non pensate che alla mancanza delle azioni possiate supplire con il proliferare delle definizioni. Non serve a nulla definirsi il partito della Costituzione a parole, se ci si rende complici dello svilimento della Carta. Non serve a nulla definirsi il partito del lavoro, se l'unica cosa che si rafforza è uno strumento dagli effetti devastanti come il reddito di cittadinanza. Insieme a Carlo Calenda abbiamo dato vita ad Azione proprio per questo: un lavoro tenace e coerente, che non ceda alla facilità di dichiarazioni che non costano nulla, a fronte di gesti che producono il contrario, perché questo è il tempo della svolta, di una svolta vera. Le sfide che abbiamo davanti (il sostegno alle famiglie e alle imprese, il piano vaccini) impongono che a questo teatro, a volte dell'assurdo e a volte dell'autoreferenzialità, si sostituisca un'assunzione di responsabilità e serietà che il Paese non può più attendere.

l'urgenza e il dovere di dare risposte e di costruire certezze per uscire dalla crisi: è il senso di questa legge. In queste settimane c'è in gioco molto del nostro destino, come nazione e come democrazia; passa dalla capacità che avremo di iniziare a costruire davvero un nuovo modello di sviluppo, innanzitutto con le infrastrutture sociali, che sono un formidabile moltiplicatore di crescita e di eguaglianza: diritto alla salute, diritto allo studio, qualità del lavoro, redistribuzione di ricchezze e opportunità, oggi sempre più concentrate nelle mani di pochi. È necessario costruire legami e costruire società, perché da soli non siamo nessuno e non andiamo da nessuna parte, come questi mesi hanno insegnato. E non c'è Italia senza una grande sfida collettiva, in particolare in questo tempo che viviamo, che non è un tempo qualunque. Servono progetto e visione; questi sono compiti innanzitutto della politica, è quanto devono dimostrare di saper avere le forze che hanno dato vita a questo Governo. La capacità di dare risposte alla crisi sociale ed economica è un pezzo decisivo della gestione della pandemia. Le cose sono connesse; per questo non bastano interventi d'emergenza, per questo serve un grande piano strutturale di investimenti per la ripartenza. Pertanto, questa legge deve servire a metterci nelle condizioni di utilizzare al meglio e con coraggio i fondi del Next generation dell'Unione europea, per cui l'Italia si è battuta con successo, riaffermando concretamente le ragioni dell'Europa del lavoro e della solidarietà. la crisi sta mettendo a rischio interi territori; mette a rischio le nostre Regioni, quelle del manifatturiero e del *made in Italy*, del valore artigiano dell'impresa diffusa, che è tutt'uno con la vita In questa legge ci sono interventi importanti che abbiamo voluto per rafforzare le aree di crisi industriale, quelle sulle quali abbiamo lottato per istituirle, al fine di proteggere i nostri distretti. Ci sono interventi fondamentali fondamentali per lo sviluppo economico e il rilancio delle Regioni del cratere sismico. In particolare c'è uno strumento, il nuovo contratto di sviluppo, con uno stanziamento di euro, che saranno subito a disposizione anche per le imprese delle aree di crisi che più stanno soffrendo, come quelle del calzaturiero. Chiediamo con forza che le misure per il taglio del costo del lavoro, previste per le Regioni del Sud, vengano estese strutturalmente a tutte le aree di crisi industriale delle Regioni colpite dal terremoto del 2016, per ridare fiducia a chi fa impresa, perché il nostro manifatturiero, il nostro lavoro operaio, il nostro artigianato sono decisivi per il nostro futuro. Di futuro parla tanta parte del disegno di legge al nostro esame e in particolare l'investimento per il diritto allo studio: ogni borsa di studio in più è un pezzo di futuro che si ricompone. Penso alle risorse per ampliare la *no tax area* e per far tornare ad iscriversi all'università i figli delle famiglie in difficoltà. Tra le norme sulla scuola ce ne sono alcune che hanno un valore speciale, ovvero quelle che rafforzano il Fondo contro le diseguaglianze e per il contrasto alla povertà educativa, per potenziare la scuola dell'infanzia e per i percorsi da di interventi vitali, per impedire che i costi della pandemia si scarichino sui bambini più deboli e tolgano loro il domani, in un Paese come il nostro, in cui la dispersione e gli abbandoni scolastici sono quasi il doppio rispetto alla media europea.

La vera rivoluzione dovrà essere quella che prevede di ridurre il numero degli alunni nelle classi, aumentare il numero dei docenti, estendere il tempo scuola e il tempo di apprendimento, innovare la didattica per dare risposte ai bisogni degli studenti, affrontare il nodo del precariato, cambiando un sistema che è ingiusto e mortifica l'insegnamento. Affrontare il nodo del precariato è ineludibile per la riapertura in sicurezza è decisivo per il rilancio della scuola dell'inclusione e, signor Presidente, è decisivo per dare forza ad una nuova leva di docenti e dare riconoscimento al mestiere più bello e più importante. investire nella funzione civile degli insegnanti e nella voglia di futuro degli studenti, perché entrambi, insegnanti e studenti, rappresentano al meglio i valori della nostra Repubblica. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

con DPCM in ordine sparso, aperture e chiusure contraddittorie, decreti in sequenza, scuole e banchi, con il problema dei trasporti che non è stato risolto, perché non ci si era accorti che le scuole sarebbero ricominciate in autunno,

un po' come per i militari al fronte. I militari al fronte che fuggono sono disertori e vanno trattati come tali. *(Applausi)*. Se il personale pubblico si rifiuta di fare i vaccini è disertore e va licenziato: non deve esserci altra valutazione e nessuna discussione.

con continui scostamenti di bilancio e misure frastagliate, senza alcun legame con un disegno logico. Cosa c'è Una importante associazione dei consumatori ha detto che il risultato del tutto saranno 862 euro in più a famiglia per ogni anno.

di euro per il fondo autonomi senza cassa è importante, ed è venuto con un emendamento dell'opposizione alla Camera. *(Applausi)*. Ma la questione seria è che un Governo che ha una visione del Paese non avrebbe lasciato a un emendamento dell'opposizione alla Camera un tema come questo;

la riforma fiscale, si prevede uno stanziamento di 8 miliardi, che poi vengono in parte assorbiti dall'assegno unico. Non ci sono soluzioni per tutto il resto: si proroga il blocco dei licenziamenti aspettando il colpo finale, perché arriveranno tutti assieme.

perché anche la parte di sovvenzione va restituita. Questo è da ricordare. Concludo. C'è un unico filo logico, contro chi produce. Per distribuire il reddito, in qualche modo qualcuno lo deve produrre. Si fa assistenza e nessuna selezione di spesa. Non è credibile. L'Ufficio parlamentare di bilancio, che è già stato citato, ha definito la legge di bilancio un coacervo di misure senza un sottostante disegno politico.

come siamo arrivati qui? Siamo ad uno degli ultimi atti di questa commedia - così pensavo qualche giorno fa - e invece non è una commedia, bensì una tragedia, perché stiamo parlando di un periodo drammatico

in quel caso ci fu anche una terza lettura perché la seconda lettura che facemmo noi portò comunque dei cambiamenti che dovettero essere poi ratificati dalla Camera, quindi non confrontiamo cose che non sono confrontabili. ricordiamo gli strappi che vengono fatti regolarmente a Costituzione e Regolamenti. L'utilizzo della fiducia, quindi uno strumento di emergenza, per

oltre alle costanti tensioni interne alla maggioranza. Tutto ciò ha portato a una tempesta perfetta. Consideriamo però anche la propaganda di regime, che ricorda un po' l'Istituto Luce del Ventennio e segue tecniche comunicative da *reality*. Non voglio dimenticare gli Stati Generali in perfetto stile Luigi XIV. E cosa dire della comunicazione voluta dall'Europa sul V-day: cerimonie simboliche, televisione *non stop* sul tema, dalla mattina alla notte, veramente h24, con commozione, interviste e fasce tricolori su tutti i canali. Questa era stata decisa dall'Europa ma in Italia abbiamo voluto, anzi avete voluto fare ancora di più, una pomposità incredibile. Io penso che tutti vogliamo uscire da questa emergenza ma non sarebbe più serio e sobrio cominciare a vaccinare in modo organizzato e continuativo e comunicare i numeri delle vaccinazioni fatte? Forse è una mentalità un po' lombarda ma guardiamo al pratico. Noi vogliamo che più persone, soprattutto partendo dai soggetti fragili e dagli operatori, siano vaccinati con regolarità, senza scene, con serietà e continuità nell'azione. Questo vorremmo. Parlando del Covid, forse un giorno qualcuno - riprendo un altro tema del quale non abbiamo più parlato - scriverà il libro «L'importanza della plastica ai tempi del Covid» perché ricordo in quest'Aula che tanto vuole fare per l'eliminazione della plastica, che forse, in questo periodo, la plastica è stata essenziale. Ricordiamocelo. Quello che è certo è che il Governo naviga a vista e vi dirò che le persone, là fuori, lo stanno capendo perfettamente. Durante i pochissimi giorni che ciascuno di noi ha avuto per dedicarsi a qualche giro nella propria città per qualche spesa,

In Alta Lombardia ci sono tantissimi imprenditori tessili, alcune aziende sono davvero di eccellenza, e l'azienda di cui vi parlo è incredibilmente solida, quindi la famiglia proprietaria è molto ricca, molto solida, appunto, sta pensando con grandissima angoscia al momento in cui dovrà licenziare il suo personale. Sono quelle famiglie che hanno avuto l'azienda tramandata di padre in figlio, ma anche il personale si tramanda di generazione in generazione, e la terza generazione che attualmente vi lavora si sa se rimarrà. Ma non parlo solo della mortificazione, della rabbia, del dispiacere, perché il vero imprenditore sa che il personale è la sua più grande ricchezza. Non è solo questo; è anche rendersi conto che ci saranno famiglie in difficoltà, che ci sarà una perdita, un pezzetto in meno di capacità professionale, di quell'arte del costruire, del fare, che rende l'Italia un Paese straordinario. Tutto questo è angosciante. Prima

ha lasciato l'Italia perché non considera più questo Paese in grado di garantire il fare impresa. Questo è assai preoccupante e dovrebbe far ragionare anche qualcuno che pensa solo sia sia importante incrementare il finanziamento del reddito di cittadinanza piuttosto che sostenere quelle imprese piccole, medie e grandi che cercano di continuare a produrre e a rendere grande e solido questo Paese sotto il profilo finanziario ed economico. Davvero è incredibile vivere questo momento; non pensavo di votare una legge di bilancio in questo modo. È successo.

sulla manovra ci sono due posizioni: la maggioranza elogia i punti forti, le opposizioni attaccano sostenendo che sia fatta di mancette, misure che rendono il provvedimento un coacervo di interventi senza senso. A me piace parlare di fatti, non di opinioni. Ritengo che fare politica sia qualcosa di più che attaccare dicendo mezze verità, nascondendo l'altra metà, cercando solo di portare acqua al proprio mulino. Passiamo troppo tempo a smentirci l'un l'altro, rischiando figure non edificanti di fronte agli italiani, ai quali non interessano le beghe di Palazzo, ma attendono solo che la pandemia finisca per poter riprendere una vita normale, riaprire i negozi, viaggiare, tornare in classe con compagni e insegnanti, Tra le situazioni più drammatiche, di cui, purtroppo, sono testimone in prima persona, c'è quella della solitudine, vissuta da tutte le persone ricoverate. Per quanto tutti noi apprezziamo lo sforzo e la sensibilità con cui il personale dei vari ospedali cerca di prendersi cura dei nostri cari, tutto questo non può mai sostituirsi alla vicinanza o all'affetto della propria famiglia. Anche la personalità più forte, vedendosi smarrita e senza certezze, rischia di lasciarsi andare, e non tutte, purtroppo, hanno o hanno avuto la forza di reagire. Ma torniamo alla manovra. Possiamo dire che per quest'anno è la quarta legge di bilancio, almeno per quanto riguarda lo sforzo di miliardi di euro messi nel piatto: cura Italia, rilancio, rilancio-*bis*, per 100 miliardi totali, e ora questa legge di bilancio con 40 miliardi Parti delle opposizioni non parlano dei grandi numeri approvati con il disegno di legge di bilancio in esame e preferiscono concentrarsi sulle misure che definiscono mancette, sostenendo che tutta la manovra sia una mancetta. Possiamo veramente definire mancette alcune misure? Magari sì, magari qualcuno dei parlamentari ha presentato e si è visto approvare emendamenti del genere da uno, cinque o dieci milioni di euro. Se lo ha fatto per ingraziarsi i cittadini del proprio collegio elettorale ha fatto una cosa deprecabile a mio avviso, che si tratti di opposizione o anche di maggioranza. Ma, se con quelle cifre si pone rimedio a una situazione che riguarda un ristretto ambito economico che afferisce a una parte della popolazione italiana, io allora non ululerei alla luna, ma guarderei tutto sistema nel complesso. Solo considerando i macrotemi ci rendiamo conto di come questa sia tutt'altro che una manovra di mance e mancette.

3,3 miliardi per la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale; 24 miliardi nel triennio per il Piano nazionale transizione 4.0; un miliardo per l'anno bianco contributivo di autonomi e partite IVA; un miliardo aggiuntivo per il Fondo sanitario nazionale, un miliardo per far fronte la campagna vaccinale con l'assunzione di 3.000 medici e di 12.000 infermieri; 3,7 miliardi nel triennio per la scuola; 1,1 miliardi per il credito d'imposta per il Mezzogiorno, oltre a 6 miliardi nel 2022 per il superbonus e mi fermo alle cifre che superano il miliardo di euro. Altro che mance o mancette! Onestà intellettuale dovrebbe portare ad ammettere che si tratta di interventi corposi e organici che toccano tutte le fasce della popolazione. Con l'assegno unico universale aiutiamo le coppie ad avere figli, cercando di invertire il calo della natalità di cui soffre l'Italia, mentre con l'esonero parziale dei contributi si supportano i piccoli imprenditori autonomi e i liberi professionisti, specie quelli giovani, che sentono in maniera particolare il peso di questa contribuzione. Con i fondi sulla sanità supportiamo ancora di più il sistema della salute in questo Paese. Vorrei ricordare che, a fronte di tagli lacrime e sangue operati nel precedente decennio per circa 37 miliardi, da quando il MoVimento 5 Stelle è al Governo sul settore della sanità sono stati messi 13 miliardi in più Con i fondi per la riqualificazione energetica e l'estensione del superbonus rimettiamo in moto l'economia senza consumare il suolo. Questa misura è formidabile e, seppur da migliorare, ha già fatto registrare un'impennata dei lavori di media dimensione, con una distribuzione geografica a macchia di leopardo e ciò significa che lavorano le piccole e medie imprese in tutto il Paese. Come si fa a non vedere l'unitarietà della legge, che tocca i segmenti vitali del nostro Paese: famiglia, piccole imprese, autonomi e partite IVA, il sistema sanitario? Questo significa che tutto un circolo virtuoso dell'economia può ricominciare a crescere. Credo a questo punto di aver dimostrato che il principio paretiano, la cosiddetta legge 80/20, è ampiamente rispettato dal presente disegno di legge di bilancio e soprattutto che è pretestuoso estendere all'intero provvedimento il commento che si potrebbe fare per una, dieci, cinquanta misure che valgono una piccola parte dell'intera manovra.

Sono circa 2.200 persone che hanno lavorato per la CRI, chi nel settore amministrativo chi in quello operativo; poi è intervenuto il decreto legislativo n. 178 del 2012, che a mio avviso ha riorganizzato in maniera disastrosa la Croce Rossa italiana, mettendo in mobilità i dipendenti e spostandoli in altre amministrazioni dello Stato, creando un ente strumentale in liquidazione (la cosiddetta Esacri) e una nuova associazione della Croce rossa italiana, privata, che però continua a ricevere sussidi dallo Stato.

Con l'aiuto del personale coinvolto nella suddetta problematica (che ringrazio), ho proposto un emendamento al decreto-legge agosto, risultato però inammissibile per materia. Tale proposta ha però riscontrato l'interesse del presidente dell'INPS Tridico, il quale ha preso a cuore quell'assurda situazione che con il provvedimento in esame So che altri stanno mettendo il cappello sopra questa misura; non mi interessa se abbiano davvero lavorato ora alla risoluzione del problema o meno. So solo che prima non l'hanno fatto e che, prima del mio emendamento e dell'apprezzamento del presidente Tridico, di voler risolvere questa situazione non c'era traccia né alla Camera né al Senato. Magari è solo una coincidenza che sia finita ora nell'articolato. Questa problematica, che ha suscitato grande scalpore, avrebbe dovuto essere risolta prima che giungesse anche all'attenzione dei noti programmi televisivi. Sono contento che finalmente si riesca a mettere ordine a un pezzetto della storia della Croce Rossa. Rossa. Andiamo avanti con la convinzione di fare il bene del Paese e ricordiamoci che non esiste una ricetta perfetta o una legge di bilancio perfetta, specie in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, ma che se la maggior parte della legge ha una sua organicità - e credo di averlo dimostrato - allora il Paese sta ricevendo lo strumento che serve per ripartire. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Ai sensi dell'articolo 129, commi 2 e 3 del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Dopo la votazione degli articoli della seconda sezione, si procederà alla discussione dell'articolo 1 del disegno di legge. Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge. Passiamo, dunque, all'esame della seconda sezione del disegno di legge (articoli da 2 a 20). Poiché non sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli da 2 a 20, si procederà direttamente alla votazione degli articoli.

Dichiaro chiusa la votazione

senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, né articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2054 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2054, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sulla fiducia avrà inizio domani, alle ore 9.